Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano", La relatrice, senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

interviene in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. La Commissione giustizia ha discusso l'Atto Senato 824 congiuntamente ad altre proposte di legge di legge (gli Atti Senato 163, 245 e 475), che, in seguito all'approvazione dello stesso, adottato come testo base, sono stati dichiarati assorbiti. Per l'istruttoria legislativa, la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali e ha dato spazio a un ampio dibattito sul tema. Di ciò ringrazio la presidente Bongiorno e i colleghi della Commissione che hanno dato il loro contributo alla discussione, consentendo di esaminare approfonditamente la complessa questione. Nel merito, il provvedimento modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque la metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a 1 milione di euro. Il disegno di legge in esame aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 12, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano riferibili al delitto di surrogazione di maternità anche se poste in essere in territorio estero, con conseguente applicazione delle pene previste dal primo periodo. La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista a determinate condizioni dall'ordinamento penale italiano. Il disegno di legge si propone così di contrastare quell'odioso fenomeno noto come turismo procreativo, per il quale molte coppie si recano all'estero per ricorrere a pratiche di maternità surrogata eludendo il divieto imposto dalla legislazione. Sulla maternità surrogata occorre rammentare che si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021, ha sottolineato che questa pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Con tale pratica, infatti, si compie la frantumazione della maternità, che viene divisa in tre parti: una donatrice di ovociti, una madre gestazionale e dei genitori committenti che poi si occuperanno del nuovo nato. Ma la domanda è: chi è la vera madre? E non è una domanda oziosa, perché il figlio ha diritto alla propria identità, a conoscere da dove e da chi proviene. Un figlio che, nel momento in cui viene tolto alla madre che lo ha partorito, interrompe per sempre il dialogo biochimico intercorso con lei durante la gravidanza, a tacere della violenza dell'atto stesso di togliere il figlio appena partorito a colei che per nove mesi lo ha portato in grembo. Non solo. La maternità surrogata offende irrimediabilmente la donna, il suo corpo per natura potente, che viene ridotto a una macchina da riproduzione, a mera incubatrice. Scinde drammaticamente la donna dalla maternità e la donna viene separata dal potere più grande: dare la vita a un nuovo essere umano, il potere più grande che si possa immaginare. La maternità surrogata è sanzionata penalmente nel nostro ordinamento, è vero, ma la norma viene facilmente elusa da coppie che si recano in Paesi in cui tale pratica è consentita, con il risultato di rendere inefficace la disposizione di legge. Di fronte a ciò il legislatore non può essere acquiescente e, se è necessario fare una nuova legge per far funzionare una legge preesistente, deve attivarsi, soprattutto quando il bene da tutelare è la dignità umana.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, di cosa stiamo discutendo? Diciamo immediatamente che stiamo discutendo non dell'introduzione dell'introduzione di un ennesimo reato per una condotta comunque non prevista nello Stato italiano. Nello Stato italiano la questione della cosiddetta GPA è già prevista come reato. Stiamo discutendo del fatto di rendere universale questo tipo di condotta. è una norma viziata sotto il profilo della ragionevolezza (è assolutamente irragionevole e spiegheremo perché) ed è totalmente disallineata rispetto alle pronunce della Corte costituzionale, che si sono occupate di quello di cui ci saremmo dovuti occupare noi, ma che invece non colposamente, bensì dolosamente, si evita di affrontare, cioè il problema della tutela dei minori, che è stato invece affrontato da numerose pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione a sezioni unite civili. civili. Siamo di fronte - e in questo obiettivamente c'è una coerenza - all'ennesima norma di carattere penale identitaria e ideologica, viziata anzi da un furore ideologico.

sembrerebbe superfluo sottolinearlo - sono reati universali perché, quanto a gravità, percezione e configurazione, sono in maniera indiscutibile percepiti come tali a livello internazionale: crimini di guerra, pirateria, tortura, genocidio. Evidentemente non stiamo parlando di questo, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che invece la

decisamente bassa. Di talché per questo tipo di reati le altre eccezioni previste sono quelle che riguardano la lesione di interessi fondamentali e diretti dello Stato. E anche qui non siamo assolutamente in questo campo, né si richiami, se si vuole argomentare, su una natura pubblicistica dell'argomento che stiamo trattando: la lesione diretta di interessi dello Stato non corrisponde e non è sovrapponibile a una natura pubblicistica. Ma vi è di più; la normativa in cui si inserisce

di certe condizioni: almeno una parte della condotta si sia verificata in Italia e su questo c'è giurisprudenza amplissima che la amplia molto; una richiesta del Ministero della giustizia (a piè pagina si registra un solo caso su questo argomento in cui il Ministro della giustizia abbia fatto questo tipo di richiesta, a testimonianza di quanto sia rilevante e di quanto sia necessario prevedere questo tipo di universalità); la doppia Ciò per giurisprudenza pacifica ovvero, e torniamo al punto di partenza, che sia previsto anche negli altri Stati. Siamo quindi completamente fuori dall'ordinamento nazionale, dalle convenzioni, dalle eccezioni già previste, dai principi generali che ci richiamano al principio di ragionevolezza,

il costante atteggiamento della maggioranza quando approccia al diritto penale. Potremmo fare un lungo elenco dell'introduzione di reati dall'inizio della legislatura. L'aspetto più grave è che molti di questi reati già esistono in Italia; li si ripropone *(Applausi)* o sotto forma di aggravanti o sotto forma di

su temi che dovrebbero essere affrontati collettivamente da tutto il Parlamento, in quanto temi che oggettivamente ci interrogano, o su esigenze che vengono sottolineate in maniera quasi normativa dalla Corte costituzionale, la maggioranza tira fuori una riedizione di reati, un *restyling* di condotte già punite, ovviamente peggiorando e creando una grande confusione. Qual è lo scheletro? Lo scheletro è che comunque tutte le pronunce, anche quelle che su questo argomento hanno espresso un giudizio e una valutazione più restrittiva quanto al bilanciamento dei beni in discussione, lasciano emergere un concetto chiarissimo: bisogna tutelare lo stato giuridico dei minori, di questi bambini. *(Applausi)*. Lo dicono tutti e, da ultimo, l'ha detto la Corte costituzionale. si potrebbe partire dalla condivisione di questo concetto e di questa esigenza? Con questa norma di fatto non solo volete evitare di affrontare questo argomento, ma pensate di perseguire un'impostazione molto ideologica rifacendovi sui bambini. Non è una terminologia molto elegante quella che sto usando. Non soltanto evitate l'argomento, ma penalizzate la tutela dei minori che ci è stata chiesta da tutte le pronunce e soprattutto dalla Corte costituzionale. Facciamocene una ragione, cari colleghi: la Corte costituzionale, che non è un organo politico, è esattamente a presidio di quei principi stabiliti dalla nostra Carta costituzionale, interpretando e applicando la quale, soprattutto nell'inerzia di questo Parlamento, si cerca di affrontare, nella rispondenza dei principi che sono a tutela di tutti, i cambiamenti che ci sono nella società.

Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824.

«Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». E la legge italiana, al comma 6, prevede che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Obiettivo, dunque, della vostra proposta è la perseguibilità del cittadino e della cittadina italiani anche nei casi in cui la surrogazione di maternità sia praticata all'estero. Spieghiamolo ancora meglio: un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile al rientro in Italia, a prescindere dal fatto che quel comportamento è invece perfettamente legittimo nello Stato straniero. Qui si pone il primo problema: la punibilità di un reato comune - perché di reato comune parliamo - commesso da un cittadino italiano all'estero è subordinata al principio di doppia incriminazione, che rappresenta un requisito imprescindibile per la punibilità, nonché uno strumento di regolamento dei rapporti internazionali tra Stati (reciprocità). Secondo la comune accezione - si badi bene - costituiscono oggi reati universali quelli percepiti come tali a livello globale, ossia i crimini di guerra, la pirateria, la tortura, il genocidio, tutti reati puniti con pene molto alte, naturalmente, fino all'ergastolo. Se aveste, dunque, un minimo di onestà intellettuale e anche di senso giuridico, il vostro intervento andrebbe letto in combinato disposto con il nostro codice penale che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, infatti prevede che qualsiasi delitto comune punito con una pena inferiore ad un minimo di tre anni - e qui la pena va da tre mesi a due anni è punibile se commesso all'estero a istanza o querela di parte, ma anche a richiesta del Ministro della giustizia. Ora, non risulta che mai, da quando questa legge è in vigore, ossia da vent'anni, alcun Ministro della giustizia abbia fatto tale richiesta, men che meno l'attuale ministro Nordio. Un filino di ipocrisia, forse, nel vostro intervento? Forse la necessità di dare in pasto ad un Paese affamato e disgregato un provvedimento bandiera, l'ennesimo, e un nemico contro cui puntare il dito e da odiare? Il sospetto è lecito, ma più che un sospetto è una certezza. Andando avanti. L'irragionevolezza dell'intervento la si coglie anche analizzando nel concreto come la norma vada ad inserirsi all'interno del sistema penale. Da un lato, infatti, la disposizione è volta a creare una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma dall'altro siamo di fronte ad una sanzione sostanzialmente bagatellare, che sarebbe peraltro totalmente priva di effettività. Essendo la pena prevista da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, come abbiamo ricordato, essa non consentirebbe la punibilità in concreto della persona, in quanto sarebbe possibile l'applicazione di molteplici istituti, come la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale, la messa alla prova. Da ciò deriva la contraddizione del vostro intervento: da un lato abbiamo un nome roboante (reato universale), dall'altro una pena minima e sostanzialmente inapplicabile. In pratica, si tratta di una misura spot che mette completamente a nudo la vostra cattiva di fronte a un provvedimento bandiera inefficace nella pratica, ma ottimo per fare propaganda sulla pelle delle persone e, quel che più ferisce, per fare propaganda sulla pelle dei più indifesi: i bambini e le bambine nati sì nati sì grazie a questa pratica, ma non da questa pratica, perché sono nati, come tutti i bambini e le bambine voluti e desiderati, da un progetto d'amore e di famiglia. Andiamo avanti perché davvero, paradossalmente, il vostro disegno di legge è discriminatorio nei confronti degli italiani - i grandi patrioti - perché opera due pesi e due misure a seconda della nazionalità di chi lo commette. Ci troviamo quindi di fronte al paradosso che una coppia di nazionalità diversa - poniamo il caso lei italiana e lui canadese - si reca in Canada, dove è perfettamente legale, legittimo e normato accedere alla pratica di surrogazione della maternità;

A voi non interessano le coppie etero, che sono però il 90 per cento di quelle che accedono alla pratica della maternità surrogata; a voi interessa soltanto colpire le coppie omogenitoriali, soltanto colpire le famiglie arcobaleno, che nella vostra visione di società devono sparire, e per fare questo siete disposti a coprire di ridicolo e ignominia anche le istituzioni più alte della Repubblica. *(Applausi)*. Tuttavia, l'ipocrisia dalla vostra sbandierata pretesa della difesa delle donne e della nostra dignità si disvela completamente qui. Avreste avuto lo strumento giuridico idoneo (e noi ve l'avevamo anche suggerito), se davvero voi aveste voluto incriminare la coercizione, ossia l'obbligo a portare avanti una gravidanza per altri, laddove la donna fosse costretta. Gli articoli 600 e 601 del codice penale prevedono, infatti, proprio la punizione dei casi di costrizione, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. presentato l'emendamento, ma l'avete bocciato perché a voi non interessa la difesa della donna, anzi soprattutto non interessa consentire che la donna che non voglia portare avanti una gestazione, sia essa per altri o per sé stessa, possa anche interromperla. Anzi, voi state minando alla base e attaccando il diritto all'aborto delle donne, quindi siete favorevoli alla gravidanza forzata. *(Applausi)*. Per questo il Movimento 5 Stelle ha aderito ufficialmente alla campagna «My voice my choice», per dare l'opportunità a tutte le cittadine europee, anche a quelle che vivono in Molise oppure in Polonia, di poter accedere a questo diritto. *(Applausi)*. Veniamo ora all'aspetto più inquietante di questa vergogna universale, che è la conseguenza che questo intervento avrebbe sui minori, sui bambini e sulle bambine. Il pericolo più grande di questo testo di legge, infatti, è che quelle tutele, già lievi, di cui questi minori non godono possano essere addirittura affievolite, andando così in contrasto con tutta un'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale e dei giudici di Strasburgo. Con la sentenza n. 33 del 2021, infatti, la Corte costituzionale ha chiesto al legislatore (a noi, a voi) di trovare un equilibrio, un corretto bilanciamento tra il divieto, oggi vigente, di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e l'imprescindibile necessità di garantire il diritto dei minori ad avere una famiglia, ripeto, una famiglia. La Corte ha indicato nella procedura di adozione nei casi speciali, l'unico strumento oggi disponibile. Tale strumento - ha sottolineato la Corte - si rivela non del tutto sufficiente a garantire l'interesse superiore del minore. Quindi, ogni intervento che vada ulteriormente ad attaccare quella già fragile tutela va in senso direttamente opposto a quello che la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo hanno chiesto.

stralciato dalla Corte costituzionale, in quanto distonico nel nostro ordinamento e distopico dal punto di vista culturale e anacronistico. In conclusione, voglio ringraziare il mio Gruppo e la mia forza politica, il MoVimento 5 Stelle, per essere impegnato davvero in tutte le sedi, dentro e fuori questo Palazzo, per contrastare questo abominio. L'impegno che, come sentirete dai molteplici interventi che mi seguiranno, va oltre quello meramente istituzionale, per diventare un impegno che investe l'umano e incarna il senso più alto del fare politica. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n.

*(Applausi)*. Saluto altresì la segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, dottoressa Filomena Gallo, e tutti i cittadini che assistono a questo dibattito

oggi reato in Italia se attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità. Ciò anche se il fatto è commesso all'estero. La disposizione penale prevede che, ricorrendo questa nuova fattispecie, l'autore sia sanzionato con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 euro a un milione di euro. Il provvedimento ha quindi il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute da chiunque, anche in territorio estero, dirette alla commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità. Si propone, dunque, di rendere universale il reato e, quindi, perseguibile anche all'estero, anche se commesso in Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è pienamente legale. che il nostro sistema giuridico consente l'introduzione di fattispecie penali universali solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato. Questo principio può essere derogato solo in una serie precisa di casi. La relazione di accompagnamento al provvedimento riconduce la GPA, quale reato universale, ai casi contenuti nell'articolo 7, comma 5, del codice penale, quindi in presenza di beni e valori, la tutela dei quali è riconosciuta di interesse dell'intera comunità internazionale. Classici casi sono, ad esempio, il genocidio o il terrorismo. Considerato che sono numerosi gli Stati, anche europei, in cui la GPA è perfettamente legale, è chiaro che ricomprendere tra tali reati la gestazione in altri sia giuridicamente del tutto infondato. Colleghe e colleghi, è pacifica l'assenza di un disvalore universale riconosciuto nella pratica della GPA, che difatti è consentita e pienamente lecita in 65 Nazioni, di cui 6 in Europa. Europa. Non solo numerosi i Paesi non vietano la GPA, ma addirittura la regolamentano e promuovono all'interno dei propri sistemi sanitari. Viene così a cadere il presupposto fondamentale della giurisdizione universale, la presenza di un disvalore comune della condotta sotto esame. Paragonare, colleghi, la GPA a reati come il genocidio, la tortura, lo sfruttamento della prostituzione minorile, la riduzione in schiavitù, è un assurdo giuridico: spero ve ne rendiate conto. Questo provvedimento viola palesemente i principi di ragionevolezza e proporzionalità che permeano l'intero ordinamento giuridico e che, in ambito penale, acquistano una particolare rilevanza a causa della connessione con altri principi, quale quello di legalità, il principio di offensività e quello di rieducazione della pena. Non solo: questo nuovo reato universale, per come è scritto, contrasta con il principio di colpevolezza di cui all'articolo 27 della nostra Costituzione, posto che sembrerebbero essere punibili condotte realizzate da soggetti la cui condotta è pienamente lecita nel Paese nel quale è stata commessa. Aggiungo che intervenire sulla GPA rendendola reato universale non solo è un abominio giuridico, ma è anche un atto di grande disumanità, colleghi, verso quei genitori e quei bambini in carne e ossa ai quali vi ostinate a non voler riconoscere alcun diritto. Infatti, anziché occuparvi di riformare la normativa in tema di trascrizioni e la legge sulle adozioni, che nel 2024 ancora non consente, se non in casi del tutto eccezionali, alle persone singole o alle coppie omogenitoriali di adottare e di introdurre una discussione pacata ed equilibrata che si basi su evidenze scientifiche e non sul pregiudizio su come regolamentare anche da noi la gestazione per altri, voi avete deciso di accanirvi, con l'unico obiettivo di alimentare lo stigma sociale contro le famiglie diverse dall'unica che avete in mente voi. Lo fate in barba alle indicazioni della Corte costituzionale, che più volte ha chiesto al legislatore di intervenire su trascrizione e adozione. Lo fate in spregio ai più elementari principi di diritto.

Signor Presidente, aggiungo la mia voce alla voce delle colleghe che hanno illustrato le questioni pregiudiziali di costituzionalità a sostegno dell'incostituzionalità di questo provvedimento. che la mia prima preoccupazione, non solo riguardo a questo provvedimento, ma alla politica generale del Governo, è che l'articolo 13 della Costituzione, che dice che la libertà personale è inviolabile, sembra venire dimenticato in quest'Aula. Noi, sostanzialmente, in questa fase stiamo lavorando soltanto come Commissione giustizia. Voglio ricordare ai colleghi che ieri in Aula abbiamo approvato

le pene, riscrivere pene e reati su comportamenti che sono già vietati e, quindi, non richiederebbero alcun intervento della maggioranza e del Governo. È evidente che, nonostante gli annunci del È evidente che, nonostante gli annunci del ministro Nordio, che ci aveva promesso il diritto penale minimo, abbiamo superato tranquillamente ogni limite del diritto penale massimo, perché l'unica cosa che fa questa maggioranza è legiferare in norma penale, introducendo reati e pene. Ed eccoci qui stamattina, ancora una volta, con un nuovo reato, che riscrive un comportamento già previsto come illegale ed illecito in questo Paese. Vorrei chiedervi se davvero non c'è niente di più urgente, fuori da quest'Aula, rispetto ad aumentare i reati e le pene. Pensate che aumentare reati e pene serva in qualche modo a gestire le complessità di una società come la società italiana?

per quali numerosi motivi questo è un disegno di legge incostituzionale. Prima di tutto, l'articolo 3 della Costituzione recita che siamo tutti uguali davanti alla legge. Invece che cosa fa questo disegno di legge? Questo disegno di legge ci dice che la GPA è reato universale se la fanno gli italiani, se la fa il nostro gregge, il gregge di Giorgia, che non si deve muovere. Infatti, se la fa Elon Musk, gli si aprono le porte di Palazzo Chigi. o il comportamento è reato universale o il comportamento non lo è, altrimenti non si va a comprare Starlink, e vorremmo anche saperne un po' di più.

che ne sa l'ufficiale dello stato civile di come è nato il bambino? Arriva un signore e dice: «Io e mia moglie abbiamo avuto un figlio in Canada» e l'ufficiale dello stato civile scrive. Se invece ci vanno due papà, l'ufficiale dello stato civile dirà: «Ma come avete fatto questo bambino?». Quindi l'antico principio *nemo tenetur se detegere*, cioè nessuno è tenuto a denunciare se stesso, se ne va a quel paese, senza che noi facciamo la minima piega. All'articolo 10 e all'articolo 11 della Costituzione è scritto che noi vogliamo tenere rapporti armoniosi nella comunità internazionale e che provvediamo a cessioni di sovranità per tenere un ordinamento pacifico e armonico. Invece che facciamo? Mettiamo due dita negli occhi

Vogliamo poi pensare a quanti minuti durerà questa legge davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea? Un minuto. Dato che in questa Unione, nonostante voi, esiste ancora la libera circolazione dei servizi - e la GPA è un servizio sanitario - e delle persone, se io, cittadino italiano, vado in Grecia, dove la GPA è lecita, e non posso accedere a quel servizio, si sta violando la libertà di circolazione dei servizi; se poi, quando torno in Italia, vengo arrestato, si sta violando la libera circolazione

Vogliamo parlare dell'articolo 31 della Costituzione, quello - cari colleghi e care colleghe - che parla della protezione dell'infanzia? Ci siamo dimenticati la protezione dell'infanzia o nella vostra visione progressiva del diritto esistono ancora i figli di serie A e i figli di serie B? *(Applausi)*. In questo Paese - grazie al cielo la differenza vergognosa, medievale tra figli legittimi, legittimati, naturali, eccetera, pensavamo di averla messa nella discarica discarica dei rifiuti della storia. Invece dobbiamo aspettare voi, il Governo Meloni, la sua maggioranza, per sentirci dire che i bambini italiani non sono tutti uguali:

che - vi do una notizia - esistono in questo Paese, vivono, vanno nelle nostre scuole, frequentano altri bambini - grazie al cielo, questo Paese è molto più civile di quanto vuole rappresentarsi qui dentro - e devono essere tutelati. Invece sapete che succede? Tutte le carte che oggi, quando si va a registrare un bambino, si portano in Comune e servono a quel bambino ad avere memoria storica della sua vita personale, non potranno più essere depositate, perché saranno la prova di un reato. Quindi, quel bambino perderà il diritto alla propria memoria storica. Lo capite questo? questo? *(Applausi)*. Poiché ancora questo Paese, unico in tutta l'Europa occidentale, non ha delle norme per riconoscere i bambini

è ovvio che quei bambini non potranno più essere adottati. E allora vi vorrei chiedere se avete per caso in mente di deportarli in qualche Albania di vostra creazione toglierli ai genitori e di darli - che ne so io - ai servizi sociali per essere educati alla moralità meloniana di cui ci state facendo esempio? questa legge non è soltanto anticostituzionale *(Commenti)*, ma è anche un dito in un occhio alla Costituzione repubblicana, come l'hanno pensata i nostri Costituenti. *(Applausi)*. Vi portate la responsabilità di approvare un disegno di legge medievale che fa vergogna a questo Paese.

Signora Presidente, questo disegno di legge vede anche il nostro Gruppo profondamente contrario per tante ragioni, che sono state giustamente ricordate negli interventi precedenti. Il provvedimento interviene Il provvedimento interviene sul tema certamente complesso che riguarda i diritti fondamentali di migliaia di persone e - secondo me e secondo noi - lo fa davvero tentando di ancorare il Paese al passato, a quel Medioevo che ha adesso citato il senatore Scalfarotto, con l'illusione davvero - fatemela dire così - di poter fermare il vento con le mani. Questo disegno di legge pretende, infatti, di sottoporre alla giurisdizione italiana chiunque realizzi una gestazione per altri, ovunque, anche all'estero. Significa - come stiamo capendo e abbiamo capito - punire con pene di reclusione da tre mesi a due anni e sanzioni da 600.000 a 1 milione di euro tutti coloro che si sono recati in un Paese estero e, nel rispetto delle leggi di quel Paese, sono diventati genitori tramite la gestazione per altri. In più, la formulazione è talmente vaga da non permettere nemmeno di comprendere quali condotte il legislatore intenderebbe effettivamente sanzionare. Si tace e non si dice nulla circa chi debbano essere gli autori della condotta affinché gli stessi siano incriminabili e quali caratteristiche debba rivestire la fattispecie, tanto da portare a pensare che la *ratio* che la *ratio* del provvedimento in esame intenda rendere perseguibile finanche il medico di cittadinanza italiana che esegua legittimamente una gestazione per altri in territorio estero, ai sensi della normativa ivi vigente, e successivamente faccia accesso, per motivi personali, nel territorio italiano. Significherebbe insomma - per spiegare quello di cui stiamo parlando - assoggettare alla stessa pena tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa procedura, compresi i medici o gli avvocati: insomma una vera e propria guerra alla gestazione per altri, ovunque nel mondo; come dice spesso la vostra propaganda, "nel globo terracqueo", nemmeno stessimo parlando di reati come il genocidio, il terrorismo o i crimini di guerra. Ora che sia questo un assurdo giuridico mi pare lampante, perché la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia operano soltanto ed esclusivamente per tutelare beni giuridici corrispondenti a interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale, mentre evidentemente il reato di surrogazione di maternità, o meglio la gestazione per altri - anche le parole sono evidentemente importanti - non è oggetto, ovviamente, di convenzioni internazionali

Voi in questo modo intervenite criminalizzando delle scelte di vita, che evidentemente non capite e non volete capire, con un provvedimento - e anche questo è stato giustamente sottolineato dai miei colleghi che non farà altro se non aumentare lo stigma sociale contro bambini e bambine già nati. Nel frattempo, però, omettete di dare attuazione alle direttive precise della Corte costituzionale, quando questa ci dice che la legge sulle adozioni deve essere modificata adottando una disciplina che dia ai bambini nati da GPA maggiori garanzie di quelle offerte dall'adozione nei cosiddetti casi particolari, richiamando la necessità cioè di salvaguardare la proporzionalità della compressione degli interessi del minore rispetto allo scopo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità. Insomma, questa nuova legge inasprirà la perseguibilità della GPA al fine di cercare di dissuadere dal ricorso a tale tecnica di procreazione, omettendo però di rafforzare la tutela dei bambini venuti al mondo a seguito di GPA, come invece chiede la Corte costituzionale. Vale lo stesso identico ragionamento per le trascrizioni, perché, quando impedite di trascrivere gli atti di nascita, realizzate una vera e propria discriminazione. Sarebbero state invece queste le priorità: consentire ai singoli e alle coppie omogenitoriali di accedere sia alle adozioni con procedure semplificate e di consentire immediatamente le trascrizioni dei bambini già nati. Ecco, è esattamente a questo che mi riferisco quando parlo di un vero e proprio tentativo di fermare il vento con le mani. Infatti la GPA - che vi piaccia o meno - è legale in molti Paesi del mondo, alcuni dei quali vicinissimi a noi. Allora l'unica strada percorribile è la regolamentazione, non certo i divieti. Invece perdurate con questa vostra sorta di così - per il panpenalismo, un'impostazione anche in questo caso clamorosamente e totalmente ideologica, con un provvedimento bandiera, un reato nuovo contro ogni cosa che non ci piace, che non facciamo lo sforzo di capire e magari illudendosi di aver risolto il problema, quando invece non sarà così. Il rischio concreto connesso a questo provvedimento è proprio il contrario, cioè che l'introduzione del reato contribuisca - come sempre accade, peraltro, in questi casi - ad incentivare il sommerso, a foraggiare il costoso mercato delle pratiche illegali, con il duplice effetto di aumentare lo sfruttamento delle donne e di porre davvero a rischio la salute della donna e quella dei nascituri, tutti costretti alla clandestinità. Sono discorsi, peraltro, che in questo Paese conosciamo bene perché hanno riempito la storia della nostra nostra vicenda politica in tutti i decenni passati. Quanto al resto, non sarà certo questo provvedimento a fermare il futuro, a fermare l'evoluzione sociale delle famiglie. Voi davvero vi comportate come quello struzzo che mette la testa sotto la sabbia per non vedere come cambiano le cose nel mondo. È stato ricordato dai miei colleghi, che hanno fatto molto bene a dirlo: i bambini e le bambine nate dalla GPA esistono già hanno vite vere, hanno diritti che vanno tutelati. Come è stato ricordato e come ho dichiarato anch'io, è la Corte costituzionale che dice che quei diritti vanno tutelati. Noi non accetteremo che esistano in Italia bambini di serie A A e bambini di serie B. Per tutte queste ragioni, voteremo a favore di tutte le questioni pregiudiziali che sono state presentate. Presidente, Forza Italia voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità, che - a nostro giudizio - appaiono viziate sotto diversi e molteplici profili giuridici e costituzionali. Ho sentito molti interventi di merito, con toni anche propagandistici. Nel mio intervento cercherò invece di concentrarmi sugli aspetti giuridici e costituzionali che - a mio avviso - attengono attengono al tema oggi in esame, con riserva poi di approfondire ulteriormente nel merito il provvedimento, perché farò anche la dichiarazione di voto finale per conto del mio Gruppo. Un primo grave errore, che ho rinvenuto sia nei testi delle pregiudiziali depositate, sia negli interventi delle colleghe e dei colleghi che mi hanno preceduto, concerne la qualificazione giuridica del nuovo reato - errore sul quale peraltro si fonda l'intero assunto delle pregiudiziali presentate - quello del reato universale. Ebbene, colleghi, questo non è un reato universale. La maternità surrogata, con l'approvazione di questo disegno di legge, non diventerà infatti mai un reato universale. Correttamente la nostra relatrice, la brava e preparata senatrice Campione, nella sua relazione non ha mai usato, per la maternità surrogata, il termine di reato universale. Invero, Presidente, secondo la dottrina giuridica, reati universali sono i reati, in genere gravissimi - sono stati ricordati - perseguibili in Italia anche se commessi da stranieri all'estero. esempio, sono reati universali i reati contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra. Parliamo, quindi, di reati commessi all'estero, anche da stranieri, però punibili in Italia. Per fare un esempio di strettissima attualità, invoca un reato universale, in particolare un crimine contro l'umanità, Zelenskij, quando in queste ore chiede al Brasile di arrestare in Brasile Putin, in occasione del prossimo G20 a Rio de Janeiro. Invero nel caso in esame non è così. Con il disegno di legge in esame ci si limita a punire un cittadino italiano che all'estero ricorre alla maternità surrogata, fattispecie peraltro - come già ricordato da tanti intervenuti oggi nel dibattito - già vietata nel nostro Paese. Un cittadino italiano, quindi, non un cittadino straniero; non viene punito lo straniero che all'estero ricorre a tale pratica, se anche poi dovesse trovarsi in territorio italiano. Quindi non viene perseguito Elon Musk - come diceva prima il collega Scalfarotto - e non verrebbe perseguito Elton John, se per caso venisse a trovarsi nel nostro Paese. Non si crea nessun nuovo reato universale. Questo è un punto che abbiamo chiarito. Passiamo al secondo punto sul quale tutti gli interventi in termini giuridici si sono soffermati: la doppia incriminazione. Il reato, cioè, dovrebbe essere previsto come reato anche nello Stato estero dove viene commesso; in caso contrario, la condotta dovrebbe essere scriminata. Anche in questo caso la vostra tesi giuridica non regge. Nel nostro ordinamento sono già previsti come reati comportamenti che appaiono leciti all'estero. Come ho già avuto modo di far notare nella discussione in Commissione giustizia, invito l'Aula a riflettere sul reato di violenza sessuale ai danni di un minorenne. Come è noto, nel nostro Paese l'età del consenso è fissata in anni quattordici; al di sotto di questa età un rapporto sessuale, pur consenziente, configura sempre un reato. Ma l'età del consenso varia da Paese a Paese. Da un semplice approfondimento di diritto comparato, si apprende per esempio che in numerosi Paesi, soprattutto del Centro America o dell'America Latina, l'età del consenso sessuale scende a tredici o addirittura a senza parlare della legge islamica, che autorizza rapporti sessuali anche con soggetti di età inferiore, pur nell'ambito del matrimonio. Appare quindi evidente, colleghi, che, qualora nel cellulare di un nostro concittadino fosse reperito un video di un rapporto sessuale avvenuto con un minorenne di anni quattordici in uno di quei Paesi dove comunque ciò è consentito, questo nostro concittadino, nonostante ciò, sarebbe perseguibile in Italia e non potrebbe invocare a sua difesa l'assenza di doppia incriminazione. Questo avviene perché la tutela dell'infanzia viene ritenuta un valore di altissimo rilievo, meritevole di tutela assoluta, a prescindere dalla latitudine del luogo ove il reato viene commesso. Altrettanto si deve riconoscere per la tutela della maternità e del diritto di un figlio ad avere e conoscere il padre e la madre biologici. Non si tratta però solo del reato di violenza sessuale; in sede di dichiarazione di voto vi suggerirò di riflettere su un altro reato. Per questo la gestazione per altri e il commercio dei neonati non possono essere tollerati, anche se avvengono in Paesi in cui ciò è lecito. Le pregiudiziali quindi vanno respinte, perché tutto del tutto infondate in fatto e in diritto.

tendiamo e vogliamo e speriamo e ci auguriamo che la maternità surrogata diventi un reato universale. Questa è la nostra posizione. *(Applausi)*. Qualsiasi norma che va in questa direzione per noi è giusta. E ciò anche perché con il disegno di legge in esame sostanzialmente evitiamo che alcuni cittadini riescano ad aggirare la legge italiana, andando all'estero dove la pratica della maternità surrogata legale, concependo quindi il bambino per cercare poi il riconoscimento giuridico nel nostro Paese. È tutto qui. Visto e considerato che questa è una nostra opinione e quindi potrebbe essere assolutamente oggetto di discussione e qualcuno potrebbe anche pensare diversamente, leggo - avendomi insegnato voi che l'Europa sta sempre sopra di tutto che sono molte le fonti giuridiche che, a causa dei gravi effetti della pratica sui più deboli, donne e neonati - abbiamo parlato dei bambini, ma ci siamo dimenticati di parlare delle donne, un piccolo particolare condannano la maternità surrogata. Il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni contro la maternità surrogata. Ricordo la risoluzione del 5 aprile del 2011

che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono utilizzati come una merce. E lo fa ritenendo che la pratica della gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani. la risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 che, al paragrafo 82, condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali. La risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, al paragrafo 48, chiede nuovamente di far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata.

tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani, prendendo di mira nel contempo soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili, evidenziandone il grave impatto sulle donne, sui loro diritti, sulla loro salute e uguaglianza di genere. E sottolinea le implicazioni transfrontaliere chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali. E poi ci sono anche delle sentenze della Corte costituzionale.

sfruttando il loro corpo per soddisfare un loro desiderio. *(Applausi. Commenti).* Questo sì che è il ritorno al Medioevo: ricchi committenti che pagano le donne povere, sfruttando il loro corpo, soprattutto donne immigrate

che mi fa venire i brividi solo al pensiero. Mi domando: ma la sinistra, che ha sempre difeso le donne e i deboli, dov'è su questo punto? Dove sono Dove sono le femministe? La cosa grave è che alcuni interventi di oggi li hanno svolti proprio delle senatrici. Ma come è possibile che il diritto della donna alla propria dignità

diversi tra loro, ma che appartengono alla sfera dei cosiddetti temi eticamente sensibili: penso a questo tema delicatissimo o, su un altro piano, al fine vita; penso al rispetto della volontà delle donne nell'applicazione della legge n. 194 del 1978. Cito questi tre temi che sono nel dibattito pubblico. Quando si parla di questi temi, si dovrebbero

estremismi e si dovrebbe cercare di fare dei ragionamenti che riguardano anche, se non soprattutto, la coscienza delle persone, anche dei singoli parlamentari. Penso quindi che trattare temi come questo debba innanzitutto significare capire. Io non ho difficoltà - il mio Gruppo lo sa, ne abbiamo parlato - a dire favorevole *tout-court* alla gestazione per altri. Io penso che invece questa possa e debba essere, per chi la vuole praticare - e a questo sono favorevole un dono, un altruismo. Questo io lo accetto, lo condivido. Penso che sia un giusto corrispondere a un bisogno, a un desiderio di maternità e paternità o comunque di possibilità di avere un figlio, anche attraverso la gestazione per altri, quando questa è un dono. Non condivido altre modalità, ma è un'opinione mia personale e io rispetto chi ha un'opinione diversa. Aggiungo anche un'altra considerazione, se mi riesce senza particolari polemiche. È noto che questa pratica, che - è vero - avveniva e avviene anche e soprattutto da parte del mondo occidentale più ricco nei confronti di Paesi e di situazioni

dietro a questo c'è anche qualche rigurgito di omofobia e ciò è assolutamente intollerabile. *(Applausi)*. Non sto insultando nessuno: sto dicendo che qui c'è anche una non detta discriminazione.

che prevedono al massimo - come fate voi - fino a tre anni. Questa è veramente una norma manifesto che voi volete sventolare, sapendo che è anche inapplicabile. Ci sono, infatti, tanti Paesi che regolano in maniera diversa la gestazione per altri. Alcuni lo ammettono come dono altruistico e basta, altri lo ammettono anche in termini commerciali, altri ancora lo vietano. Quindi, se non c'è reciprocità,

una sessione di libertà al Parlamento, senza vincoli di mandato, e senza che si sventolino bandiere partitiche. Ogni parlamentare dovrebbe esprimersi liberamente con la propria coscienza, senza essere ricattato da

Ci sono opinioni diverse su come tutelare l'interesse del bambino. La Corte costituzionale ce lo ha detto più volte. Fatelo. Fatelo. C'è chi pensa che sia giusto procedere alle iscrizioni automatiche nei registri anagrafici. Le borboniche circolari dei prefetti che il Ministero ha fatto inviare sono francamente ridicole e offendono anche la sentenza della Corte costituzionale, oltreché il buonsenso. C'è chi pensa, invece, che la via maestra possa essere quella delle adozioni velocizzate, quasi in tempo reale. Queste soluzioni (ognuno può scegliere quella che vuole, in quanto

Bisogna che tutti noi ci arrendiamo a un fatto: la società cambia, il mondo cambia. Io stesso, che sono un *boomer* del Novecento, non mi rendo conto di alcuni cambiamenti

Questo mondo è dentro di noi prima che ve ne rendiate conto, ma norme di questo tipo dicono che non ve ne rendete conto.

Signor Presidente, ringrazio la relatrice, senatrice Campione, per la sua esauriente introduzione a questo argomento i colleghi della maggioranza, senatori Zanettin e Romeo, che hanno portato forti argomenti sui fondamenti giuridici e su documenti europei che hanno condannato in modo molto chiaro e netto la surrogazione di maternità. Ringrazio soprattutto i colleghi dell'opposizione, che hanno presentato e sostenuto le questioni pregiudiziali, perché ci hanno rivelato qual è il pensiero dietro la difesa della pratica della cosiddetta surrogazione di maternità. Il pensiero è che va bene che ci sia il commercio di bambini, va bene ridurre le donne in schiavitù e lasciare che le famiglie ricche possano approfittare di donne che si trovano in situazioni di bisogno, molto spesso, anzi quasi sempre, in Paesi di quello che si chiamava il terzo mondo, certamente meno ricco del nostro. *(Applausi)*. Va bene per voi, per una serie di ragionamenti: perché poi ci sarà la Corte di giustizia europea; perché c'è il tale regolamento. C'è il regolamento della libera Il servizio di schiavitù e di acquisto dei bambini non è un servizio!

che può darsi siano veri. Non lo sappiamo perché, essendo una pratica illegale, non lo sappiamo. È scritto che l'80 per cento delle surrogazioni di maternità viene praticato da coppie eterosessuali. Può darsi. È una pratica vergognosa allo stesso modo! *(FdI)*. Proprio la senatrice Maiorino ha parlato di una nostra presunta intenzione di limitare il diritto all'aborto stabilito dalla legge n. 194. È falso, è completamente falso! Ricordo, invece, che nei contratti commerciali cui vengono sottoposte le madri surrogate, quelle che effettuano la surrogazione di maternità, ci sono degli impegni per cui, siccome il bambino che hanno in grembo è merce altrui, perché comprata dagli altri, queste donne, per contratto, possono abortire solo se lo decide la coppia, padroni. Questa è limitazione del diritto all'aborto, questo lo è! *(Applausi)*. Così come è una limitazione alle libertà personali l'impegno a non assumere una serie di farmaci, ad avere un certo stile di vita durante questa gravidanza per altri,

per cui i ricchi hanno comprato il bambino, la donna povera non si può curare e può abortire solo se lo decidono i padroni!

c'è gente che compra i bambini. Allora, dobbiamo dire che va bene e riconoscere il diritto ad essere immediatamente, senza ritardo, riconosciuti come genitori, pur essendoci una genitrice (e a volte anche un genitore) che chissà dov'è, che è stata tacitata con dei soldi. Sappiamo che ci sono state delle cause, in Paesi come gli Stati Uniti d'America, dove la donna che ha portato avanti la gravidanza ha cambiato idea e voleva tenere il bambino. C'è stato un caso, portato anche qui in Senato, di una donna che voleva tenere il bambino. Tra l'altro, caso anomalo, anche l'ovulo era suo,

madri, è chi vuole prevenire l'approvazione di questa norma.

perfetta, con tutti i valori a posto, riguardante i cani e i gatti. *(Applausi)*. Questo regolamento, all'articolo 8, dice che è vietato allontanare i cuccioli dei cani e dei gatti dalla madre prima dei sessanta giorni, se non per gravi motivi certificati dal veterinario. *(Applausi)*. Allora, la tutela delle madri dei cani e delle madri dei gatti deve essere almeno messa sullo stesso piano della tutela delle madri alle quali il bambino viene tolto subito per contratto. Ci avete accusato di ideologia. Siamo d'accordo, se per ideologia si intende difendere la dignità delle persone, delle madri, dei bambini, che hanno diritto a sapere chi è il loro padre, chi è la loro madre, hanno diritto a non essere merce.

non volevamo intervenire in dichiarazione di voto, ma mi sembra doveroso e imprescindibile, anche perché abbiamo appreso con favore dal senatore Zanettin che non stiamo per approvare un reato universale. Dovrebbe spiegarlo a Giorgia Meloni e a tutto il Gruppo Fratelli d'Italia che, con roboanti annunci sul loro sito ufficiale, il 3 luglio 2024, scrivono: «Con il via libera della Commissione giustizia del Senato al disegno di legge che introduce il reato universale di maternità surrogata, fortemente voluto da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni, diciamo basta…» e via discorrendo. *(Applausi)*. Quindi Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno mentito sulla pagina ufficiale del loro Gruppo

nessuno può sapere come sia nato quel bambino; il dubbio viene solo se la coppia dinanzi all'ufficiale giudiziario è omosessuale, oltretutto solo se è composta

passa sotto silenzio. Quindi ce l'avete solo con le coppie omosessuali maschili; ce l'avete coi papà. Vogliamo salvare le mamme, ma spariamo addosso ai papà. Il senatore Romeo ha fatto un ampio *excursus* sulle risoluzioni approvate dall'Unione europea, in cui specifica chiaramente donne vulnerabili, Paesi in via di sviluppo, sfruttamento commerciale, abuso nei confronti di donne che siano finanziariamente e socialmente vulnerabili, su cui nessuno di noi è in disaccordo. Siamo totalmente d'accordo su questo, ma esiste una norma che si chiama solidaristica, per la quale non c'è sfruttamento, non c'è passaggio di denaro, non c'è commercializzazione. Facciamo finta di negare questa evidente verità, che esiste per esempio in Canada, che non è un Paese sottosviluppato *(Applausi)*, o vogliamo dire che Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, Paesi dove questa norma è legale, siano Paesi poveri e senza diritti, come ha detto il senatore Romeo? Quindi, apprendiamo che tre grandi potenze mondiali sono Paesi sottosviluppati, dove non c'è democrazia. Dopodiché, si è parlato tantissimo della questione contratto e commercializzazione. misura solidaristica, com'è ben specificato, ad esempio, nel disegno di legge presentato dalla mia forza politica, con prima firma Castellone e che ho sottoscritto anch'io, perché in esso si parla di una forma solidaristica. Sapete che cos'è la solidarietà? Vi faccio un esempio: donazioni di organi e trapianti. È vietata anche la commercializzazione degli organi e nessuno si permette di dire che si possa vendere un rene o un polmone a fini commerciali Infatti, si parla di tratta d'organi e quello è un reato. Ebbene, vi informo che se io volessi donare un rene a un mio familiare, o a un mio amico che ne ha bisogno per un'insufficienza renale, Io mi posso privare per tutto il resto della mia vita di un mio organo, ma voi mi volete dire che se io voglio portare avanti una gravidanza per una mia amica, che magari ha la sindrome di Rokitansky, non lo posso fare. Eppure io l'utero non glielo regalo, me lo tengo. *(Applausi)*. Resta mio, non è una

abbiamo una lunga discussione generale in cui tutti potranno intervenire. Colleghi, non mi costringete ad interrompere la seduta, non mi costringete ad interrompere la seduta, c'è una lunga discussione generale in cui tutti potranno intervenire. Prego, senatrice Pirro. Quando i colleghi, arrivati dal Medioevo, mi lasceranno parlare... Quindi, i colleghi maschi della maggioranza stanno cercando di dirmi che l'utero non è mio? E di chi è, vostro? Dello Stato? Di chi è? Fino a prova contraria, i miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio

il mio utero? Abbiamo appreso che l'utero delle donne italiane non è di loro proprietà, ma è dello Stato: siamo al comunismo degli organi. Il comunismo vi piace solo quando pare a voi. Quindi, ripeto, posso donare un rene, ma non posso prestare il mio utero, se lo voglio fare. Io donna italiana, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, indipendente economicamente, non posso fare quello che mi pare del mio corpo: quindi siamo anche al divieto di aborto, perché è lì che vogliamo arrivare. Se dobbiamo preservare la natalità, io non sono libera di decidere cosa fare del mio corpo? mio corpo? Spiegatemelo, perché è questo quello che arriva dai banchi della maggioranza. *(Commenti)*. Io ritengo fondamentale che vengano votate queste pregiudiziali. Colleghi, se non si riduce il brusio dovrò sospendere la seduta. Vi prego, c'è una lunga discussione generale in cui si può intervenire. Un'altra delle cose sentite è che si è contrari a questa pratica perché se l'ovocita è della gestante poi ci sono poi ci sono dei vincoli e non può decidere di tenere il bambino. È per questo che le cose vanno regolamentate; è per questo che abbiamo presentato un disegno di legge. Le cose vanno non vietate, ma regolamentate. Noi chiediamo che ci sia la maternità surrogata solidaristica, e all'interno del nostro disegno disegno di legge si prevede che assolutamente il materiale genetico - gameti, ovociti e spermatozoi - non appartengano alla gestante o eventualmente al coniuge, e che arrivino da un'altra fonte, in modo da non instaurare nessun legame biologico che possa portare a contenziosi. Insomma, usciamo dal Medioevo e votiamo a favore di queste pregiudiziali.

Signora Presidente, ancora una volta abbiamo un Governo che si sta cimentando su temi di diritto con approssimazione dilettantistica, e lo fa perché evidentemente lo scopo principale di questa maggioranza e di questo Governo è quello di utilizzare quest'Aula per finalità propagandistiche. Quindi non si fanno scrupolo nel fare delle evidenti forzature su temi e principi di diritto che sono incontestabili. Il Governo vuole dire la sua sulla maternità surrogata ed ha diritto a farlo; però, dato che in Italia una legge che vieta la maternità surrogata esiste già e dato che non vogliono neppure metterla in discussione, si sono inventati questo fatto del reato universale.

Volete fare la voce grossa e in sostanza che cosa fate? Volete estendere il divieto che esiste in Italia anche al di fuori dei confini nazionali, ma non seguendo le norme del codice penale. Prima la collega Maiorino vi ha fatto un'elencazione dettagliata parlando di come funziona il sistema penale italiano e quando un reato commesso all'estero può essere punito nel territorio italiano. Non voglio riaprire questo capitolo, però quello che voglio dire è che voi in questo caso state dicendo che la legge italiana insegue gli italiani in ogni angolo della Terra. Quindi, se un italiano va negli Stati Uniti o in Canada, dove questa condotta non costituisce reato, sarà punito al suo rientro in Italia. Quindi la legge italiana si applica in ogni angolo della terra. Scusate, colleghi, ma non vi suona un po' come un delirio di onnipotenza? Colleghi, un conto è dire che esistono reati universali: questi reati sono universali perché sono riconosciuti tali dalla comunità internazionale, non perché lo dice l'Italia o perché lo dice la Meloni. Sono reati che sono universalmente riconosciuti come reati universali. La maternità surrogata non è e non potrà essere reato universale, per il semplice fatto che in molti Paesi, come gli Stati Uniti o il Canada, è riconosciuta come una pratica legale. State cercando di confondere la regolamentazione con una casistica di cui nessuno sta parlando. Voi parlate della commercializzazione, che è cosa diversa rispetto al tema che dovremmo oggi affrontare in Aula.

valida in ogni angolo della terra. Forse, però, ci sarebbe bisogno di una buona dose di umiltà, per capire che non siamo gli imperatori del mondo. Voi state cedendo al fascino dell'impero, l'impero del diritto italiano, che deve essere valido e imporre una verità morale a tutti i Paesi del mondo e deve interferire anche all'interno di territori dove ci sono altri Stati sovrani.

Volete affrontare i problemi sociali non per risolverli. Fate dei provvedimenti, come il decreto sicurezza, che mirano non a risolvere i problemi, ma ad usare la politica del manganello. Adesso c'è un'altra novità: non vi basta più lo Stato autoritario, ma volete anche uno Stato confessionale, volete interferire sulle libertà morali dei cittadini, nelle scelte più intime delle persone. Volete fare i moralizzatori del diritto, con una moralizzazione sistematica che ignora i problemi psicologici che si andranno a creare in quei bambini che si troveranno ad avere dei genitori incriminati per il semplice fatto di averli voluti mettere al mondo. Colleghi, ma io dico, perché questo desiderio di controllare tutto? Perché questa paura del pluralismo? Non sarà che avete paura che il pluralismo possa mettere in discussione le vostre convinzioni, questa idea di essere depositari di una verità assoluta? Guardate che in democrazia non esiste una verità assoluta, esiste una verità che si mette in discussione La moralizzazione estrema, questa moralizzazione del diritto, è estremamente pericolosa, perché ricordatevi che la moralizzazione del diritto genera anche dei nemici immaginari. Ricordatevi la caccia alle streghe: è solo la forza della ragione che può arginare questo delirio collettivo. suggeriva l'Illuminismo, appunto. L'Italia è un grande Paese, però voi state gettando un'ombra su questa grandezza; state mettendo in ridicolo l'Italia sul palcoscenico internazionale e dinanzi al mondo intero dei giuristi. *(Applausi)*. L'Italia può essere un Paese grande, ma deve porsi come esempio di una democrazia pluralista che rispetta le differenze e rispetta anche il diritto sancito in altri Stati sovrani.

potessero essere invincibili. Però vedete, colleghi, alla fine sono stati proprio i dinosauri che si sono estinti.

di cambiare la normativa che riguarda un reato che tale rimane. Dai toni che ho sentito nella discussione finora, mi pare invece che si cerchi di discutere una cosa diversa, attribuendo colpe a prescindere, come si suol dire. Vedo però che poi la discussione non interessa molto, visto che i banchi di fronte a me sono in gran parte vuoti. Vorrei partire da una parola che considero fondamentale in questa discussione.

tutto tondo. Mi domando perché non ho sentito la parola sfruttamento in quest'Aula quando abbiamo discusso delle donne indiane delle terre di Latina e della loro impossibilità di chiedere soccorso per un lavoratore che era stato

del lavoro che si svolge anche nel nostro Paese prevede lo sfruttamento. Mi viene in mente in realtà che noi usiamo questa parola solo quando riguarda la sfera riproduttiva. Se riguarda la vita quotidiana delle persone, la loro condizione di indigenza, di sfruttamento e di impossibilità di determinare alla loro vita, allora la parola sfruttamento scompare. Non appena si parla della sfera riproduttiva, improvvisamente questo tema

il tema. È possibile che le donne siano comunque ritenute soggetti vulnerabili non in grado di prendere decisioni autonome su se stesse? Dobbiamo ogni volta ricominciare da lì, cioè dal fatto che noi siamo esseri senzienti, non siamo soltanto fattori riproduttivi. Forse allora avremmo diritto di parola dentro tutto questo,

siamo anche in grado di giudicare ciò che è sfruttamento e ciò che invece è volontà propria. Poi ognuno può decidere e ognuna soprattutto può decidere se vuole o meno affrontare questa discussione, il tormento che essa provoca e la necessità di decidere se farlo o non farlo. Ha diritto però di farlo lei. farlo lei. Io non ho mai pensato che si possano comprare i bambini e quindi non penso che possano essere delle partite commerciali di compravendita, ma rivendico il diritto che le donne possano decidere del loro corpo fino in fondo perché quello che c'è dietro una parte della discussione che ho sentito stamattina non è se la gestazione per altri è commerciale o meno, ma se le donne possono decidere di loro stesse o se sono piccole, vulnerabili e incapaci e quindi qualcun altro deve decidere per loro.

corso di una campagna elettorale in una Regione ho sentito dire che le donne devono fare i figli. No, le donne decidono se fare i figli o non farli, hanno diritto di determinare loro stesse. E allora credo che quando un Paese torna ad avere il problema di discutere della libertà delle persone su loro stesse siamo troppo vicini a ciò che si chiama Stato etico, lo stesso che condanniamo quando invece parliamo di questioni di politica internazionale.

per riproporre un reato che peggiora una condizione precedente, perché le norme non sono neutre e possono decidere poi forme di discriminazione che nella normativa precedente non c'erano. Ebbene, invece di dedicare tanta energia a inventarsi nuovi reati e distrazioni di massa rispetto ai problemi del Paese, perché non discutiamo seriamente di cosa potremmo fare dal punto di vista del contrasto effettivo allo sfruttamento? Perché non discutiamo del fatto che dobbiamo smetterla di considerare le donne soggetti deboli da tutelare e cominciamo invece a porci il problema di perché sul mercato del lavoro non godono di Perché non diciamo insieme in quest'Aula che in Sicilia si sta facendo una discussione insopportabile che vuole ridurre la rappresentanza delle donne? Perché poi, quando parliamo delle cose che riguardano i nostri poteri, improvvisamente quello maschile deve comunque emergere e sovrastare.

anche chi è nato. La cosa vera che c'è, alla fine, dentro questa modalità, ma anche dentro altre leggi che abbiamo dovuto discutere in quest'Aula in questi tempi, in questi tempi, è che alla fine noi stiamo negando ai bambini e alle bambine di essere uguali agli altri bambini e bambine. Stiamo decidendo che ci sono dei bambini che hanno diritto di essere cittadini italiani e di avere tutte le opportunità e altri bambini e bambine che invece queste opportunità non le hanno. Lo abbiamo recentemente deciso anche in un'altra situazione, perché abbiamo deciso in quest'Aula che i bambini possono andare in carcere e la mia paura - lo dico esplicitamente è che se poi si vuole fare una bandiera della norma di cui stiamo discutendo, potremmo scoprire che questi bambini, quando tornano nel nostro Paese, devono denunciare il fatto che sono figli di un reato e possono anche direttamente essere accompagnati alle patrie galere, a proposito di uguaglianza dei diritti E allora, da questo punto di vista, siccome diciamo sempre che invece apprezziamo le convenzioni internazionali e ne vogliamo essere attori - non lo siamo, per esempio, sulla tratta e lo sfruttamento, ma potremmo invece esserlo su altre

a quei bambini e a quelle bambine di non subire nessuna discriminazione, ma direi di più: dovremmo garantire a quei bambini e a quelle bambine di non avere addosso uno stigma,

cui la nascita di quel bambino o di quella bambina è segnata già da uno stigma è un modo per rendere quel bambino colpevole di cose per cui colpa non ha, salvo che non vogliamo, in una versione sempre più medievale del nostro Paese, tornare al fatto che le colpe dei padri ricadono sui figli,

ma possono determinare nella loro finta neutralità delle grandissime discriminazioni. Questa norma ne introduce varie; la prima che introduce è quella per cui l'autodeterminazione delle donne è *sub iudice* del valore e dei giudizi che dà lo Stato o che dà la parte maschile dello Stato. La seconda che introduce è quella che i bambini e le bambine non sono tutti uguali e non hanno gli stessi diritti. La terza, anche se il presidente Romeo non è riuscito a esprimere fino in fondo questo concetto, è che noi pensiamo di introdurre norme vendicative nei confronti delle coppie omogenitoriali e in particolare delle coppie omogenitoriali omogenitoriali maschili. La domanda è: perché? Non è vero che quella fattispecie non fosse già vietata, quindi non ce n'era alcun bisogno e il fatto che si introduca questa legge in realtà segna una cosa che a me onestamente fa paura: devo ricominciare ad affermare che io sono libera e che nessuno può decidere di me e della mia vita. Signor Presidente, parlo per primo da questa parte del "gregge", come qualcuno ci ha definito; un gregge che, però, è composto da persone che ragionano col proprio cervello, che pensano e non rispettano *Diktat,*

Inizio questo mio intervento con una frase di una grande donna femminista, che ha scritto: la verità è che le leggi dello Stato non possono ignorare le leggi della natura. È una frase di Oriana Fallaci, sicuramente non scritta e non pensata in riferimento all'utero in affitto, alla maternità surrogata o alla gestazione per altri (GPA), che dir si voglia, ma che racchiude in sé lo stesso senso della nostra legislazione e della nostra vita. Nel caso della procreazione, la legge della natura recita che ogni nato è figlio di una donna e di un uomo. È una notizia clamorosa, ma oggi, 16 ottobre 2024, cento delle bambine e dei bambini è nato dall'incontro dell'ovocita di una donna con il seme di un uomo. Ciò però non significa che la nostra contrarietà a questa pratica dell'utero in affitto, a differenza di quanto abbiamo sentito da quasi tutta l'opposizione, supportata da molte associazioni LGBTQ+, sia una battaglia contro la famiglia omogenitoriale, perché, com'è stato ribadito, quasi il 90 per cento delle famiglie

pratica aberrante, che trasforma il concepimento e la nascita in merce e umilia la dignità della donna, donna, che non presta un organo, ma partorisce un figlio che non può essere merce. *(Applausi)*. Non si tratta di donare o vendere un rene: si tratta di donare o vendere un figlio. È una contrarietà, la nostra, che inizia con il quesito di chi sia effettivamente il genitore del nascituro. Sarà quello individuato seguendo il criterio del *favor legis,* quindi quello per cui saranno la legge e il contratto conseguente, sottoscritto dalle parti, a stabilire i ruoli genitoriali, indipendentemente da ogni legame biologico affettivo o esistenziale, o si dovrà seguire il cosiddetto *favor veritatis*, per cui si dovrà tener conto dei legami biologici esistenziali? Nel caso in cui la legge decidesse di stabilire quali sono considerati i genitori, al di fuori, naturalmente, dell'istituto dell'adozione, quale diritto vorrebbe tutelare questa legge? È giuridicamente concepibile un diritto al figlio? Contro chi potrebbe esser fatto valere: nei confronti del *partner*, anche non in grado di figliare, nei confronti della società o nei confronti dello Stato? No, le persone sono da considerarsi soggetto e non oggetto di diritto. Il diritto al figlio non può essere né configurato, né rivendicato dalle coppie che siano omosessuali o meno, perché contrasta con la natura e la dignità del figlio. La dignità viene violata ogni volta che si attribuisce un prezzo a qualcosa.

può avere dignità. La donna che presta gratuitamente, in pochissimi casi, o vende o affitta, nella maggior parte dei casi, il proprio grembo per la gestazione è ridotta a un'incubatrice, interrompendo il legame biologico tra se stessa e la creatura dentro di lei. I bambini diventano progettabili e acquistabili da genitori individuati per legge o per contratto.

di cui si possono scegliere altezza, peso, colore dei capelli, degli occhi e anche della pelle e gruppo sanguigno. Le stesse agenzie forniscono, sempre a pagamento, gestanti di cui si può scegliere stato civile (*single*, sposate, divorziate) e fascia d'età (dai diciotto ai situazione è completamente contrastante con il desiderio naturale di genitorialità. Il figlio arriva non progettato; magari si sogna come lo si vorrebbe, ma non si progetta. Comunque esso nasca (con capelli biondi, senza capelli, con occhi verdi, blu o neri, con la pelle più o meno chiara o scura, alto o basso, grasso o magro), è sempre il più bello per i propri genitori. Coloro che non possono avere figli, oppure, potendoli avere, ricorrono comunque all'istituto dell'adozione (dopo un'accurata scelta e dopo aver dimostrato la loro stabilità morale e materiale), non possono scegliere il figlio che potranno adottare e che diventerà loro. Gli arriva così come stabilisce la legge. la legge. Non scelgono prima che tipo di bambino o bambina e di che età potranno avere nella loro famiglia. Lo accolgono per amore verso i figli e non per avere un figlio più o meno bello, più o meno alto, più o meno biondo. Questa possibilità di scelta trasforma un pur comprensibile desiderio in un diritto per pochi. È noto, infatti, quanto costi l'utero in affitto negli Stati dove tale

Questo trasforma il desiderio in un sogno per pochi ricchi. Ma chi paga il prezzo vero? Sono sempre le gestanti, solitamente la parte debole: le donne povere, che prestano il loro corpo e il loro grembo per figli di altri, non sapendo però che devono anche rinunciare alla volontà di tenerselo. Non si può dimenticare

il feto che porta in grembo. Quel feto non potrà mai tenerselo per lei, anche se cambia idea. A questo noi vogliamo far scadere la la cosa più alta che la natura ci ha dato: la possibilità per le donne di avere figli, figli che dovranno dimenticare e che non conosceranno mai la propria madre naturale, pur sapendo - e e questo lo prova la scienza - che il legame tra chi è partorito e chi partorisce è indissolubile. Gli studi di psicologia dello sviluppo hanno reso palese tutto ciò. Legittimare, con la pratica dell'utero in affitto, l'interruzione di questo percorso che si crea tra la madre, il feto e poi il figlio che esce dal suo utero, non da quello di un altro, non da quello di chi l'ha comprato, ci

Ci espone a rendere la nascita un mercimonio. Questo non lo diciamo noi. Non lo dice questo gregge retrogrado di centrodestra, di destra o di Fratelli d'Italia. Questo lo dicono le cento femministe che hanno firmato una lettera, nell'aprile del 2023, contro questa pratica. Lo dicono stilisti di grido, dichiaratamente omosessuali, per i quali il bambino deve avere una madre e un padre, che se due omosessuali decidono per amore di stare assieme qualche rinuncia la devono fare, perché il bambino deve avere una madre e un padre. Insomma, tutto quello che viene raccontato, *fake* e più neanche tanto *news*, su bambini di serie A e serie B, non è vero. Basta che un genitore riconosca il figlio all'anagrafe italiana, infatti, ed il bambino avrà diritto a tutto ciò cui hanno diritto i bambini che hanno due genitori anziché uno; e l'altro genitore lo può sempre adottare. Noi non vogliamo bambini di serie A e serie B, assolutamente, ma respingiamo con forza le accuse di chi invece dice che noi questo facciamo non tutelando i diritti dei bambini. Noi lo facciamo per tutelare i diritti dei bambini. È una battaglia, la nostra, per non adagiarsi sul fatto che la riflessione pubblica accolga passivamente i traguardi della scienza e della tecnica, dimenticandosi la legge della natura, e per chi, come me crede, anche i precetti della religione.

utilizzerò questo tempo in discussione per sottoporre a questa platea delle domande che ho rivolto per prima a me stessa, non sempre trovando risposta. Chissà che oggi qualche mente saggia non possa illuminarmi.

che mi hanno fatto già sorgere il primo dubbio. È o non è questo il luogo, il Parlamento, dove da rappresentanti del popolo si lavora per qualcuno e non contro qualcuno? Sono io che mi sono persa qualcosa, in una legislatura da deputata e in una quasi a metà da senatrice?

contro chi o contro cosa dovrebbero andare questi ed altri provvedimenti. Non chiedo per un amico, chiedo proprio per me stessa, perché quelle che vedo io sono persone. In In questo caso specifico sono bambini e qui mettete pure il punto esclamativo, se vi aggrada. È di questo che stiamo parlando ed è questo che rende ancor più deplorevole l'azione che state portando avanti. In Italia, com'è stato ricordato e come sicuramente vi sarà noto, la maternità surrogata è già vietata e penalmente sanzionata dalla legge n. 40 del 2004, che norma la procreazione medicalmente assistita. Ribadiamo, per coloro che ci ascoltano fuori da qui, ma anche perché non si sa mai avessi capito male io, cosa vuole fare la maggioranza. La maggioranza vuole criminalizzare questa pratica, anche quando viene effettuata dai cittadini italiani all'estero, in Paesi in cui è legale e regolamentata. Qui delle due l'una: o io devo tornare all'università o questo è un obbrobrio giuridico. *Spoiler*, notizia: mi dispiace per quelli che vogliono essere difesi dall'ideologia LGBT e da cui può sembrare, leggendo le parole della relatrice cui facevo riferimento prima, abbiate avuto una sorta di mandato, di mandato, ma non si può fare, quindi dovete trovare armatura ed elmetto in qualche altro strumento. Non per infierire, ma c'è un'altra notizia che, per onestà intellettuale, mi tocca darvi. Ad avvalersi dello strumento della maternità surrogata all'estero, dov'è legale e dove noi non possiamo andare a dire cosa sia legale e cosa no, sono per il 90 per cento coppie eterosessuali. Volete sapere contro chi veramente va un provvedimento del genere, chi danneggia e chi non tutela? I bambini. Pur di alzare le barriere ideologiche siete pronti - è questo torna sempre - a rischiare di creare nuove discriminazioni. Quale diritto superiore stiamo tutelando, se condanniamo un bambino alla privazione di una relazione giuridica con chi lo ama e chi lo accudisce? Siamo soltanto violando i principi di convenzioni internazionali e le indicazioni della stessa Corte costituzionale, che si è pronunciata sull'argomento con la sentenza n. 33 del 2021. La Corte, ponendo al centro la dignità della donna, da una parte, e i diritti del bambino nato attraverso queste pratiche, dall'altra, è costretta a ricordarci che, quando una nuova vita viene al mondo, lo Stato non può ignorarne l'esistenza. Questo bambino, questo individuo, ha diritti, incluso quello di essere riconosciuto come figlio e di avere genitori che lo accolgano, lo proteggano e lo crescano, siano essi biologici o di intenzione, ovvero genitori che non hanno contribuito col proprio patrimonio genetico a concepire il minore, ma che con lui hanno intenzione di instaurare un rapporto familiare. Ma voi immaginate cosa potrebbe succedere se il genitore intenzionale, cittadino italiano, che ha fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero in un Paese in cui è legale, per timore di sanzioni, rinunciasse a trascrivere l'atto di nascita del figlio, lasciando quel bambino senza un legame giuridico con uno dei due genitori? Vi chiedo quale sia il vero obiettivo di questa proposta: vogliamo davvero tutelare donne e bambini o stiamo solo cercando di imporre un modello di famiglia? Ma davvero il vostro odio e la vostra paura per le famiglie omogenitoriali arrivano al punto di voler discriminare i bambini, i loro bambini, per le scelte di vita dei loro genitori? La famiglia è dove ci sono amore e cura, non dove ci si adatta a uno schema prestabilito; che poi - permettetemelo - Avete davvero riflettuto su tutte le conseguenze delle vostre azioni, innanzitutto - lo ripeto ancora una volta - su bambini che non hanno alcuna colpa, ma che invece hanno soltanto diritti, come tutti gli altri? I bambini e le famiglie non devono pagare il prezzo di una vostra cieca battaglia, guidata da un'ideologia reazionaria e oscurantista. Abbiamo il dovere di normare, sì, ma con giustizia e umanità, senza perdere di vista il bene supremo, il rispetto della dignità e dei diritti di ogni individuo, a prescindere dal modo in cui sia venuto al mondo, in questo mondo, che noi abbiamo il dovere di fargli trovare giusto e civile. *(Applausi)*.

dire. Credo personalmente che i temi oggetto della discussione odierna richiederebbero non dico pacatezza, ma sicuramente, sicuramente, com'è stato detto, meno furore ideologico, toni più rigorosi, un po' più seri, un atteggiamento anche meno propagandistico, oserei dire - proverò ad argomentare perché - e anche forse un po' più di coerenza e di onestà intellettuale. Vengo al tema e lo farò a partire da me stessa, non nascondendo che intanto, su questo terreno, mi sembra difficile che qualcuno abbia delle verità assolute che possa affermare con assoluta certezza cosa è giusto e cosa è sbagliato. Affrontiamo temi stamattina che dovrebbero un po' attraversarci tutti, in termini almeno di dubbi. Poi i dubbi sono, come spesso si dice, sinonimo di intelligenza, ma soprattutto - io dico in questo caso - di onestà.

i diritti dei bambini, quelli che non hanno fatto nessuna scelta e che sicuramente, in questo contesto, sono i soggetti più vulnerabili, ai quali abbiamo il dovere, tutti insieme, come Stato e come comunità, di garantire una crescita all'interno di un una condizione di affetti e di certezze, anche di diritti e di *status*. è poi il desiderio di diventare genitori, che dev'essere rispettato per tutti e credo che anche su questo terreno dovremmo interrogarci un po' di più e meglio. È un desiderio che non può certo diventare mai senza limiti, ma che è assolutamente legittimo, da guardare con attenzione e del quale mi sento di farmi carico. Poi, anche per ragioni di passioni politiche che ho maturato in questi anni, tema sicuramente per me principale è il rispetto della dignità della donna, del suo corpo e della sua inviolabilità; anche, come diceva la senatrice Camusso, delle sue libertà di scelta. Insomma, sono temi - mi sembra - abbastanza complicati per essere derubricati in qualche applauso

grande strumento di governo, anche perché in tempi forse di vacche magre e di conti che non tornano, una norma in più o in meno nel codice penale costa zero, crea un po' di consenso, parla un po' alla pancia ed è molto facile.

lo è, secondo me, sia sul carico di disvalore sociale che voi volete attribuire e sul quale potrei dirvi che in alcune circostanze mi troverei d'accordo con voi; lo è sul piano giuridico, ma lo è anche sul tema dell'opportunità politica e di una drammatica occasione che avete sprecato

Io verrò dopo con tante perplessità, ma questo per dirvi come può essere assurdo il vostro provvedimento: lui l'ha fatto in buonafede, ritorna in Italia e noi che facciamo con quel ragazzo? che facciamo con quel ragazzo? Non gli riconosciamo il figlio? Non lo riconosciamo e smantelliamo quella famiglia? Non lo so, questo per dirvi l'abominio giuridico che avete prodotto.

confermato. Vi devo dire che l'ho registrato innanzitutto con molto dolore, perché speculare su queste cose mi sembra veramente oltre il limite del possibile

e non vi abbiamo sentito. Analogamente, dovrei ricordare al senatore Romeo che in quest'Aula il senatore Pillon addirittura diceva, nel caso del doppio cognome - e lei era sempre su quei banchi affianco a lui, ad applaudire

apprezzato molto il tono dell'intervento della senatrice Camusso, quando ha parlato di libertà di scelta. Penso che su quei temi ci dovremmo interrogare, perché io, per esempio, non ritengo che la prostituzione possa essere una libertà di scelta, ma credo che la legge Merlin abbia rappresentato un grande baluardo e un traguardo nel confronto, quando si è prefissa di punire. Si è affrontato Si è affrontato il tema con serietà e con rigore, con un confronto nelle Aule parlamentari, fuori dal furore ideologico, che è quello che invece voi mettete questa mattina nella discussione e dentro il provvedimento. Vi dico che personalmente non ho problemi a riconoscere che, secondo me, la GPA rischia di minare l'inviolabilità del corpo di una donna. Penso che sarebbe sbagliato girarsi dall'altra parte rispetto al fatto che è sicuramente uno strumento più disponibile nelle mani di chi può, a dispetto di chi è in una condizione di povertà - semmai sotto di scelta o meno - e non so quanto effettivamente sia libera quella scelta (non perché la persona sia fragile, ma perché è messa in una condizione di fragilità e di vulnerabilità). Credo che questi temi li dovremmo semplicemente affrontare con serietà e personalmente mi pongo così.

che potevamo arrivare a riconoscere i diritti delle donne, anche perché in questo Paese tale fattispecie è già reato e non c'è niente da aggiungere, perché non ci avete sfidato dicendo di provare a costruire una legge che limiti e vincoli il rispetto della tutela dei minori con una scelta chiara, quella indicata dalla nostra giurisprudenza e dalla nostra dottrina, dal 2017 al 2022 e ad oggi, con pronunce chiare, che penso possano definire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato? La Corte costituzionale ci ha indicato la strada e ci ha detto di cambiare e modificare, intervenendo sulle adozioni in casi particolari. Perché non ci avete sfidato su quel terreno? Perché non abbiamo costruito insieme un percorso di questo tipo? Perché? Perché vi interessava ancora una volta solo una norma manifesto propagandistica, che in questo caso però specula sui diritti delle donne, ma soprattutto dei minori. Quella era una risposta seria e rigorosa, che richiedeva però a voi forse un approccio diverso, più puntuale, meno propagandistico, meno da applausi, forse anche più difficilmente spiegabile; era necessario sicuramente costruire un percorso di maggiore condivisione. Eppure, la nostra elaborazione giurisprudenziale ce la indicava in maniera chiara. Per questo vi dico dispiace davvero molto per i toni, ma soprattutto per il modo in cui siamo arrivati a proporre il testo che oggi licenzierete. Poteva essere un'occasione per fare tutti insieme un passo in avanti; invece abbiamo tolto diritti ai bambini, non abbiamo tutelato di più e meglio quelli delle donne e sicuramente non abbiamo fatto un servizio all'interesse generale del Paese, ma probabilmente soltanto al vostro consenso e al vostro elettorato.

le rivolgiamo un saluto speciale, perché ricordiamo l'81° anniversario del disumano rastrellamento del Ghetto di Roma. Lo sdegno, che il presidente La Russa ha già manifestato, per la deportazione ci impone di riconoscere oggi il dovere della memoria come fondamento irrinunciabile di umanità, della nostra umanità.

Ci inchiniamo di fronte ai deportati, agli sterminati e ai sopravvissuti, che sono i testimoni di una verità storica assoluta. In loro ricordo invito l'Assemblea ad osservare un momento di silenzio e di raccoglimento.

il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare». Ebbene, Presidente, io e il mio Gruppo oggi ci sentiamo e vogliamo essere un po' partigiani, perché non possiamo e non vogliamo assolutamente rimanere indifferenti davanti a questo provvedimento sulla gestazione per altri, che ci ci è stato proposto con parole che a nostro avviso configurano un'aberrazione liberticida e un *nonsense* legislativo. Vogliamo usare la nostra volontà politica e umana per condannare questo provvedimento e lo facciamo nei termini del buonsenso, della denuncia politica e di un accorato appello, che rivolgiamo a tutti e a tutte. La ministra Roccella ha definito l'Italia un Paese all'avanguardia su questo tema. Ma all'avanguardia, scusate, rispetto a chi e rispetto a cosa? Quello che leggiamo è quanto di più lontano dalla consapevolezza dei nuovi indirizzi dell'evoluzione culturale e politica non dico dell'Italia e dell'Europa, ma dell'intera umanità; e non sto esagerando. esagerando. Pensiamo a tutti i tetti di cristallo - per dirla con le parole della presidente Meloni - che l'umanità infrange ogni giorno, come la progressiva, dolorosa e inesorabile conquista della parità femminile o il diritto di vivere una vita piena e felice, a prescindere dalla propria identità sessuale. Sono percorsi da cui non si può tornare indietro, a meno che non si perda il contatto con la realtà del mondo nel quale viviamo. L'evoluzione ci porta verso nuovi lidi e nuove frontiere, così come la scienza che oggi ci consente di fare e pensare cose inimmaginabili fino a poco tempo fa. Allo stesso modo, stiamo sviluppando nuove forme di cultura e non possiamo definirci all'avanguardia, se invece non ne prendiamo atto e non legiferiamo di conseguenza, in modo consapevole e rispettoso del diritto di tutte le persone. La gestazione per altri è tra queste nuove frontiere. Noi invece cosa facciamo? Cosa fa il Governo? Cosa fa questa maggioranza? Si è espressa ad esempio contro la proposta del certificato europeo di filiazione con cui l'Unione europea vuole garantire a tutti i bambini a tutte le bambine il riconoscimento di essere figli dei propri genitori, a prescindere dalle modalità riproduttive e dall'orientamento sessuale dei genitori stessi. Questo è possibile perché abbiamo infranto quei tetti di cui si parlava.

Devono quindi esistere una legislazione consapevole e responsabile e soprattutto un sistema giuridico e politico, come dice la nostra Costituzione con chiarezza, in cui lo Stato è in funzione della persona, non viceversa: la persona non è in funzione di questo Stato e di questo Governo. Cosa dice ancora questa maggioranza? Cosa dice oggi? Vuole trasformare la gestazione per altri in un reato universale, perseguibile ovunque in questo globo terracqueo, seguendo gli aspiranti genitori, anzi, diciamo perseguitandoli anche nei Paesi in cui è legale. I reati universali - semmai

Questa maggioranza vuole legiferare per punire la costituzione di una famiglia, pagare l'amore e la voglia di essere genitori con il carcere, ovunque essa venga ricercata, a prezzo spesso di sofferenze e sacrifici. Non esistono solo sfruttamento e mercificazione, ma anche altro. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, recita che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

Non c'è verità, c'è solo un comodo espediente populistico per avere il consenso parlando alla pancia del Paese. La Lega addirittura in questo suo dialogo con la pancia ha proposto un emendamento che prevede la reclusione fino a dieci anni e una multa di 2 milioni di euro. Quanta ossessione! Come definire tutto questo? Sicuramente degno solo di una politica feroce e violenta rispetto all'esercizio del diritto dell'individuo totalmente - ribadiamo - lontano dalla realtà.

concreta di perseguibilità all'estero, dove la GPA è legale; l'irragionevolezza del provvedimento, che colpevolizza chi desidera essere genitore, dopo aver provato ogni possibilità; irragionevolezza, perché punisce i bambini e le bambine, che con questa legge diventeranno invisibili e privi di tutele. Presidente, qui non si tratta di un mero capriccio, ma di un desiderio frustrato, che si è scontrato spesso con la natura, con la burocrazia e con leggi obsolete. Ci sono poi le modalità di lavoro che ci hanno portato a oggi.

È così che dovrebbe essere qui, con grande attenzione da parte soprattutto di questo Governo, che dice di aver superato la sua matrice ideologica, evolvendosi in ideologia completamente diversa da quella fascista, di cui Matteotti è stato vittima. Ci dovrebbe essere, quindi, più attenzione, attenzione, ci dovrebbe essere rispetto per le prerogative del Parlamento. Certo, ci possiamo scontrare, perché siamo diversi, ma poi da questo scontro deve nascere qualcosa qualcosa per il bene comune dello Stato rispetto al quale ci siamo impegnati di servire con fedeltà, lealtà e onestà. Quel che succede, invece, è che voi avete fretta, avete sempre fretta, come se si rincorressero delle emergenze, quindi questa è un'emergenza? Noi pensavamo che le emergenze fossero altre, il lavoro, le retribuzioni da fame, le persone che non riescono ad arrivare a fine mese, le donne che non riescono a riempire il carrello della spesa e stanno lì a vedere se i soldi che hanno in tasca bastano per comprare quello che hanno nel carrello della spesa, con molta vergogna e umiltà comunque devono lasciarlo là, perché non se lo possono permettere. *(Applausi)*. Oppure un'emergenza potrebbero essere le aziende che chiudono, che ci ricattano per non chiudere, per mantenere in attività le lavoratrici e i lavoratori o che ci propongono soluzioni alternative prive di alcun valore sociale, commerciale e industriale. Pensavamo fossero queste le emergenze. Avete sempre fretta, non ci permettete dubbi, osservazioni, contraddittorio; è scavalcata totalmente la prerogativa del Parlamento, dove appunto si dovrebbe parlare delle nuove frontiere dell'evoluzione culturale, dell'esistenza di posizioni diverse, di ideologie differenti, di sensibilità diverse e quindi fare sintesi, magari, con leggi laiche rispettose del diritto dell'individuo e di quelle Carte internazionali di cui spesso siamo stati tra i primi firmatari: la Carta dei diritti dell'Unione europea e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Proprio il nostro Parlamento dovrebbe ancora parlare dell'autodeterminazione delle donne, anche alla luce dell'emergenza culturale dell'educazione di genere: i dati dei femminicidi in Italia sono un bollettino di guerra. Invece no, no, entriamo a gamba tesa nella sfera dei diritti individuali che, come dice la parola, sono diritti che attengono solo alla persona. richiesta che rivolgo a tutti e a tutte: la famiglia non deve essere assolutamente un'arma politica, ma soprattutto non perpetuiamo quel brutto vizio di far decidere ai Governi sul corpo delle donne. Questa è una cosa gravissima, è una deriva pericolosissima. Parliamo di erosione dei diritti civili, ma noi non siamo questo, l'Italia non può essere questo. Se continuate così, se questa è la strada che volete percorrere, si rischia veramente di trasformare l'Italia in uno dei satelliti degli Stati più oscurantisti che stanno emergendo in Europa e questa cosa è gravissima. Ma poi, per cosa? La maternità non è solo gravidanza, è un sistema complesso di presa in carico, di cura, che esiste anche laddove non c'è parto, anche laddove non si può partorire. Concludo con un pensiero rivolto ai bambini, anche questa volta con una citazione. Ho iniziato con un mio conterraneo e finisco con una mia conterranea, Michela Murgia,

«Il bambino, la bambina, abbraccia quel che trova e ama quel che offri da abbracciare. Si spera che si cerchi di dargli il meglio, certo. Ma chi decide cosa è questo meglio?». Signor Presidente, colleghe e colleghi, in altre circostanze sarei stata ben felice di intervenire su un disegno di legge volto alla modifica della legge n. 40 del 2004; sarei stata ben felice di votare un disegno di legge volto ad abrogare la parte dell'articolo 13 che dispone il carcere per quei ricercatori italiani che volessero derivare cellule staminali embrionali dalle blastocisti umane sovrannumerarie destinate al congelamento distruttivo. Da decenni - lo ricordo a tutti - quelle cellule embrionali staminali umane, che a noi viene vietato di derivare dalle blastocisti, vengono importate dall'estero (non comperate, importate nell'ambito di progetti di ricerca) e poi si continuano a studiare, anche nel mio laboratorio. cellule staminali embrionali umane interessantissime, perché da queste vogliamo ottenere le cellule specializzate che poi si vorrebbero sostituire nelle varie malattie degenerative. Le importiamo senza infrangere nessuna legge, ma con un insostenibile carico di ipocrisia, perché noi non deriviamo queste cellule, ma lasciamo fare questa parte ad altri che ritengono immorale questa parte, la lasciamo fare agli altri) e poi importiamo i loro prodotti importantissimi e nei nostri laboratori e nelle nostre università pubbliche

oggi quelle cellule staminali embrionali umane sono in sperimentazione clinica per il morbo di Parkinson, dopo aver passato studi, verifiche e validazioni di ogni tipo in vent'anni di ricerca. *(Applausi)*. Io spero che se ne parlerà - vorrei far questo - a fine novembre qui in Italia, non solo per il morbo di Parkinson, ma anche per il diabete e per la degenerazione della macula dell'occhio. ricerche che hanno un carico emotivo, morale, tecnico, scientifico importantissimo, perché sono dedicate alle persone e a generare speranze per quei malati e quelle famiglie che evidentemente queste speranze non possono crescersele da sole. Invece, anziché essere qui a festeggiare per la liberazione della scienza da un divieto alla ricerca scientifica ideologico e ipocrita, oggi siamo qui a discutere l'allargamento della punibilità di scelte riproduttive compiute da cittadini italiani in Stati a noi prossimi in cui queste scelte sono perfettamente legali e regolamentate. La gestazione per altri in forma solidale, infatti, è legittima, come sappiamo, in Paesi come Olanda, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Grecia, Portogallo, Gran Bretagna, Ucraina, molti Stati degli Stati Uniti e Canada. È una pratica, quindi, seguendo la logica, che di tutta evidenza non può essere considerata come un reato con un disvalore sociale universale. Qualunque cosa si pensi legittimamente di questa scelta, io faccio fatica a comprendere come si possa paragonare la gestazione solidale alla stregua di reati gravissimi che, questi sì, evidentemente hanno una portata universale: penso alla pedofilia, al terrorismo o ad atti di genocidio. Colleghi, io non sono un'esperta, ma leggendo la documentazione tecnica a corredo di questo disegno di legge sono molti ed evidenti i problemi (già venivano citati) che nasceranno in concreto dalla norma che stiamo introducendo e con queste premesse è certo che ancora una volta i tribunali di ogni ordine e grado saranno chiamati a giudicarne l'applicabilità, compatibilità con la disciplina europea, ragionevolezza e forse anche costituzionalità. Ebbene, qualunque sia l'esito di questa attività, il rischio è di essere di fronte ad un nuovo manifesto ideologico, che d'altronde da sempre connota la legge n. 40 del 2004, piuttosto che alla volontà di affrontare razionalmente un tema che dovrebbe vedere nella libertà e autodeterminazione delle persone e nel benessere psicofisico del minore, in qualunque circostanza sia venuto alla luce, la nostra stella polare. In questo contesto, non posso che esprimere il mio voto fortemente contrario al disegno di legge in

attenti più di altre volte alle vite concrete delle persone coinvolte, parlarsi e non fronteggiarsi, soprattutto quando si legifera su come si viene al mondo, sull'inizio della vita. Siamo tutti nati da donne, come il femminismo ci insegna, ma diverse possibilità sono aperte riguardo al modo in cui questo oggi è possibile

che rende mute le relazioni e le pratiche sociali che portano alla vita. Lo stesso vale per il fine vita, così difficile da affrontare, come è noto, nonostante i richiami della Corte. Qui invece tutto pare urlato e si vuole piantare una bandierina ideologica che chiude ogni possibile discussione e rimanda a mai la vera priorità su cui pure la Corte costituzionale ci ha richiamato: i diritti delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali. Oggi però siamo chiamati ad altro e davvero questo disegno di legge è l'ennesima arma di distrazione di massa di questa maggioranza per non parlare dei problemi di questo Paese, del bilancio che ci aspetta, delle difficoltà delle famiglie e dei ritardi che stanno mettendo a rischio l'attuazione del PNRR. Parliamo sapendo che questo tema della gestazione per altri è complesso e suscita dubbi e dibattito. Esistono opinioni diverse pure all'interno del mio partito, anche se su questo disegno di legge la contrarietà è condivisa. Qui ho invece sentito comizi comizi di uomini sulla dignità delle donne e sulla loro libertà. Davvero *timeo danaos et dona ferentes.* Ma qui si parla, in realtà, non di GPA; la vera questione su cui siamo chiamati a votare è il limite fino a cui può spingersi il diritto penale in una democrazia. Lo so che per voi non ha limiti. Non so più quanti reati avete prodotto da quando governate. Qui siamo al panpenalismo universale: aggettivo ambizioso per un qualcosa fin troppo umano, come le norme penali. Francamente avrei sperato in qualche sussulto laico e liberale da parti di pezzi della maggioranza. Altro che garantismo! Il diritto penale può spingersi oltre i confini del proprio territorio solo a condizioni definite, come ha spiegato anche la senatrice Rossomando e gli altri che sono intervenuti sulla pregiudiziale. La GPA, per quanto dibattuta, non rientra in nessuno di questi casi. Siamo di fronte a una scelta ideologica, strumentale, giuridicamente inconsistente e gravemente incostituzionale. Il diritto penale può invece - questo sì, lo farà - mortificare e stigmatizzare scelte procreative che nel Paese in cui sono realizzate sono legittime. Quindi davvero dovremmo riflettere su quest'uso ideologico e simbolico, su quanto sia pericoloso per la democrazia e su dove ci condurrà questo precedente. Infatti, oggi rischiamo di aprire per la prima volta un precedente per cui qualunque condotta potrà essere annoverata tra quelle punibili in nome di questa forza simbolica del divieto. Soprattutto, questa dimensione sovranazionale serve a segnalare la condanna senza appelli della della pratica criminale, con inevitabile criminalizzazione - è stato detto - di chi vi ricorre e, in particolare, stigmatizzazione dei figli di pratica illegittima. Abbiamo già visto all'opera questo intento perché il fantasma della GPA, pur essendo usata soprattutto da coppie eterosessuali, si aggira ogni volta che parliamo della possibilità di riconoscere i diritti delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali.

Lo avete fatto con le circolari contro i Comuni che stavano riconoscendo i figli delle coppie omogenitoriali. Si tratta di un passo indietro, un muro alzato nei confronti di famiglie che tali sono all'estero e che qui non verrebbero riconosciute. Si ritorna, come giustamente ha sottolineato la sociologa Chiara Saraceno, che di famiglia se ne intende, alla discriminazione sulla base del modo di venire al mondo, come succedeva con i figli illegittimi. con i figli illegittimi. Sono stata anch'io una bambina molti anni fa, figlia di genitori separati prima che esistesse la legge sul divorzio e ricordo lo stigma. Frequentavo le elementari e ricordo la crociata contro il divorzio e cosa ha significato quel dibattito pubblico che prepotentemente entrava e giudicava quanto avessi di più caro: mia madre, mio padre, me stessa e mia sorella. A me questo pare un punto dirimente. Non si può parlare di persone e di bambini come merce. A tutti i bambini vanno riconosciuti stato giuridico, genitori e diritti civili. Quello sulla loro origine è un interrogativo irricevibile, se diventa ostativo al riconoscimento dei diritti fondamentali. *(Applausi)*. È questo l'unico effetto vero che avrà questa norma ed è questa la priorità che noi, come legislatori, avremmo dovuto affrontare. Ci sono bambini reali, relazioni, bambini diventati grandi, che questo dibattito lo ascoltano, lo vedono. Invece, questa maggioranza chiude e mette all'ordine del giorno il cosiddetto divieto universale. Chiamatelo come volete: non è un divieto universale, ma questi sono bizantinismi. Il tema è questo: rendere criminale ovunque la gestazione per altri, con questi effetti sulla vita dei dei bambini, delle bambine e di queste famiglie. È una scelta ipersovranista, anche ridicola di fronte a quello che avviene in tanti Stati Stati vicini a noi, anche quelli che non hanno riconosciuto la GPA, ma fanno politiche di riconoscimento e di tutela delle persone nate Questo provvedimento espone famiglie italiane al diritto penale, a processi e a sanzioni. Sarà anche complicato fare questi processi, perché non ci sarà collaborazione da parte di quegli Stati dove, chiaramente, pratica non è un reato. Sarà, soprattutto, angoscia di queste famiglie e di questi bambini: non parliamo, poi, in caso di condanna dei loro genitori. Ecco, questo è il rispetto che voi dimostrate verso le vite e le esperienze che non rientrano nel modello di famiglia e genitorialità da voi ritenuto l'unico possibile: la spada del diritto penale, l'angoscia dell'esposizione alle procure. Ciò non riguarda solo le persone LGBTQ, ma riguarda tutti noi, riguarda l'idea di democrazia che abbiamo, l'idea di diritto che abbiamo. Riguarda la civiltà che vogliamo costruire.

Perché chi lo chiama utero in affitto davvero riduce le donne a un corpo muto, come faceva Aristotele: le donne sono come un uomo sterile; il maschio apporta la forma e le donne sono solo contenitore, corpo e materia. materia. Se noi avessimo avuto lo spazio politico per fare una discussione vera, penso che avremmo dovuto ragionare, nelle differenze che esistono, sul fatto che la maternità surrogata, intesa sempre come sfruttamento delle capacità procreative delle donne, quando è sfruttamento, è una condotta grave. Se, però, questo diventa un divieto assoluto, fino a criminalizzare la consapevole e libera scelta della gravidanza in solidarietà, questo appunto mette in discussione la costruzione dell'autodeterminazione sessuale e riproduttiva delle donne. È un tema aperto, complicato e difficile, su cui ci sono opinioni diverse, ma è di questo che si deve discutere, se si vuole davvero fare fare i conti con la libertà delle donne. Ma questa discussione non si può aprire. Qui c'è solo un'ideologia piantata sulla vita delle persone.

e la stiamo estendendo anche all'estero per i cittadini italiani. Abbiamo visto che la legge vigente ha una grande efficacia in Italia, ma vogliamo sradicare il fenomeno del turismo procreativo. Sempre in punto di diritto, ho sentito molti interventi che richiamavano sentenze della Corte costituzionale. Non so quali sentenza abbiate letto voi, ma c'è una frase di una delle sentenze, la n. 272 del 2017, che descrive la maternità surrogata e dice che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». *(Applausi)*. Come vede, senatrice D'Elia, non lo diciamo noi, lo dice quella suprema Corte che voi avete sbandierato più volte durante i precedenti interventi.

Prima ascoltavo l'intervento della senatrice che diceva che lei ha vissuto lo stigma sociale, in quanto bambina figlia di genitori separati; ma un diritto non glielo ha tolto nessuno e quel diritto era di avere la mamma, di avere il papà. Io adesso vorrei analizzare bene questo fenomeno, perché io sono stanca di sentir dire a noi che non vogliamo proteggere il bambino. *(Applausi)*. Se c'è un genitore biologico, quel genitore biologico può trascrivere all'anagrafe quel bimbo, che avrà la sua carta di identità, che avrà il suo codice fiscale, che sarà uguale a tutti gli altri bambini Basta con questa retorica, falsa, opportunista! *(Applausi)*. Invece andiamo a guardare che cosa tutela veramente il bambino. Il bambino è un oggetto di diritti? È un oggetto di diritti altrui, che può essere acquistato, venduto, prodotto, come un prodotto su Internet che si ordina e magari si decide che lo si vuole biondo con gli occhi azzurri? O è un essere umano, o è quello che noi crediamo che sia - ed è il principio a fondamento di questa norma - ossia un soggetto di diritti. Quel nascituro è un soggetto di diritti. Allora siete voi che infierite sul soggetto più debole di questa storia, che è quel nascituro, che crescerà nel ventre, ma di chi? Di una madre, la madre con cui si crea quel rapporto preziosissimo, unico, unico, che sentirà battere il suo cuore, che sentirà i primi scalci di quei piccoli piedini che crescerà nel proprio ventre. Non avrebbe il diritto di sapere, a prescindere dai contratti, chi è quella madre? C'è un altro motivo per il quale siamo felici di votare questo disegno di legge: perché protegge - questa sì - la dignità della donna. Senatrici, ma come? Anni di battaglie per la valorizzazione della donna che cosa stanno portando? A trasformare quella donna, priva di dignità, a mendicare dei soldi per poter essere ridotta a un forno nel quale si va a mettere una vita per poi togliergliela in cambio di denari? Questa per voi è la civiltà? Questa è la libertà della scienza di cui altri parlano? Beh, io credo che la libertà finisca dove comincia la libertà altrui, dove comincia la libertà di un nascituro di sapere chi è la sua mamma, chi è il suo papà e di quella donna che non deve vivere lo sfruttamento. Ho sentito parlare di GPA. Cos'è la GPA? Il Gran Premio d'Argentina? Ma abbiate almeno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: la maternità surrogata, l'utero in affitto. Questo è! Abbiate il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. Per noi la maternità resta unica, insostituibile, quel rapporto preziosissimo e, come molte cose preziose, delicato. Ho ascoltato una volta due padri che mi raccontavano la loro esperienza nell'avere ordinato i loro bambini in America e si lamentavano. Sapete di cosa si lamentavano? Del fatto che fosse costata un pochino troppo quell'operazione. Era costata troppo, perché non avevano previsto che la donna avrebbe dovuto subire un parto cesareo e quel parto cesareo gli era costato di più. Io ho provato tanta pena per quella donna, di cui tutti si disinteressavano, anche del fatto che avesse subito quel parto cesareo. cesareo. Credo che invece sarebbe rilevante e importante ricordare quella maternità che, come dicevo, è assolutamente unica

Quando qualcuno ci ha detto da quegli scranni "arrendetevi, voi non potete fermare il vento con le mani",

il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare».

mi trovo veramente in imbarazzo ad entrare oggi in questa discussione generale, perché sto assistendo alla fiera dell'ipocrisia, alla fiera dell'ipocrisia, tanto più grave quanto più vergognosa, perché insiste sulla pelle dei bambini e non voglio addentrarmi in tutti gli aspetti giuridici che chi mi ha preceduto ha evidenziato in maniera ineccepibile. Dal punto di vista del merito giuridico della questione, faccio solo riferimento alla sentenza n. 33 della Corte costituzionale, che forse è scappata all'attenzione della collega Mennuni che mi ha preceduto, dove c'è un fortissimo richiamo da parte della Corte costituzionale nei confronti del legislatore italiano, perché strumenti come l'adozione in casi particolari sono dei palliativi a cui si fa ricorso perché c'è un vuoto normativo. Qui sarebbe necessario intervenire con un provvedimento che vada a legiferare su una materia su cui il Parlamento italiano, nelle mani di questa maggioranza, sta continuando a lasciare alla giurisprudenza e ai procedimenti la necessità di intervenire; questo perché non si trova l'adeguato soddisfacimento del superiore interesse del minore ad essere riconosciuto nei suoi diritti di figlio. Questo concetto è rafforzato dall'articolo 8 della Carta europea sui diritti umani, in cui vi è la necessità di far assurgere questo legame di filiazione come riconoscimento giuridico dei bimbi, comunque nati. Tra l'altro, io sono Vice Presidente nella Commissione politiche europee purtroppo ho già assistito a questa sfilata di ipocrisia da parte di diversi esponenti della maggioranza, che in occasione della sottoposizione alla nostra Commissione della proposta di Regolamento europeo sul certificato di filiazione sono venuti esattamente a ripetere questa manfrina.

lo stesso legiferare su un reato che già è previsto come tale nel nostro ordinamento, al semplice scopo di piantare la bandierina dell'universalità di questo reato, fa il paio con i provvedimenti che questa maggioranza ha ritenuto di dover assumere, per esempio, in tema di sanità. In tale settore invece di assumere medici e rafforzare il sistema sanitario è fatto il decreto liste d'attesa, che non ha risolto minimamente il problema delle liste d'attesa e che è pura propaganda elettorale; ad oggi, infatti, come ha evidenziato Gimbe in un recente rapporto, 4,5 milioni di cittadini italiani che rinunciano a curarsi. E siccome tutto si tiene nella narrazione di questo Governo, la maggioranza, invece di intervenire rispondendo alle esigenze vere dei cittadini che hanno bisogno di un salario minimo, perché sotto i 9 euro l'ora è sfruttamento e non è lavoro, si si inventa una legge delega al Governo con cui mette in lista d'attesa le esigenze di 3,5 milioni di lavoratori italiani che purtroppo non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. posso inoltre non ricordare il tripudio di demagogia e di propaganda che riguarda il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari italiani e delle famiglie italiane che vanno al supermercato e non riescono a riempire il carrello della spesa. Qui abbiamo avuto un tripudio: il carrello tricolore, il *bonus* befana, il *bonus* Natale. Vi do un'idea per il prossimo *bonus*: chiamatelo direttamente "*bonus* pesce d'aprile", perché la sostanza reale di questi provvedimenti è la presa in giro delle reali esigenze dei cittadini. Non ruberò altro tempo, perché la maggioranza, da questo punto di vista, di fronte alla realtà si volta dall'altra parte, come insegna a fare loro la Presidente del Consiglio, che si lava le mani su questioni sicuramente di impatto non solo nazionale, ma anche internazionale, come abbiamo avuto modo di ricordare ieri, per esempio, per quanto riguarda la situazione dei conflitti esteri. di fronte alla realtà di questa maggioranza, che ipocritamente parla di piedini che scalciano nella pancia della mamma, come ha appena finito di fare la collega Mennuni, mi chiedo: come mai, quando Giorgia Meloni è stata invitata da Elon Musk a ritirare il premio in America, non si è rivoltata e indignata verso di lui dicendogli "delinquente reo confesso che non sei altro, il tuo premio tienitelo insieme a quelle due gravidanze di maternità surrogata che oggi ti fanno padre"?

questo mio suggerimento. Laddove l'anno prossimo l'ambito premio di Elon Musk dovesse essere conferito al senatore Romeo,

Signor Presidente, senatori colleghi, direi che la prima cosa che bisognerebbe richiedere a tutti noi, quando si affrontano questi temi, è una cifra maggiore di umanità. perché è veramente difficile affrontare questioni che riguardano la sofferenza delle persone, da tutti i lati: da quello di chi vuole essere genitore ma non riesce a diventarlo; da quello decide o in modo più o meno libero - poi entrerò su questo tema della libertà - di essere una madre gestante. Secondo me, non è una scelta così semplice come può sembrare. C'è poi il tema dei bambini e dei bambini non riconosciuti. Credo che l'umanità servirebbe a tutti per ricalibrare i nostri interventi e cercare di dare un contributo del Parlamento più alto rispetto a questi temi. Ciò poi ci aiuterà nel futuro ad affrontare quello che non abbiamo fatto oggi, cioè i nodi reali e concreti di quello che accade attorno al variegato ed estremamente eterogeneo mondo delle gravidanze e del desiderio di genitorialità. Vorrei sgomberare subito il campo da un equivoco evidente, da questo dibattito così aspro, soprattutto nella fase delle pregiudiziali, che ha portato, per volontà della maggioranza a mio parere, a essere questa una discussione estremamente divisiva e ideologica, al punto tale che, rispetto a questo provvedimento di Fratelli d'Italia, se una persona come me, ad esempio, ritiene un obbrobrio giuridico l'istituzione di un reato universale di questo tipo, debba essere favorevole alla GPA o alla maternità surrogata (chiamatela come volete). Credo che questo sia un grandissimo errore, perché istituisce un paradosso molto pericoloso e fa di questa una vicenda ideologica, dove tutto viene tagliato a metà in modo netto, quando di cose nette qui ce ne sono sempre di meno. È un paradosso che però è facile per la propaganda politica, che ha voluto sventolare con questo provvedimento una bandiera ideologica, che nulla fa sulle questioni, ancora tutte aperte, del mercato globale costruito intorno a un desiderio sempre più forte di genitorialità. Non fa nulla di ciò che poteva essere fatto sul piano giuridico per quanto riguarda il supremo interesse dei bambini (lo diremo dopo) e non fa nulla sul piano sociale su un tema apertissimo in Italia, come quello delle adozioni, estremamente scomodo; questa è una strada quasi impossibile per gli eterosessuali nel nostro Paese e totalmente impossibile per le coppie omosessuali o per i *single*. Argomento scomodo, che continuiamo a non affrontare e che fa parte del tema del desiderio della genitorialità. Poi c'è il tema sanitario della preservazione della fertilità nel nostro Paese, che è una questione emergente e urgente dal punto di vista sanitario. A sette anni dall'approvazione della norma che ha portato il mio nome, che ha inserito tra i livelli essenziali di assistenza la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa,

a sei inseminazioni in modo gratuito nel Sistema sanitario nazionale (parlo di Sistema, perché è sia nel pubblico che nel convenzionato), ma il costo oggi per queste sei inseminazioni nel privato si aggira intorno ai 40.000 euro; più o meno quanto costa una maternità surrogata in Ucraina *no limits*, cioè con accesso illimitato a inseminazioni e con un sistema molto lontano dai nostri occhi sulla preservazione della salute della donna. Capite quindi che c'è, a a mio parere, un'ipocrisia di fondo perché laddove potremmo agire veramente sugli strumenti a nostra disposizione già presenti nell'ordinamento nazionale o innovando quello che c'è per facilitare la genitorialità di chi oggi vuole essere genitore, non lo facciamo. Facciamo invece una norma penale restrittiva e molto punitiva, come questa, totalmente inutile tra l'altro (poi vi diremo anche per quale motivo), e di fatto non facciamo nulla per scoraggiare un mercato che oggi costa quanto andare a fare un ciclo di procreazione medicalmente assistita in una struttura privata in una qualsiasi città della nostra Nazione (senza ovviamente avere un'assicurazione di risultato). Inoltre non si fa nulla sull'applicazione della legge così com'è oggi, anche nella parte più facile, cioè la punibilità della promozione del commercio. Se navigate su Internet, troverete pubblicità, promozione e commercio di tutto, dai gameti alla GPA, con tanto di contratti di logistica. Mi chiedo come mai, almeno dall'inizio di questo *iter* parlamentare, questa maggioranza parlamentare e governativa, che ha così a cuore questo tema, non abbia perseguito

tutto, in italiano, da strutture italianissime, quindi *contra legem*. Per sgomberare il campo da dubbi o equivoci, vorrei sottolineare che ero e resto profondamente contraria all'uso della maternità surrogata, che ritengo l'ultima delle forme assunte nella lunga storia di sfruttamento della donna, privata della propria libertà di scelta e ridotta a fattrice da un meccanismo mercantilistico legato a logiche di consumo e all'estremizzazione di una cultura neoliberista. e cultura tutto può essere oggetto di scambio e consentito grazie a un contesto sempre più diffuso che tende a sdoganare pratiche lesive della dignità personale, facendole passare per una libera scelta

però a vedere i siti dove si commercializza, ci si rende conto che la maternità surrogata altruistica, se esiste veramente, esiste solo in due Paesi, in Portogallo e in Canada. In tutti gli altri luoghi, anche in Grecia, dove è proibito accedere alla maternità surrogata non altruistica, il listino prezzi è di circa 81.000 euro. Questo è l'ambito, il contesto reale, non ipotetico o teorico, nel quale noi ci stiamo muovendo. Il mio, ovviamente, è un punto di vista personale. Io non parlo a nome del Partito Democratico, ma esprimo la mia posizione su un tema delicatissimo e relativamente nuovo nel dibattito politico e lo faccio da un punto di vista laico e femminile e, se mi permettete - spero che nessuno si offenda

femministe. Ci sono posizioni molto diverse in quest'Aula, sotto certi aspetti anche inconciliabili, trasversali negli schieramenti e anche tra chi ha posizioni comuni su alcuni aspetti, ne troviamo altri in cui la pensiamo diversamente. E non può essere che così, viste la delicatezza del tema del tema e la difficoltà a parlarne in modo sereno e pacato. Invito chi usualmente è meno interessato alla questione a fare semplicemente quello che ho fatto io ieri sera: una semplice ricerca con lo *smartphone*, digitando "come faccio GPA in Europa". Subito compaiono siti delle maggiori agenzie internazionali in italiano con prezzario, assistenza legale, assistenza sanitaria, differenti tipologie contrattuali e soluzioni per tutti i gusti. Emerge chiaramente che il mercato è differente tra Europa, USA e Asia, differente per eterosessuali e omosessuali, e vorrei dire che la maggioranza delle coppie, il 90 per cento di esse, è eterosessuale; sono coppie eterosessuali molto benestanti che accedono a un servizio essendo spesso fuori dall'età in cui nei loro Paesi è consentito accedere alla procreazione medicalmente assistita eterologa, e cioè dopo i quarantasei anni o i poi lo strano caso della Grecia di cui vi ho già parlato. I luoghi più gettonati sono quelli dove fai quello che vuoi e la gestante è di fatto privata di qualsiasi libertà una volta firmato il contratto; la questione centrale di chi sostiene la pretesa di poter disporre di un altro essere umano. Una donna e un neonato non possono essere oggetto di una rivendicazione la sua salute, la sua integrità psicofisica, compreso l'aborto, l'abbandono del bambino, se non perfetto o se nel frattempo i genitori decidono di non volerlo più. La La cosa che fa più impressione è che la madre gestante non può cambiare idea, non è più padrona del proprio corpo in virtù di un contratto. L'essere madre non è più una scelta della donna. Sono secoli che discutiamo di cosa sia la libertà e solo da poco lo facciamo in merito alle donne e da pochissimo sul rapporto tra maternità e libertà. E per un estremo paradosso questa oggi viene confusa ad arte con la disponibilità, come se disponibilità a fare qualcosa e libertà coincidessero quando in tutte le nostre azioni cerchiamo di capire come e quando la libertà sia condizionata da fattori esterni, come ambiente, istruzione e povertà, e come questa sia compressa o ampliata da questi fattori. E quindi è libertà quella in cui il nostro corpo e la capacità procreativa diventano oggetto di uno scambio commerciale? commerciale? Personalmente mi sono scandalizzata per le donne asiatiche relegate nei villaggi più poveri, trasformati, nel decennio scorso, in *factory*. Ma oggi sono molto preoccupata per quello che avviene in Ucraina, dove donne che sono libere scelgono liberamente di sottoporsi alla gestazione, perché questo diventa l'unico modo per sostenere la loro famiglia dal punto di vista economico. A questo punto, quindi, dico che abbiamo tanto parlato di libertà, ma c'è libertà e libertà e sicuramente la libertà di chi è povero, di chi non è istruito e di chi non è libero è diversa da altre. Tuttavia,

ci ha divisi, non ha portato le soluzioni che volevamo. Ma, anche dal punto di vista giuridico, è soltanto un manifesto e lo ha affermato in modo molto chiaro il capogruppo Romeo, dicendo che anche se non funziona, anche se non è costituzionale, serve a dare un segnale.

La Corte costituzionale la ascoltiamo quando e come ci pare. La Corte costituzionale ha tracciato chiaramente il quadro, indicando che si devono contemperare due diritti che a loro volta devono stare in piedi: da una parte, non bisogna sdoganare la pratica della gestazione per altri rendendola di facile attuazione; ma, dall'altra, c'è lo strumento dell'adozione e le adozioni speciali, come sono fatte oggi in Italia, non sono più compatibili con il ruolo di genitorialità. È lì, allora, che bisognava incidere e questa è l'altra occasione persa, quella di costruire un quadro

ho apprezzato i toni di quei pochissimi esponenti dell'opposizione che hanno cercato magari di ragionare sul merito di questa legge, e non semplicemente di trincerarsi dietro le solite accuse di oscurantismo, di ritorno al Medioevo, di totalitarismo, cioè tutto quell'armamentario che quotidianamente da due anni viene rivolto contro questa maggioranza

fa parte integrante di quanto da noi annunciato in campagna elettorale - quindi siamo stati votati come coalizione anche per portare avanti

della pratica di utero in affitto in Italia e la estende ai cittadini che lo fanno all'estero. Non è una legge contro qualcuno: è una legge in difesa di qualcuno. È una legge, innanzitutto, in difesa dei minori, dei bambini - checché se ne sia detto in quest'Aula - perché difende il loro diritto sacrosanto, il loro diritto naturale, ontologico di avere un padre e una madre, di avere la possibilità di difendere quel legame, che non è solo biologico ma è anche emotivo, con la madre che gli ha dato la vita. Quel minore non può essere oggetto di scambio, ma soprattutto non può essere oggetto di mercato. È stata richiamata la possibilità della gestazione solidaristica,

ed è una pratica rispetto alla quale noi, con questa norma, non diamo un segnale, ma costituiamo un tassello importante nel nostro diritto non accettando

Ci sono - credo - 170 Paesi nel mondo, ci sono una serie di pratiche per noi assolutamente illecite, non legittimate, illegali:

che discriminano per legge gli omosessuali; ci sono Paesi del mondo che applicano applicano la *sharia,* o comunque le leggi di diritto religioso, nell'ambito del diritto dello Stato. Tutto questo in Italia non accade, non lo ammettiamo. Personalmente, sono tra coloro i quali, per esempio, sono contro la pena di morte,

viene considerata oggettivamente disumanizzante. Noi non vogliamo contrastare il diritto ad avere figli, ma vogliamo dire che il diritto del minore è prevalente,

che fino adesso sono stati frutto di maternità surrogata, non rimangono figli di nessuno: la legge italiana, comunque, li tutela. Togliamo questa narrazione, questa sì demagogica e oggettivamente falsa. Raccontiamo che noi da domani metteremo un ulteriore tassello per contrastare la pratica della schiavitù commerciale, che in molti Paesi è concessa. *(Applausi)*. Diciamo che stiamo compiendo un piccolo atto di civiltà e che lo fa il Parlamento con un proprio atto: non il Governo con un atto d'imperio, ma il Parlamento, che dibatte, discute e va avanti.

finale. Vorrei citare non un pensatore cattolico, conservatore o di destra, ma un autorevole esponente del mondo femminista. Sylviane Agacinski, accademica di Francia, femminista e filosofo, dice che abbiamo a che fare non con gesti individuali motivati dall'altruismo, ma con un mercato procreativo globalizzato nel quale i ventri sono affittati. È stupefacente e contrario ai diritti della persona e al rispetto del suo corpo il fatto che si osi trattare una donna come un mezzo di produzione di bambini. Per di più, l'uso delle donne come madri surrogate poggia su condizioni economiche sempre più diseguali. I clienti, che appartengono alle classi sociali più agiate e ai Paesi più ricchi, comprano i servizi dalle popolazioni più povere sul mercato neocolonialista. Questo non l'ha detto un pericolosissimo esponente del pensiero della destra retrograda, oscurantista, cattolica. C'è tanta gente che ha a cuore realmente quel in cui crede, ossia i diritti delle donne, che viene dalle battaglie femministe e che queste cose le ha scritte. Sono state richiamate prima delle prese di posizione importanti anche di associazioni femministe. Su questo tema mi sembra che una norma semplice, chiara e precisa dal punto di vista legislativo sia intervenuta con chirurgica efficienza a porre un argine importante a delle pratiche che oggettivamente stanno debordando. Veniva richiamata prima - e sono d'accordo che andrà affrontata in ulteriori provvedimenti - la pubblicità incredibile che c'è di questo mercato. mercato. Questo Governo e questa maggioranza hanno cercato e cercano costantemente con umiltà, ma anche con determinazione, di impostare l'azione di governo a favore delle famiglie, della natalità e dei minori non per un motivo semplicemente ideologico,

una battaglia ideologica *sic et simpliciter* tra destra e sinistra, tra conservatori e progressisti, e dovremmo anche discutere di quali progressisti. Siamo qua per difendere il diritto delle madri a non essere pecore da gregge e il diritto dei bambini di non essere agnellini da commerciare. Questo noi stiamo facendo oggi.

che dal vocabolario di tutti i membri di questa maggioranza sembra essere improvvisamente scomparsa. La parola solidarietà, solidarietà, in tutte le sue declinazioni, trasformazioni in aggettivi, avverbi e tutto quello che volete e che ci consente la grammatica italiana, è scomparsa dai vostri dizionari. Eppure, Eppure, è uno dei concetti base su cui si fonda la nostra Costituzione. Non vogliamo che nessuna donna sia costretta, per ragioni di sudditanza psicologica, morale ed economica, a vendersi e a dover subire una gravidanza non voluta. però tutto un ventaglio di emozioni, possibilità e disponibilità che va al di là delle pratiche commerciali. Come ho già avuto modo di dire in quest'Aula, credo che questo tema possa essere facilmente affiancato affiancato e sovrapposto a quanto avviene nell'ambito della donazione di organi. Anche lì c'è sfruttamento della povertà e delle condizioni di fragilità. E, quindi, ci sono delle regole ben chiare, nei Paesi che si ritengono più sviluppati e più democratici, che stabiliscono quali siano le regole per una donazione solidale, sicura e senza pagamenti commerciali, senza violenze e senza sopraffazione. Non capisco per quale motivo non si possa affrontare il discorso della gestazione per altri con la stessa laicità, in uno Stato laico, disciplinandola in maniera solidaristica. Questo non vuol dire costringere una donna che non voglia sottostare a una pratica di questo genere a farlo. nel modo in cui agite voi, costringete una donna, che invece vuole sottoporsi a questa pratica, a non farlo. State facendo voi una violenza sul corpo delle donne. Voglio essere più esplicita.

perché volete ammantarvi di un'aura che poi, in realtà, non avete. L'obiettivo è quello di perseguire la pratica laddove venga svolta

ragionevolmente sicuri che sia nato per gestazione per altri e, quindi, fate scattare la persecuzione legale. Invece, se davanti all'ufficiale di anagrafe arriva una coppia eterosessuale, su che base scatta il procedimento? Questo punto non è chiaro e vorrei che lo spiegaste ai cittadini italiani. Oltretutto, dovreste anche spiegare che, nel 90 per cento dei casi in cui si ricorre a gestazione per altri, a ricorrervi sono coppie eterosessuali. Questo perché esistono difficoltà nella procreazione all'interno delle coppie eterosessuali: udite, udite! Che notizia! Sembra che nessuno se ne sia accorto. Di sicuro non ve ne accorgete voi, che non fate altro che parlare di denatalità, supporto alla famiglia, sostegno alla maternità. Quelli contrari ai bonus nella legge di bilancio che state per varare hanno tirato fuori una cosa di berlusconiana memoria, il bonus ai nuovi nati: quanto siete originali! Eppure, Eppure, a quelle donne che, per una ragione fisiologica, che è la sindrome di Rokitansky, non possono autonomamente portare avanti una gravidanza, anche se hanno le ovaie, ma possono mettere a disposizione i loro ovociti, il loro patrimonio genetico per avere un figlio, che sia anche anche biologicamente loro, questa cosa la vietate, Quelle donne le discriminate. Quindi, che maternità volete salvaguardare? Come Come la volete fare la lotta alla denatalità, se, in ogni cosa che fate avete un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne? Le discriminate quando aumentate l'IVA sui prodotti dell'igiene intima femminile. Le discriminate quando aumentate l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Seggiolini pannolini, latte in polvere: per tutti questi prodotti le donne italiane devono pagare di più. Però, a parole siete a favore dell'aumento della natalità. Aumentate l'assegno unico: adesso, forse, riusciamo a toglierlo dal calcolo dell'ISEE. Dico forse, perché non è ben chiaro come lo vogliate fare. È più di un anno che annunciate questa misura e ancora non è entrata in vigore. Quindi, siete malati di "annuncite" di sicuro. Poi, nella pratica, vi dimenticate i decreti attuativi. Vi dimenticate di mettere le gambe alle norme che proclamate ai

per calunnia un parlamentare, cosa che sapete benissimo nei fatti non si può fare, noi quereleremmo il senatore Malan per queste affermazioni fatte in quest'Aula. Noi non vogliamo commercializzare in nessun caso i bambini. Siete voi che fate propaganda sulla pelle dei bambini. Se non fosse così, non vi opporreste alle adozioni delle coppie omosessuali. Se non foste discriminatori, razzisti, omofobi - e chi più ne ha più ne metta - nei confronti delle coppie omosessuali, allora li avreste approvati gli emendamenti che sono stati depositati a questo disegno di legge per favorire l'adozione per casi speciali. *(Applausi)*. E invece no, per la vostra furia oscurantista di persecuzione di chi è diverso da voi e la pensa diversamente da voi, voi i bambini non li tutelate. O meglio, li volete tutelare prima che nascano e prima che siano effettivamente dei bambini, quando magari sono ancora un ammasso di cellule nel grembo di una donna; ma poi, una volta che sono nati, li discriminate e non consentite che vengano iscritti all'anagrafe come figli dei genitori che li hanno voluti *(Applausi)* - sì intensamente - e li vogliono crescere con amore. con amore. Siete profondamente ipocriti in tutti i provvedimenti che varate. Si vede una ipocrisia sottesa, un finto buonismo che emanate da tutti i pori. Lo dimostrano le dichiarazioni fatte in quest'Aula: un collega di Fratelli d'Italia - adesso non ricordo chi fosse - ha detto che tra madre e figlio durante la gestazione si instaura un legame profondo e indissolubile. Questo è vero, credo, nella maggioranza dei casi per fortuna, ma non in tutti. Non è assolutamente così sempre: ci sono donne che deliberatamente decidono, dopo aver portato avanti una gravidanza, di lasciare il bambino che è nato in ospedale, non riconoscendolo. Se voi foste coerenti con le parole che avete appena pronunciato, porterete avanti il disegno di legge, depositato alla Camera, sul diritto alle origini dei bambini che poi vengono dati in adozione, non riconosciuti alla nascita, perché oggi quei bambini devono aspettare cent'anni dalla nascita per sapere quali sono le loro origini e da dove arrivano. Allora, basta: squarciamo questo velo di ipocrisia. Se volete davvero salvaguardare i bambini, fate finalmente qualcosa di serio in questo caso. Altrimenti

durante la discussione generale questo provvedimento, ho sentito molti appelli alla pacatezza, al ragionamento, alla civiltà dello scambio. Queste sono buone regole del dibattito parlamentare. Però, mi perdoni, Presidente: quando si discute di temi etici è giusto essere pacati ed equilibrati; quando c'è invece un attentato alla libertà delle persone; quando si utilizza il diritto penale come una clava; quando si varano norme che sono scritte per essere discriminatorie, perché il portato di questa legge vuole dare un messaggio di discriminazione al Paese e vuole vittimizzare una parte del Paese, che ci si scaldi è del tutto normale, che la passione politica prevalga è del tutto normale. Quindi, io rivendico il calore del mio intervento in sede di dichiarazione sulla questione pregiudiziale di incostituzionalità, perché penso che la manovra astringente delle libertà personali che sta facendo questo Governo richiede di essere manifestata in quest'Aula con tutta la passione e il calore che sono necessarie. L'uso di questo diritto penale deve finire qui: non è più tollerabile. Io questo lo dico e lo ripeto. Dopodiché, dobbiamo anche demistificare e chiarire questo dibattito. La destra sta cercando di portare qui dentro un dibattito sulla GPA, sulla gestazione per altri. Noi non ci stiamo occupando di questo. Va detto chiaramente che la gestazione per altri in Italia è vietata: punto e basta. È vietata dalla legge n. 40, tant'è che non era necessario in alcun modo fare una nuova legge, perché il punto è che il dibattito sulla GPA in questo momento non è aperto. Ci sono persone favorevoli e persone contrarie. Le dico subito che intervengo in discussione generale e non in dichiarazione di voto, per avere la libertà di dire quello che penso, perché so che nel mio Gruppo ci sono sensibilità diverse. Dunque, non farò la dichiarazione di voto perché intendo intervenire in discussione generale con la massima delle libertà. E allora, con la massima delle libertà, dico che questa norma, e in genere il pensiero politico che c'è dietro la legge che stiamo approvando, sono negativi per i bambini, per le donne e per una particolare minoranza di questo Paese, che sono gli omosessuali maschi. È negativo Si attaccano i bambini: questo è chiarissimo. C'è un pensiero politico che va al di là di questa norma, perché in questo Paese alcuni sono bambini a diritti diminuiti. Quando il Ministero dell'interno, attraverso un prefetto, fa una circolare ai sindaci per dire di non trascrivere degli atti di nascita, crea dei bambini a diritti diminuiti. Signor Presidente, io me ne vergogno *(Applausi)*. Mi vergogno di vivere in un Paese dove ci sono bambini ai quali lo Stato nega la genitorialità. Avere due genitori è un punto di forza per il bambino; avere due eredità, avere due persone che ti vengono a prendere a casa, avere quattro nonni è forza per il bambino. Ma la Repubblica italiana

C'è un tema sulle donne. Signor Presidente, la mia opinione personale - come ho detto, intervengo in discussione generale per questo - è che il dibattito sulla GPA nasconda molte altre cose. Nasconde il fatto che lo Stato vuol dire alle donne cosa possono e non possono fare del proprio corpo: questo è il pensiero. Ci fosse anche una donna, una e una soltanto, che decidesse liberamente di dire a un'amica o una sorella «avrò questo bambino per te», c'è lo Stato che le dirà: «guarda, ragazza, tu non capisci abbastanza, tu non sei abbastanza libera. Te lo dico io. La dignità del tuo corpo mi dice che tu non lo puoi fare, anche se lo vuoi». vuoi». Si introduce sempre questo pericolosissimo e pelosissimo concetto della dignità. Chi la decide la dignità? Quando un malato chiede di accedere al suicidio medicalmente assistito, noi diciamo che siamo per la dignità della vita. Ma la dignità della vita di quel malato la decide quel malato; non la decidiamo né io, né lei, né quest'Assemblea, signor Presidente. Lo Stato dovrebbe fare una e una sola cosa: determinare che la donna che ha deciso di prestarsi alla GPA lo faccia in modo libero da costrizioni e dal bisogno, che è esattamente quello che c'è scritto nel disegno di legge dell'associazione Coscioni, presentato a mia prima firma, perché io penso che quello che si debba fare non è vietare, bensì regolamentare. Vogliamo evitare gli abusi? Facciamo una legge che dica che si può fare questo, ma quest'altro non si può fare. Tant'è vero, signor Presidente, che in quella legge io scrivo che costringere una donna in qualsiasi modo, anche per ragioni di bisogno economico, va equiparato alla riduzione in schiavitù. L'ipocrisia generale è che noi condanniamo questo reato con un massimo di due anni di reclusione. Allora, se sono due anni, così grave non è: è un reato che si dice La donna che viene costretta va protetta con vent'anni di reclusione, e non due. *(Applausi)*. Ma la donna che decide liberamente non deve mai avere la Repubblica che le dice: «donna, non sei in grado di decidere per te, te lo diciamo noi». Quanti maschi ci sono in quest'Aula? Le leggi le facciamo ancora noi maschietti e andiamo dalle donne a dire cosa possono fare. Io sono un uomo del secolo scorso e sono rimasto a quella bellissima frase, quando le femministe andavano in piazza e dicevano: «L'utero è mio e me lo gestisco io». Ebbene, lasciamo che siano le donne a gestirsi il proprio utero. *(Applausi)*. Se in questo Paese una donna può legittimamente decidere di partorire e abbandonare suo figlio e immagino e spero che nessuno di voi voglia toglierle questo diritto - una donna ha anche il diritto di decidere di prestarsi per motivi solidaristici, per dare il figlio che ha avuto per motivi nobili. poi una terza minoranza, quella degli omosessuali maschi. Oggi il senatore Verini ha detto che in questo Parlamento c'è omofobia. Ma questo Paese è intriso di omofobia, signora Presidente. Non lo dico come un'offesa, lo dico come una constatazione. L'omofobia è l'idiosincrasia per le persone omosessuali. Noi pensiamo ancora che gli omosessuali non siano come gli altri; nel fondo della testa di molti qui dentro c'è che due uomini e due donne non sono in grado di tirar su dei bambini. E la dimostrazione è che questo è l'unico Paese dell'Europa occidentale dove non riusciamo non dico a introdurre il matrimonio egualitario, ma neanche a parlarne. Non si può: tutti contrari. *(Applausi)*. Io ho depositato un disegno di legge e non riesco neanche a farlo calendarizzare, da nessuno.

che vieti l'odio omofobico e transfobico, non la si riesce a fare; non si riesce a fare una legge contro l'odio. Ma che comunità nazionale è una comunità nazionale che non riesce a dire che l'odio in questa casa non è ammesso, che l'odio in questo Paese non è il benvenuto? Cari colleghi, tirate fuori il coraggio civile di dire che l'odio in Italia non deve avere spazio; sono trent'anni che ci dividiamo su questo. Ma io sono fiducioso, sa, signor Presidente, perché penso che alla fine voi oggi approverete questa legge, ma essa sarà destinata alla sconfitta. Sarà sconfitta dai giudici. dai giudici. Mi sono dilungato questa mattina sulle tematiche giuridiche, cosa che non ho voluto toccare adesso. La Corte europea dei diritti dell'uomo butterà subito questa legge nel cestino e lo stesso farà la Corte costituzionale. Lei si immagina un tribunale dei minori in Italia o un tribunale che condannerà due persone che hanno avuto un figlio? In che Paese potrebbe mai succedere una cosa del genere? Sarete sconfitti dai giudici e poi sarete sconfitti dal tempo, che lo vogliate o meno, siamo nel 2024 e questo non lo potete fermare in nessun modo, non potete portarci al Medioevo. *(Applausi)*. Non è possibile, perché il progresso umano è una linea

perché quando ci sono persone che decidono di avere un figlio e che magari sono aiutate da una donna che, spinta dalla solidarietà e dall'amore, decide di realizzare quel progetto, quel progetto ha una forza che spiana le montagne. Per cui, se pensate di riuscire a sconfiggere l'amore, sappiate che siete destinati a perdere.

Signora Presidente, intervengo per dichiarare la nostra contrarietà all'introduzione del reato universale sulla maternità surrogata. L'idea stessa di introdurre un reato universale, ovvero perseguibile nei confronti di un cittadino italiano anche all'estero, anche in quei Paesi in cui questa condotta è legale, è un'aberrazione giuridica che credo verrà dichiarata incostituzionale dalla Consulta e credo che sarà censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione europea. L'idea di reato universale dovrebbe essere utilizzata in casi straordinari, serve per punire i criminali di guerra, non chi diventa genitore. Ma anche nel merito del provvedimento voglio manifestare la mia personale contrarietà. Ritengo che sia assolutamente doverosa e necessaria una forma di regolamentazione che tuteli la dignità delle donne contro la mercificazione del corpo per fini riproduttivi, contro il turismo procreativo, contro l'idea che essere genitori sia solo una questione di prezzo o di costo, ma regolamentare è una cosa, criminalizzare il desiderio di genitorialità e un'altra. Così facendo, state discriminando e punendo le famiglie LGBTQIA Plus, le famiglie arcobaleno, che sono ricorse a questa pratica. Così facendo, state punendo e discriminando le coppie italiane, le famiglie eterosessuali che non riescono ad avere figli e che devono ricorrere a questa pratica. Ricordatevi che esiste la pratica della gestazione per altri volontaria, quando la donna genera un figlio per consentire ad altri di avere la gioia della genitorialità senza alcuno scambio di denaro. A proposito di denaro, il senatore Romeo nel suo intervento ha citato spesso l'espressione «ricchi committenti». Quanta ipocrisia, quanto poco coraggio! Perché non dire un nome e un cognome? Quando parlava dei ricchi committenti, probabilmente si riferiva a Elon Musk, oggi dovrebbe essere considerato un criminale che andrebbe punito in Italia con la reclusione da sei mesi a due anni. Diteglielo questo mentre gli chiedete di investire i soldi nelle infrastrutture digitali in Italia.

ad un altro grave errore che avete commesso - e arrivo alla conclusione - quando non avete voluto votare a favore del regolamento europeo per il riconoscimento dei figli fuori dai casi di adozioni speciali. Bisognava tutelare lo *status* giuridico dei minori, per evitare che le colpe dei padri potessero ricadere sui figli, ma non avete voluto il coraggio di approvarlo perché travolti dal furore ideologico proprio contro la gestazione per altri, contro le famiglie omosessuali. Questa è la verità per la quale allora non abbiamo approvato questo regolamento e oggi ci troviamo ad approvare questa norma. Quell'errore di ieri, insieme a questa votazione di oggi, credo che siano - al momento - due delle pagine più tristi e oscurantiste di questa legislatura.

Signora Presidente, io vorrei mantenere un comportamento calmo e pacato, come alcune colleghe e colleghi prima di me hanno tenuto e come i colleghi della maggioranza ci hanno raccomandato. Devo dire che, però, in questo caso potrebbe venirmi anche molto semplice, perché purtroppo le telecamere del Senato non possono inquadrare l'ala della maggioranza, ma vedrebbero che i banchi sono assolutamente vuoti, certificando l'assoluto disinteresse per un tema così cruciale, che ha un impatto così fondamentale sugli aspetti più profondamente umani dell'esistenza

la controparte. Eppure è difficile mantenerlo, perché mantenere un comportamento pacato sarebbe come accettare di prendere parte ad una messa in scena; sarebbe accettare di dire che non è vero che c'è quel carico di ipocrisia, di ideologia e di strumentalizzazione intriso profondamente in questa norma. Se io mantenessi Se io mantenessi un tale atteggiamento, sarebbe ipocrita da parte mia e sarebbe un tradimento del mio mandato, perché è sotto gli occhi di tutti che questa è una norma ipocrita, ideologica e strumentale. Infatti, c'è un'immagine che continua ad aggrapparsi alla mia mente ed è quella di una signora dai biondi boccoli ed il sorriso estasiato che in quel di Washington riceve un premio. Lei è la nostra Presidente del Consiglio, lui è Elon Musk, che la premia

quell'uomo sia anche il padre non di uno, ma di ben due figli ottenuti attraverso la maternità surrogata. Nessuno della maggioranza, nessuno dei compagni di partito di Giorgia Meloni ha avuto un sussulto di coscienza per dirle:

io il motivo. La distinzione vera che fa questa maggioranza e questo Governo non è neanche tra coppie eterosessuali e omogenitoriali, ma è una distinzione molto più profonda della società,

provvedimento. Abbiamo dovuto anche assistere all'intemerata del senatore Romeo in quest'Aula, con un'accorata quanto incredibile difesa delle donne. da parte del senatore Romeo. Donne fragili, vulnerabili e alla mercé della legge del mercato: guarda un po', alla mercé di quella legge che fanno i ricchi. Ma come pensate di essere credibili quando il vostro eroe è Elon Musk? *(Applausi)*. Come pensate di essere credibili quando, non più tardi della settimana scorsa, avete votato un provvedimento che restringe il limite delle intercettazioni per i magistrati a anche per i reati del codice rosso? E vane sono state le nostre implorazioni di stralciare quantomeno i reati che riguardano la violenza di genere. Ora venite a farci la morale sulla difesa della dignità delle donne, quando non vi siete fatti scrupoli nel mettere a rischio ulteriore le vittime di violenza, pur di perseguire il vostro obiettivo, ossia mettere il bavaglio alla magistratura in modo che non possa interferire nei vostri affari. Non avete credibilità. Non avete credibilità. È per questo che questo dibattito non può essere pacato. Il senatore Malan, rispondendo a quanto da me affermato, ha ribadito nuovamente che nessuno mette in discussione la legge n. Ma voi pensate davvero di poter mentire così sfacciatamente alle italiane? Penso al fondo dedicato alle associazioni antiabortiste perché possano entrare nei consultori e il punto presente nei vostri programmi politici che prevede l'inserimento della tortura per le donne che scelgono di abortire con l'ascolto del battito del feto. Questo dimostra che a voi mancano i fondamenti del diritto e che non siete credibili quando parlate della difesa della dignità delle donne. Siete talmente abituati alla menzogna che, alla fine, siete stati persino costretti ad ammettere in quest'Aula che non state istituendo un reato universale. Lo ha chiarito proprio poco fa il senatore Zanettin, la vostra stessa *leader* e quanto tuttora si legge sul sito del partito Fratelli d'Italia: maternità surrogata, reato universale contro *business* esecrabile. Non avete alcuna credibilità. Come vi ho già ricordato, i reati riconosciuti come universali sono, ad esempio, i crimini di guerra e il genocidio. Ma voi, con la vostra presidente Meloni, non avete proferito una parola contro il genocidio in atto a Gaza, quello sì, reato universale. *(Applausi)*. Non avete proferito una parola contro il criminale di guerra Netanyahu almeno fintantoché si è limitato, si fa per dire, a sterminare civili inermi, donne e bambini, al punto da astenervi su qualunque risoluzione chiedesse il cessate il fuoco, salvo quando la sua ira si è poi abbattuta contro le nostre basi. Volete però bollare come criminali universali due persone che vogliono mettere al mondo un figlio e come frutto di reato quel figlio o quella figlia. Legiferate su persone e storie che neanche conoscete e che, però, non esitate a dipingere come malvage e a mettere alla pubblica gogna. Avete mai pensato di parlare con quei bambini e quelle bambine? Alcuni di loro sono cresciuti, hanno compiuto diciotto anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di poterci parlare. Sapete cosa ha detto Lia, da poco diciottenne? Ha detto che la cosa più brutta, che più l'ha ferita nel profondo, è stata sentirsi dire che lei è un prodotto, prodotto, una merce. Ed è esattamente quello che state continuando a fare anche oggi in quest'Aula. Sembrate non rendervi conto che queste persone esistono e hanno dei sentimenti, ma voi vi rifiutate anche di parlarci. Dite di difendere i bambini, ma in Commissione avete avuto il coraggio di presentare un emendamento. Vi è mancato il coraggio di ripresentarlo qui in Aula, ma in Commissione avete presentato un emendamento che recita, testualmente, che i bambini e le bambine nate da maternità surrogata devono essere messi in orfanotrofio e dati in adozione. Ma quale credibilità avete? *(Commenti)*. Ha poco da ridere, collega. Si vada a leggere l'emendamento della Lega, proprio loro che oggi strillavano in difesa dei bambini. Non siete credibili, perché almeno avreste potuto facilitare le adozioni sia per persone etero che per persone omosessuali. Mi viene in mente l'esperienza di Luca Trapanese. Conoscerete Luca Trapanese e la sua Alba, che dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, come anche

che vi mandano a dire quanto segue: «Care senatrici, cari senatori, siamo Carlo e Christian, due papà che hanno appena rimboccato le copertine ai propri figli dopo aver letto loro tre favole della buona notte. Se solo li sentiste ridere quando gli raccontiamo la storia di Gino, il pinguino birichino, vi accorgereste che non possono essere il frutto di un reato universale, come vorreste farci credere voi oggi. Sapete che, prima di addormentarsi, fanno a gara per trovare le somiglianze con i loro due papà? Sapete che di notte, quando fanno un brutto sogno, vengono nel nostro lettone, perché è lì che si sentono al sicuro? Sapete che ogni anno voliamo negli Stati Uniti per passare del tempo insieme alla famiglia della nostra mamma surrogata? Lei si chiama Krista, una donna straordinaria, che ha scelto liberamente di aiutarci a coronare un legittimo desiderio. Sapete poco di noi, eppure molti di voi oggi sono pronti a relegarci nel girone infernale dei peggiori criminali sulla faccia della terra. Lo stesso girone di quelli che uccidono, spacciano, stuprano, sterminano. I veri criminali universali, mentre noi siamo solo due papà, che ogni giorno cercano di fare del proprio meglio per crescere due brave persone. Parlate di famiglia tradizionale, senza sapere che anche nella nostra famiglia rispettiamo una tradizione: quella di esserci l'uno per l'altro, sempre. Parlate del diritto di un bambino ad avere un padre e una madre, senza sapere che l'unico diritto che conta davvero è quello di avere due genitori che, come noi, non smetteranno mai di prendersi cura dei propri figli. Malgrado non sappiate molto di noi e del nostro percorso, siete oggi chiamati a decidere del nostro presente e del nostro futuro. Per questo, senatrici e senatori, vi chiediamo di fermarvi e di stoppare questo mostro giuridico. Fatelo per le nostre famiglie, che oggi rischiate di condannare ad un futuro di odio e pregiudizio. Fatelo per i nostri figli, ai quali rischiate di spegnere quel sorriso capace di illuminare tutti i buchi neri del mondo. E fatelo per tutti quei bambini e bambine che potrebbero nascere da una scelta d'amore. Perché sì, esiste una via corretta alla gestazione per altri, quando è un gesto libero, volontario e consapevole. Soprattutto, fatelo per voi stessi, perché l'unico vero reato universale di questa proposta di legge è negare la scelta d'amore che ha generato la nostra famiglia».

non starò qui a ripetere argomenti che descrivono la mostruosità giuridica di questo provvedimento o a sottolineare come, di fatto, discrimini le coppie omosessuali. Io voglio qui introdurre una nuova dimensione, di cui finora non ho sentito parlare, cioè la dimensione della malattia. La sterilità, signori, è una malattia. Ci sono donne che nascono senza utero e perfettamente in grado di produrre gameti. Ci sono donne che hanno alterazioni morfologiche dell'utero, che impediscono loro di avere una gravidanza. Ci sono donne che hanno tumori dell'utero, alle quali deve essere asportato. Ci sono donne che vanno incontro a chemioterapia,

all'estero rientrano in questa casistica. Noi qui stiamo licenziando un provvedimento che prevede il reato universale per un'opzione terapeutica, perché la GPA, nel caso della sterilità, è un'opzione terapeutica come tutte le altre e vi ricordo che la Costituzione garantisce le cure in caso di malattia. Quindi, noi qui stiamo creando una situazione per la prima volta in cui un'opzione terapeutica diventa reato universale. Penso che dovremmo riflettere su questa assurdità e forse l'avremmo dovuta anche sottolineare, al momento della sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Di fatto, stiamo negando a migliaia di persone un'opportunità terapeutica che la scienza e la tecnologia offrono in questo momento e trasformiamo tutto questo in un reato universale. Però, attenzione, vediamo un attimo che cos'è poi la GPA in termini tecnico-scientifici. Altro non è che una donazione temporanea di organo reversibile: questo è dal punto di vista tecnico, quindi è molto assimilabile alla donazione di organo, ma con il vantaggio che, nel caso della consapevolezza e della libera scelta, è totalmente reversibile e noi qui ne stiamo facendo un reato universale. Allo stesso tempo, sempre parlando di organi, non definiamo reato universale il traffico di organi, che invece, quello sì, dovrebbe essere un reato universale, perché quello è un reato che colpisce le persone più deboli ed è una piaga dei Paesi sottosviluppati, come l'Africa e l'India. Dove sta la coerenza di questa maggioranza? Dove sta un provvedimento che definisce reato universale il traffico d'organi? Mostrate la vostra faccia. Voi, di fronte a una vergogna di questo genere, state zitti e punite le donne sterili, garantite dalla Costituzione per la terapia, come dei criminali. Penso che questo è l'argomento su cui tutti noi dobbiamo riflettere e vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso.

solo la mamma può capire, solo quando cresce dentro di te una creatura puoi parlare e solo quando capisci che dal tuo corpo può nascere una nuova vita, la difendi con i denti e non la tratti come un oggetto. Solo se sei donna e capisci che dal tuo corpo dipende una vita, non la tratti come mercificazione. Solo se sei donna e accetti il tuo corpo, il grande dono che ti è stato dato, accetti tutti i cambiamenti che la maternità comporta. Nei primi tre mesi si affermano mutamenti in modo particolarmente evidente: essere incinta significa mettere il proprio corpo temporaneamente a disposizione del nascituro e i cambiamenti fisici sono tanti e a questi mutamenti il corpo reagisce con sintomi in parte spiacevoli. Questi disturbi legati alla gravidanza danno espressione a un conflitto interiore, perché due esseri convivono in un unico corpo. Ma ci sono donne, donne ricche che non l'accettano, perché il loro corpo cambia. Che cos'è invece la maternità? La maternità è un servizio alla vita, non deve essere un uso del corpo per benefici economici; non è un semplice compito femminile, ma un atteggiamento che tutti sono chiamati a coltivare, partendo proprio dalla consapevolezza che in fondo ognuno di noi ha bisogno di un grembo materno accogliente che ti faccia sentire amato. La nascita di un figlio, se ci pensiamo, è una cosa serissima perché riguarda una vita che viene al mondo e tutti noi ne abbiamo la responsabilità. Dal giorno in cui la donna sentirà che diventerà madre ha inizio un viaggio che non è circoscritto solo al miracolo di dare la vita, ma assume anche un'altra dimensione. La dignità della donna è legata certo alla sua libertà di scegliere, in ragione però del rispetto della sua femminilità, quale dono per lei e per l'intera società. La donna deve sentirsi libera, paritaria, rispettata e tutelata nel vivere questo dono, però spesso la donna è vittima di pretese, di sudditanze passionali che mettono a repentaglio la sua dignità e la sua libertà. Ne sono testimonianza, purtroppo, i numerosi femminicidi. La maternità non è sempre un percorso rose e fiori, tanto più se per anni un figlio non arriva, o se la madre ha la sventura di perderlo dopo qualche settimana o addirittura in corso di gravidanza. La maternità è un percorso difficile, in particolare quando la donna deve confrontarsi con il resto del mondo, deve essere giudicata da familiari e marito, che non è in grado di condividere la totalità delle emozioni. Una coppia che non riesce ad avere figli per motivi naturali, oppure per condizioni di salute di uno dei membri della coppia o di entrambi, dovrà affrontare ostacoli supplementari, tribunali, le complicanze burocratiche dell'adozione, il dilemma etico tra fecondazione artificiale e metodi naturali per la fertilità. È qui che dobbiamo intervenire; è qui dobbiamo aiutare le coppie; è qui che dobbiamo lottare per semplificare; è qui che possiamo incidere sulla denatalità del nostro Paese. Fino alla metà del decennio del 2010, l'India era considerata la capitale mondiale della maternità surrogata, ma ha compiuto negli anni passi in questa direzione. Le nuove leggi hanno limitato i servizi di maternità surrogata, andando direttamente a concederlo alle coppie che hanno almeno cinque anni di matrimonio e, naturalmente, un certificato di infertilità comprovata. Inoltre, la maternità surrogata è stata limitata a un parente stretto della coppia. Anche in questo caso, permetterla solo all'interno di legami parentali può causare gravi condizioni di sfruttamento. I costi altissimi rendono meglio l'idea della realtà che sta dietro questa compravendita di bambini, che molti vorrebbero legalizzare e che questo Governo con questa legge è deciso a combattere, fino a punirlo come reato universale, ossia perseguibile anche se commesso fuori dai confini italiani. *(Applausi)*. Quanto costa la maternità surrogata? In Ucraina, con consulenza legale gratuita, garanzia di trascrizione, test materno, numero illimitato di tentativi e risultato garantito, 70 per cento di riuscita al primo tentativo, senza limiti d'età, costa circa 40.000 euro. A Cipro ci sono addirittura le offerte speciali e piacevoli sorprese. Vi sembra normale? I bambini non si comprano al supermercato. Nessuno considera il bambino? Abbiamo sempre parlato delle donne, abbiamo parlato dei bambini già nati; parliamo invece del bambino in divenire che Ebbene sì, molti studi dimostrano che il bambino in utero percepisce già le emozioni della madre e tra di loro si crea un legame da cui scaturisce la base relazionale futura. L'attaccamento prenatale influisce sullo sviluppo psico-infantile. Cosa accade quando un bambino nasce, ma si sente rifiutato già nel ventre, a causa magari di una violenza, di un atto non voluto oppure, in questo caso, addirittura di una compravendita? Come può crescere questo bambino? Ce lo vogliamo chiedere? bambino? Ce lo vogliamo chiedere? Posso ripetere, se volete, la lettera che Oriana Fallaci ha scritto a Pierpaolo Pasolini, in cui riporta le sue parole dopo che lei gli ha regalato il libro «Lettera a un bambino mai nato». Lui scrive: «Non voglio sapere cosa v'è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità». la maternità». Ci sono persone misogine, ci sono persone che detestano le donne, ma poi pretendono di avere un figlio con la GPA? Vogliono sfruttare le donne per soddisfare le loro esigenze? Come detto in precedenti interventi, dal punto di vista legislativo - lo ha detto anche il capogruppo Romeo - in Parlamento europeo sono state votate tante risoluzioni contro la maternità surrogata. La Cassazione si è pronunciata per questo volevo leggere direttamente quanto scrive: «La maternità surrogata si pone oggettivamente in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante». E ancora: «nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione, che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale e non al mero accordo fra le parti». delle istituzioni, l'impegno che possiamo prendere è quello di educare direttamente alla relazione, l'educazione sessuale di coppia che porta in sé la naturale fecondità. Se la relazione è stabile fra soggetti adulti, l'apertura della vita può essere il concepimento qualificante di quel rapporto d'amore, anche tramite PMA, nel momento in cui ci sono dei problemi. Se questo non è possibile, ci sono le adozioni o forme di aiuto e supporto ai bambini orfani e bisognosi. Concludo, signor Presidente, con una poesia di Alda Merini, perché con l'arrivo di un figlio impariamo così tante cose che a un certo punto sembra che si capovolgano i ruoli, dandoci l'opportunità di crescere come persone più consapevoli,

La poesia dice: «Ti ho generato col solo pensiero figlio e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada. Però sei diventato un'ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo e a mia volta son diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero. Forse, quando morirò, partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo perché figlio, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto. Figlio, figlio mio sognato, figlio ti ho solo pensato non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai». Signor Presidente, Governo, senatrici e senatori, entrando da quella porta, quella lì, saremmo tutti chiamati, anzi richiamati, a svestirci delle nostre appartenenze, quelle religiose, ideologiche, culturali e sociali, e a legiferare e votare esclusivamente nell'interesse delle cittadine e dei cittadini italiani, che ci hanno temporaneamente conferito la loro rappresentanza; Presidente, queste identità non ci abbandonano: ci abitano, ci vestono, ci accompagnano, talvolta ci accecano, ci motivano nel lavoro che siamo chiamati a svolgere in quest'Aula, entrando da quella porta. Illusorio dunque l'appello che qualche ora fa il senatore Verini aveva provato a rivolgere alla maggioranza, a confrontarci con pacatezza nel merito, con coscienza, acribia, senza vessilli, oltre le barricate, su una questione che rileva di ciò che è più intimo dell'intimo e che quindi richiederebbe, almeno virtualmente o virtuosamente, ragionevolezza, assennatezza, ascolto. Non mi è sembrato di sentire - mi sarò distratto, sarò di parte e lo sono questo ascolto, coperto dalle ovazioni e dalle grida che hanno salutato l'intervento del presidente Malan. Lo dico consapevole di non essere tra i più disciplinati in quest'Aula e perché, sempre soltanto poche ore fa, vociavo all'indirizzo del senatore Romeo, invitandolo a uscire da quella che mi era sembrata un'ipocrisia e a dire esplicitamente, con la parresia che la Lega di Salvini e Vannacci rivendicano, chi fosse il reale destinatario della sua intemerata. Peraltro, senatore, credo sia la prima volta che la sento parlare a favore delle donne ucraine. Sono commosso. *(Applausi)*. Entrando da quella porta, Presidente, dicevo che dovremmo ma non ci lasciamo alle spalle chi siamo, nel bene e nel male. Io, ad esempio, e mi scuso di quest'audacia, sono cattolico, apostolico, romano, pure romanissimo (si sente), dunque un cattolico sbilenco, manchevole, sbagliato, ma - e parlo di me e per me - sono per la GPA. So che in Italia, ma non in altri Paesi, è un reato; le leggi vanno rispettate e, se ne si ha la forza e il coraggio, cambiate. E so che secondo il magistero forse, anzi certamente, sarei un cattivo credente, non un buon cristiano, perché non penso che la GPA sia un peccato o una bestemmia. Usciamo allora dall'ipocrisia, questa la mia preghiera. Penso che questa vostra manganellata sul reato universale sia profondamente sbagliata, non fondata dal punto di vista del diritto, crudele nei confronti dei minori, inefficace quanto a monito e deterrenza. Lo hanno detto molto meglio di me i colleghi che mi hanno preceduto e - fatemelo dire - le colleghe del Partito Democratico

dei cattolici; forse credete di mandare un segnale minaccioso alla comunità LGBTQ, tralasciando peraltro il fatto che le coppie che intraprendono questa strada, che ha le sue gioie e le sue afflizioni, siano nella grandissima maggioranza eterosessuali, ma sappiate che anche questi mondi sono più larghi e inquieti, più tormentati di questa vostra difesa pelosa. E poi lo chiedo a lei, Presidente, per suo tramite. Che vi hanno fatto di male, 'sti bambini? *(Applausi)*. Che vi hanno fatto i minori per essere diventati il principale fronte del vostro furore legislativo, il nemico? Giovani da punire, da zittire, da mettergli da mettergli il grembiule, da proibirgli i *social*, i *rave* da vietare, minori da mandare o da lasciare in galera, ragazzi da sbattere in gattabuia perché ecovandali, oggi figli colpevoli soltanto di essere tali,

Ho sentito parlare di natura e di diritto naturale. Mi dispiace, con tutto il rispetto, non mi è parso di scorgere né l'Areopagita né Konrad Lorenz nella filigrana delle argomentazioni. Vogliamo davvero banalizzare la relazione tra desiderio e diritto come fosse uno scontro o aprire una discussione su tecniche e sessualità, sulla laicità? Siamo stati all'altezza? Non è facile per nessuno di noi, colleghi, però mi chiedo perché non si scorgano nel vostro campo queste inquietudini. Perché non c'è questo travaglio? Perché la pensate davvero tutti allo stesso modo? Perché i vincoli di coalizione sono più forti delle coscienze dei singoli? Per il partito? Ma davvero? La disciplina di partito sulla gestazione? Invocate la libertà, mostratela! mostratela! Esercitatela! *(Applausi)*. Un dissenso, uno, anche piccino, a mezza bocca, un equivoco; no, niente. La mamma contro il *gender*, le manette contro l'amore, la schiavitù contro la responsabilità. Sono Sono un credente miscredente, come tutti i credenti, credo, spero; sono un cattolico che sogna un giorno di essere non un cattolico, ma per la GPA, bensì un cattolico e dunque per la GPA, perché al cuore del messaggio cristiano della nostra umanità c'è solo l'amore; questo scandalo, questo errore, niente altro, più più forte del dogma e della disciplina. Ci siamo soltanto noi, deboli della nostra forza. Colleghi, come dice il mio teologo di riferimento, il prete di «Fleabag» ci vuole forza per fare ciò che è giusto. Spero ne abbiamo. Spero che ne siate consapevoli una volta entrati da quella porta e spero siamo tutti quanti all'altezza di questa debolezza,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la legge n. 40 del 2004, la cosiddetta legge sulla procreazione assistita, vieta e sanziona la maternità surrogata solo in Italia. Noi oggi, con questo disegno di legge, siamo chiamati a fare chiarezza e a porre fine a una ipocrisia, perché tutti sappiamo che il divieto è facilmente aggirabile, se si concepisce il bambino dove la pratica dell'utero in affitto è consentita.

la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», ma comporta anche il rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne economicamente bisognose o in condizioni disagiate, che verrebbero indotte ad accettare la gravidanza solo per necessità, dovendo poi consegnare il bambino a terzi.

definirsi progresso sfruttare le condizioni di fragilità delle donne pagandole per portare avanti una gravidanza commissionata da altri. No, Presidente, questo non è progresso, questa è inciviltà. Le donne hanno combattuto tanto, abbiamo combattuto tanto e ancora lo stiamo facendo. Abbiamo raggiunto tanti risultati e adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo tornare indietro? Dire che il provvedimento è contro le coppie omosessuali, come qualcuno nel dibattito ha detto, è pretestuoso, perché i dati statistici ci dicono che sono soprattutto le coppie etero che ricorrono a questa pratica. Dire, come ho sentito dire dall'opposizione, che con questa proposta di legge verrebbero negati i diritti dei minori, è fuorviante. Questa legge infatti nulla ha a che fare con i diritti dei minori, che sono comunque garantiti, non è mai impedito il riconoscimento riconoscimento del bambino da parte del genitore biologico e la tutela da parte di entrambi i genitori è possibile con il ricorso all'adozione in casi particolari. dire, come ho sentito dire dall'opposizione, che la maternità surrogata può avvenire per solidarietà e per altruismo è ipocrita. Questo proprio non si può sentire, perché sappiamo tutti che non è così che funziona. Intorno a tutto questo c'è mercanteggiamento e avviene sulla pelle delle donne, altro che solidarietà e altruismo. Si tratta di una reale umiliazione per la donna e per la vita che sta nascendo dentro di lei, perché entrambi durante la gravidanza stabiliscono un legame indissolubile di simbiosi e di empatia. In questa pratica, l'allattamento al seno non è previsto, quando sappiamo tutti che ha aspetti positivi innegabili sia per le mamme che per il bambino, per non parlare poi del microchimerismo fetale, per cui le cellule del feto sarebbero in grado di migrare nel sangue e nel cervello della mamma rimanendoci fino a trentott'anni dopo il parto, cosa che spiegherebbe il rapporto particolare tra madri e figli. Mi ha molto impressionato, perché è emblematico, il caso del figlio di Elton John, che, strappato dal seno materno, non ha fatto altro che piangere per ben due anni, tanto che il cantante ha deciso di far prelevare il latte dal seno della mamma biologica, una ragazza orientale che vive a 10.000 chilometri di distanza da Londra, e farlo arrivare tutti i giorni in Inghilterra con un *jet* privato per lenire la sofferenza del bambino. Per lui la storia di Gino, il pinguino birichino, non è stata sufficiente. Alla luce di tutto questo e di ciò che ruota intorno al miracolo della vita, separare una madre da un figlio, se non per cause di forza maggiore, è una barbarie che uno Stato civile non può avallare. La compravendita di bambini sin dal loro concepimento non può e non deve essere incoraggiata, perché questo sì che rappresenterebbe una regressione culturale e sociale e un ritorno a quello schiavismo in cui le donne erano costrette a vendere i propri figli per sopravvivere economicamente. È questo che vogliamo? Siamo sicuri che vogliamo questo? Combattere, scoraggiare la maternità surrogata è una battaglia di civiltà. Dietro la pratica dell'utero in affitto c'è un *business*, un mercato vero e proprio. Le agenzie che offrono servizi di maternità surrogata in Europa sono molte e il prezzo varia a seconda delle loro richieste. Anch'io ho fatto qualche ricerca per vedere un po' come funzionava: si parte addirittura dal pacchetto base per arrivare al pacchetto *vip*, senza limiti, della serie soddisfatti o rimborsati, con garanzia al 100 per cento di avere un bambino. I prezzi salgono a seconda dell'età della madre, dei donatori, dei quali si può scegliere altezza, età, peso colore dei capelli e degli occhi, gruppo sanguigno. Le agenzie mettono a disposizione dei *book* fotografici così da permettere di scegliere anche dal punto di vista estetico. Negli Stati Uniti i prezzi sono decisamente più alti che in Europa, ma arriviamo quasi a 80-160.000 euro. Sono tanti soldi ed è chiaro che solo poche coppie possono permetterselo. In India, il *business* della maternità surrogata vale circa 2,3 miliardi di dollari all'anno. Le donne "volontarie" sono reclutate sono reclutate nelle zone più povere e partoriscono più di 1.500 bambini all'anno. Molti aspiranti genitori vanno in India attratti dai prezzi bassi, che generalmente si aggirano tra i 25 e i 30.000 dollari. Le donne che entrano nel circuito legale delle cliniche per la maternità surrogata guadagnano fra gli 8 e i 9.000 9.000 dollari a gestazione. Le donne che invece non entrano nel circuito illegale vengono pagate ancora meno, tra i 3 e i 5.000 dollari e i contratti firmati ovviamente non prevedono alcun tipo di supporto medico post-parto. Una giovane donna indiana è morta all'ottavo mese di gravidanza: il neonato, che era stato commissariato da una coppia di americani, è stato salvato da un parto cesareo. L'utero in affitto costituisce un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso questa pratica, rendendoli di fatto equiparabili a delle merci e a dei prodotti ed è chiaro che dietro queste attività vi sia un vero e proprio giro d'affari che coinvolge di fatto donne povere o disagiate. Quello che però non capisco e che mi sono chiesta anche ascoltando il dibattito se siamo tutti d'accordo nel provare sdegno, nello stigmatizzare i femminicidi e gli stupri, e nel dire che è necessario un cambiamento culturale che inizi dalla scuola e che insegni il rispetto della donna e del suo corpo, e perché, se siamo tutti d'accordo nel mettere in atto quanto è possibile perché le donne maltrattate dentro casa denuncino i propri aguzzini, nonostante ne dipendano economicamente, di fronte alla pratica dell'utero in affitto, che altrettanto calpesta la dignità della donna, oltretutto mercificandone il corpo, ci sia chi è contrario a questo disegno di legge, che di fatto ha lo scopo di perseguire tale pratica, a prescindere da dove avvenga, proprio a tutela della dignità di tutte le donne del mondo. Questo io non lo comprendo: è un controsenso. Non è che, poiché la pratica della maternità surrogata avviene all'estero, possiamo chiudere un occhio. La nostra coscienza non ce lo permette. È ora di uscire da quest'ambiguità e prendere una posizione chiara, come ha fatto il Parlamento europeo, che ha definito la pratica dell'utero in affitto inaccettabile e ha ribadito che costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani; come ha fatto la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha considerato lecito il divieto dell'utero in affitto e non un limite alle aspirazioni genitoriali; come ha fatto in Spagna il Governo Sánchez, che ha inserito la maternità surrogata tra le manifestazioni di violenza contro le donne; come hanno fatto anche molti movimenti femministi, che hanno manifestato il loro profondissimo dissenso. Detto questo, signor Presidente, mi avvio alla conclusione ribadendo che ritengo questa una grande battaglia di civiltà e desidero ringraziare l'onorevole Varchi, prima firmataria del disegno di legge in titolo, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata la prima firmataria nella precedente legislatura, e la relatrice Susanna Campione, per la sua puntuale relazione. Mi auguro, anzi auguro a tutte le donne, che chi pensa di votare contro ci ripensi, esca dagli schemi ideologici e prenda una posizione netta contro questa che è una pratica barbara, barbara, che uno Stato civile non può e non deve avallare.

di considerare lo sfruttamento della maternità surrogata come un reato grave, da punire, secondo il codice penale, fino a un massimo di quindici anni. Signor Presidente, questa è anche la richiesta richiesta della Commissione europea, che nell'ultima direttiva antitratta, approvata il 17 maggio 2024, chiede proprio questo agli Stati membri, cioè di punire come reato e di inserire nel codice penale lo sfruttamento della maternità surrogata. Noi equipariamo lo sfruttamento della maternità surrogata all'induzione in schiavitù. Basta propaganda, basta parlare di reati che sappiamo non potranno mai essere considerati tali, perché sono pratiche lecite all'estero. Invece,

Vorrei segnalare a quest'Assemblea che, mentre noi siamo qui a discutere, bambini già grandicelli o grandi stanno sentendo il Parlamento del Paese del quale sono cittadini

ovviamente dai compagni di scuola che avranno ascoltato le conversazioni nelle case. Qual è l'impatto che noi, anzi,

di orfani che non sono, perché hanno l'altro genitore che è come gli altri. Non mi arrendo a un'idea zootecnica della genitorialità e rivendico la nostra umanità. Siamo animalità e razionalità, diceva qualcuno molto tempo fa. La genitorialità umana non è fatta soltanto

La norma che state disgraziatamente andando ad approvare vi impone e ci impone, come Parlamento di una Repubblica democratica che si occupa di tutti (anche dei bambini che non votano, ma che sono il nostro futuro), di assicurarci che questi bambini stiano bene e abbiano tutta la protezione, l'amore e il sostegno

come necessario. Volete prendere questa sciagurata decisione politica? Almeno passatevi una mano sulla coscienza e fate in modo che i diritti di questi bambini non siano toccati.

Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1. Sugli ordini del giorno,

parere è favorevole, se così riformulato: eliminate tutte le premesse, impegna il Governo «a garantire, nel superiore interesse del minore, un'adeguata conoscenza e una puntuale applicazione della sentenza della Cassazione, a sezioni unite, del 30 dicembre 2022, n. 38162, con la quale si individua il percorso dell'adozione in casi particolari, già presente nel nostro ordinamento e ampiamente applicato, per consentire al *partner* del genitore biologico di assumere la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore».

nei termini che ho già letto per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, che posso rileggere, eventualmente: eliminate tutte le premesse, impegna il Governo «a garantire, nel superiore interesse del minore, un'adeguata conoscenza e una puntuale applicazione della sentenza della Cassazione, a sezioni unite, del 30 dicembre 2022, n. 38162, con la quale si individua il percorso dell'adozione in casi particolari, già presente nel nostro ordinamento e ampiamente applicato, per consentire al *partner* del genitore biologico di assumere la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore».

ci sia niente da salvare in questo breve articolo, che di fatto ha la sola finalità di rimestare discriminazione, odio e stigmatizzazione nei confronti di bambini, come ho detto anche nell'intervento precedente, la cui nascita viene considerata, appunto, non soltanto un reato, ma un reato universale. È una norma che evidentemente, come pure molti colleghi hanno sottolineato questa mattina, è rivolta in particolare

come il vice ministro Sisto, ha dato parere favorevole a un ordine del giorno del senatore Gasparri secondo cui l'ufficiale dello Stato civile o l'ufficiale consolare dovrebbe chiedere alle coppie: «Scusi, com'è nato suo figlio?».

«Scusi, signora, potrei sapere com'è nato suo figlio?». E non voglio entrare nell'esame delle possibili risposte, per restare nell'ambito della decenza, però, se non dovessimo metterci a piangere, ci verrebbe da ridere. Questa è una norma che non serve a niente, perché sappiamo benissimo che sarà disapplicata e che la Corte di giustizia dell'Unione europea la troverà in violazione di una serie di norme dei Trattati istitutivi dell'Unione. Sappiamo benissimo che è irragionevole, perché introduce in modo appunto irragionevole un reato universale su un reato semi-bagatellare, punito con due anni di reclusione. È proprio una norma manifesto che serve a coprire l'inazione e l'inattività del Governo: mentre non si riesce a fare la legge di bilancio, perché mancano i soldi, si manda, tipo *panem et circenses*, qualcosa a distrarre l'attenzione, un'arma di distrazione di massa, parlando alla pancia del Paese e dicendo le cose che abbiamo sentito quest'oggi. È proprio una norma che ripugna alla coscienza civile, perché non aggiunge nulla. Io ho sentito colleghe anche dell'opposizione esprimersi in modo contrario rispetto all'idea della gestazione per altri, ma dire anche che questa norma non aggiunge assolutamente niente; ho sentito parlare di un'occasione sprecata. Insomma, mi pare di poter dire che nella sua brevità e nella sua

faccio un appello, sebbene io sappia che andrà nel vuoto come un messaggio in una bottiglia, affinché anche il resto dell'Assemblea voglia votarlo.

e lo sono anche per il dibattito a cui ho dovuto prestare attenzione questa mattina. Signor Presidente, io non sono tra quelli che, in quest'Aula e nel Paese,

coi colleghi e le colleghe - dirò semplicemente che per me un bambino non si vende, non si compra e nemmeno si regala *(Applausi)*. Oggi però non trattiamo di questo. Oggi noi non discutiamo se inserire o no nel nostro Paese una legge sulla GPA, anche se credo che i convincimenti personali, come il mio, d'altra parte, debbano prestare molta attenzione

discutiamo di che fine fanno i bambini, nati attraverso la GPA in un altro Paese dove questo è legittimo, quando i genitori vogliono rientrare in Italia Questo è il tema del dibattito di oggi. Il disegno di legge in esame è una legge contro i bambini, purtroppo una delle tante che non mettono al centro innanzitutto la persona del bambino e della bambina. Voi vi immaginate un padre e una madre o due padri e due madri che rientrano nel nostro Paese insieme al bambino e devono sborsare una cifra davvero rilevantissima, come se il reato fosse terribile, rischiando anche la galera? Che fine fanno questi bambini? Vanno negli orfanotrofi? Vengono dati in adozione ad altri? Per quanti anni - magari per tutta la vita - dovranno portarsi addosso lo stigma di essere nati in un modo diverso? Sappiamo bene che il nostro Paese non riconosce troppa benevolenza a tutto quello che è diverso. Ho ascoltato con attenzione i tanti riferimenti rispetto alla dignità della donna. Credo che parlare di dignità della donna nel nostro Paese sia molto, molto importante, in tutte le sue sfaccettature. in termini di promiscuità in un centro immigrati, con minori e bambini, anche piccoli, insieme agli adulti. Anche quella è dignità della donna e, in questo caso, di una donna bambina. Credo che quando tocchiamo questi temi, che sono etici, anche di convincimento e di sentimento personale, dovremmo avere molto più rispetto innanzitutto per i soggetti a cui sono rivolti. Noi, attraverso questa legge, inventiamo un altro reato e andiamo a punire altri bambini che avranno un percorso di vita molto, molto complicato. Tanto tempo e tanto ingegno li dovremmo invece riservare a una legge diversa sulle adozioni, che riconosca anche il diritto della persona, il diritto individuale,

la cosa peggiore che può essere fatta a un bambino sia privarlo della madre.

che vanno a incidere sulla legge n. 40 del 2004, sui quali noi, come Gruppo, voteremo dando libertà di coscienza, perché non hanno a che fare in particolare

che questa sia l'occasione di fare un ragionamento sulla legge n. 40, che è una legge ideologica. Oggi ho estremamente apprezzato l'intervento della collega senatrice a vita Cattaneo,

partorire e di lasciare il bambino nella struttura sanitaria dove lo ha partorito. Immagino che nessuno voglia togliere questo diritto alle donne. Io

dimostra. In questo caso voterò in quella direzione, rivolgendo un invito a ripensare a una legge oscurantista, che tra l'altro in gran parte è stata demolita dalla Corte costituzionale, che ne ha ravvisato gli evidenti elementi contrari ai valori di base della nostra Repubblica. Aggiungo che alcuni degli emendamenti che abbiamo votato prima si riferivano a un inasprimento delle pene quando la GPA sia dovuta a una costrizione, a utilizzare uno stato di bisogno, per esempio della donna, che in quel caso non si presta, ma viene costretta a portare avanti una gravidanza per altri. È una norma che la senatrice Castellone ha inserito nel suo disegno di legge e io nel mio, perché ci viene da dire che, se una donna viene costretta, altro che due anni di reclusione, bisogna darne venti di anni di reclusione. Vietare non è mai un buon modo; quello che bisogna fare è regolamentare. Quando c'è un abuso, se c'è un abuso, bisogna andarci giù anche con la mano pesante. Così come bisogna riconoscere - ripeto, parlo a titolo personale - che quando invece c'è una libertà e una piena autonomia

e spiegandole come funziona il mondo. Se ci sono degli abusi, se qualcuno si permette di approfittare dello stato di bisogno o della minorata volontà di una donna, bisogna equiparare questo alla riduzione in schiavitù e bene ha fatto la collega Castellone a presentare quegli emendamenti che infatti ho votato a titolo personale.

la procreazione medicalmente assistita che riguarda le donne a tutte le coppie, a quelle coniugate, a quelle conviventi, a quelli unite civilmente e alle persone *single*. Quando infatti si parla di dignità autonomia delle donne, bisogna anche poter riconoscere loro la capacità di autodeterminarsi e decidere su quello che è il proprio corpo, come avviene in tutti i Paesi europei. Poco fa senatore Malan, e mi è sembrato di sentire anche un suono di violini di sottofondo, ha detto che la cosa più importante per i bambini è la mamma, che non gli si deve togliere. Ebbene voi togliete le mamme ai bambini, perché siete voi che con i vostri provvedimenti e i vostri comportamenti avete fatto sì che venissero cancellate le mamme nelle coppie di donne. Ricordo ad esempio 33 nel Comune di Padova. *(Applausi)*. A quei bambini voi la mamma l'avete tolta. Allora diciamo che la vostra mamma non va tolta, quella astratta, teorica, che esiste soltanto nella vostra mente. Quella va rispettata, le mamme vere, reali, in carne e ossa, con i propri figli, invece, si possono anche cancellare con un tratto di penna. Invito

dico esplicitamente che il mio ragionamento non è tanto sulla questione dell'emendamento 1.15. Ho approfittato, lo dico in maniera palese, della votazione di tale emendamento per dirvi una cosa della della quale sono convinta. Io voterò contro l'istituzione di questo reato. La discussione che però ho ascoltato questa mattina

Parliamoci con grande chiarezza: istituire un reato su questa cosa è una follia per i ragazzi e i bambini che sono coinvolti. Dico però con altrettanta franchezza - e lo voglio dire esplicitamente in quest'Aula - che per me la GPA è una cosa intollerabile e lo sfruttamento di una donna su di essa non è una considerazione che non può passare dai ragionamenti che stiamo facendo. Stiamo attenti, colleghi e amici, perché c'è un tema che riguarda un errore, cioè l'istituzione di un reato nel momento in cui si dovrebbero affrontare con più serietà e articolazione certi ragionamenti. Ma ce n'è però un altro dal punto di vista di principio, che non può non passare attraverso l'idea che anche le donne che sono sottoposte a gestazione per altri (GPA) sono sfruttate. Altro che «l'utero è mio»! Quando una donna è in condizioni di sfruttamento per motivazioni sociali ed economiche, deve essere considerata in quanto tale. Lo dico perché mi sono trovata molto in imbarazzo in una discussione ideologica e voglio affermare il mio punto di vista. Con la stessa chiarezza e nettezza con la quale oggi mi esprimerò contro questo reato, vi dico anche che la posizione personale che ho sul tema della GPA è nettamente contraria e che il discorso è un po' più complesso rispetto a come sento articolare il ragionamento anche oggi in quest'Aula.

espresso in maniera molto chiara qual è l'imbarazzo del nostro partito su questa proposta di legge. Io vorrei dire una cosa però ai colleghi Capigruppo, che sono anche colleghi a cui con amicizia mi rivolgo: credo che bisognerebbe ricordarsi

tranquillità nel mio Gruppo e di confrontarmi con il mio Gruppo anche con chi ha opinioni diverse. Lei, però, ha parlato di un argomento che non è l'argomento del giorno. Siccome voi

giusto? Non abbiamo discusso, oggi, di una proposta di legge che elimina la GPA come reato. Oggi discutevamo del fatto che la GPA potesse essere estesa come reato anche quando viene praticata dai cittadini italiani che sono all'estero. Questo era l'oggetto, ma questo non l'abbiamo discusso oggi, cioè voi non avete considerato la cosa più elementare, che è il lavoro parlamentare. Noi dovremmo fare un lavoro di realtà, non un lavoro di retorica. La retorica serve a eccitare gli animi, ma governare serve a risolvere i problemi.

che questo non è il modo per scoraggiare l'elusione della legge, tutti gli esperti auditi vi hanno detto che questo è un modo sbagliato perché il vostro obiettivo è chiarissimo. Voi volete avere una maggiore deterrenza rispetto alla legge. Dico

300 chilometri di deserto, passa sei mesi in un centro di detenzione in Libia e voi pensate che possa scoraggiarlo il fatto che aumentate il tempo di detenzione da trenta a quarantacinque ma governare è un'altra cosa! Non vuol dire venire in Aula, fare un esercizio di retorica e proclamare princìpi. Vuol dire capire come si fa a evitare che si eluda la legge dello Stato, ma voi oggi non avete affrontato mai questo problema. Questo è un problema serissimo, perché allo stesso tempo la Corte costituzionale ha detto che la vera urgenza che avevamo non era quella di inventarci una norma bandiera da portare in Aula, come dire, da buttare in pasto alla retorica; alla retorica; questo non è un esercizio di parresia, non è dire la verità agli italiani. La vera cosa di cui c'era bisogno e urgenza era fare una legge sugli affidi per garantire il supremo interesse del minore. *(Applausi)*. Di quello dovevamo parlare oggi. Questo vi ha detto la Presidente quando abbiamo parlato di incostituzionalità. Perché avete continuato a sbandierare ideologie per dividere l'Assemblea inutilmente? Avete perso anche oggi un'altra occasione.

L'ordine del giorno G1.102 chiede semplicemente di introdurre, con il primo provvedimento utile, strumenti normativi volti a consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero del bambino nato da gestazione per altri, il che significa fare esattamente ciò ciò che ci chiede la Corte costituzionale, ossia rafforzare gli strumenti di tutela dei minori. Questo dovrebbe essere appunto oggetto della vostra preoccupazione e della vostra azione di Governo. Confido pertanto in un ripensamento e in un voto favorevole rispetto a questo impegno.

cerchiamo di spiegare il meglio possibile la giurisprudenza, che dice che si può ricorrere all'adozione in casi particolari. La domanda è precisamente, come pensiamo che un tribunale per i minorenni possa dare un bambino in adozione per casi particolari, quando abbiamo stabilito che i suoi genitori sono perseguibili penalmente, anche avendo commesso il reato all'estero? L'adozione in casi particolari viene uccisa da questa norma. Una delle conseguenze di questa norma sciagurata che stiamo andando ad approvare è che, come dicevo, gli atti legati alla nascita di questi bambini e quindi la loro memoria storica di chi sono e da dove vengono diventano *corpus delicti*, quindi debbono essere tolti di mezzo. Questi bambini non avranno più un pezzo di carta che dice loro da dove vengono. Del resto, vengono da un reato, da un crimine universale, quindi chi vorrebbe vedere il crimine universale dal quale viene? Evidentemente non avranno la possibilità di avere un atto del Comune che li registra, perché mica il Comune può registrare il frutto di un delitto; tra l'altro, di un delitto universale, equiparabile al genocidio, ai crimini contro l'umanità, alla riduzione in schiavitù e al terrorismo internazionale e compagnia cantante. è inutile che ci prendiamo in giro: qui bisogna che sia messo agli atti del Senato, *in secula seculorum*, che questa norma è fatta per colpire i genitori e, in particolare, quei genitori che dovranno autodenunciarsi perché non potranno tenere nascosto il fatto di aver utilizzato la GPA. L'intenzione è quindi colpire i genitori, ma le vittime collaterali saranno i bambini.

un organo della Repubblica italiana si rivolga a un privato cittadino chiedendogli spiegazioni su temi legati a come si è riprodotto. Ma ci rendiamo conto, Presidente?

riprodotto? Non sta né in cielo, né in terra. Rendiamoci conto delle cose che facciamo.

«Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.» È semplicemente la declinazione di quello che dicevo prima. Comunque questo bambino sia nato, questo bambino ha diritto a non subire pregiudizio dalla legge e che i genitori di fatto siano riconosciuti come i genitori del bambino. Qui si può votare sì o no: se si vota no, si dice che si è contrari al fatto che i bambini abbiano dei pregiudizi da questa legge. a chi ci guarda, a chi ci ascolta, di osservare bene questa votazione. Qui il testo è chiaro: non ci sono infingimenti, non ci sono possibilità di nascondersi. La proposta è chiara: si può votare sì o no. La responsabilità è nei confronti del Paese.

ci consente di svelare, di fronte a un voto contrario da parte della maggioranza, l'intento strumentale della proposta e anche ideologicamente poco umano di ciò che volete far approvare a questa Camera. Come hanno dimostrato molti interventi dei senatori e delle senatrici del Partito Democratico, noi, nonostante fossimo consapevoli alla fine siamo entrati nel merito. nonostante fossimo consapevoli di questo carattere politico, siamo entrati nel merito. Questo perché, se si entra nel merito, ci si accorge che la questione che questo disegno di legge non affronta, ma alla quale rinvia ed evoca, è una questione profonda, una questione di prospettiva, di futuro; è anche una questione di diritti fondamentali e di antropologia dalla quale muoviamo. Vi rubo pochi minuti, perché intervenire sul merito della questione che la legge dice di voler trattare, ma non tratta, è difficile. Io credo, però, che alla fine, come hanno fatto molti colleghi del mio Gruppo, non ci si deve sottrarre. Io sintetizzerei così i princìpi che dovrebbero guidare una discussione e poi una determinazione seria, responsabile da parte del Parlamento. Primo principio: non ci può essere alcuna legislazione, alcuna scelta giuridica che produce un danno ingiusto a dei bambini. È un criterio di cui non possiamo non tenere conto. Poi c'è un secondo criterio: non tutti i desideri è giusto che si trasformino in libertà o in diritti. Anche questo è un criterio. Bisogna dire, naturalmente, quali sono i desideri, che non è, a nostro avviso, giusto che si trasformino in diritti. Io ho ben chiaro che ci sono dei desideri legittimi, che però non hanno il crisma per diventare diritti, a mio avviso. Poi dobbiamo, secondo me, individuare un altro principio: che non tutti i beni è giusto che siano sottoponibili alle dinamiche del mercato. Non tutti i beni devono poter essere acquistati o venduti secondo le leggi della domanda e dell'offerta. Quindi, non ogni desiderio può diventare un diritto, non ogni bene può essere sottoposto alle regole del mercato. Non è possibile arrecare danni ai minori. Non è possibile discriminare. Aggiungo, per non

Tuttavia, come si compone questo quadro difficile di princìpi? Come si compone la tutela del bambino, il limite al desiderio, la non mercificazione di ogni bene? Alla fine, penso che il criterio guida per comporre queste esigenze sia quello di porre al centro, come questione da affrontare con serietà e con rigore,

Bisogna verificare e trovare il modo di fare sì che la donna, di fronte alle scelte che ha il diritto di compiere, di fronte alle questioni nelle quali l'ultima parola è della donna, sia davvero libera, sia davvero libera, non sia costretta dal bisogno, non sia costretta dal contesto culturale; non sia, insomma, una donna che solo apparentemente sceglie in maniera libera. Questo, secondo me, è il criterio che avrebbe dovuto condurre tutta la discussione. Allora, avrebbe potuto essere una discussione seria, una discussione che sviscerava i problemi, le contraddizioni e le ipocrisie, ma voi questa discussione non avete voluto svolgerla.

l'intento strumentale sia insito nell'emendamento, che, se venisse approvato, disconoscerebbe né più né meno tutta la norma, perché riconoscere il rapporto filiale che si è instaurato con i genitori di fatto significherebbe riconoscere la maternità surrogata. Penso che sia molto chiaro quello che noi oggi andiamo a votare. Lo dico con estrema chiarezza anche al senatore Delrio, di cui di cui apprezzo l'intervento e il tentativo, perché a proposito di contraddizioni bisognerebbe incominciare a parlare un po' delle contraddizioni che ci sono anche all'interno del suo partito, perché nel momento in cui sono contrario alla pratica dell'utero in affitto e della maternità surrogata, lo sono in Italia e per la maggior parte lo sono anche se la pratica avviene all'estero. Questo mi sembra abbastanza palese. Rispetto ad alcuni discorsi più coerente che da parte dell'opposizione arrivasse un disegno di legge per far sì che anche in Italia la pratica della maternità surrogata diventasse lecita. Sarebbe stato più coerente. Io non riesco a capire quale sia il filo del fatto che non ci avete convinto e avremmo potuto discutere di altro. È molto semplice: per evitare che la norma venga aggirata in Italia, noi dobbiamo introdurre questo reato e far sì che diventi universale. Altrimenti una coppia va all'estero, ricorre alla pratica all'estero, arriva in Italia, avviene il riconoscimento e di fatto la maternità surrogata viene riconosciuta. È talmente semplice. È talmente semplice. Comprendo naturalmente lo sforzo che è stato fatto da lei per tentare un po' di riequilibrare una posizione che immagino all'elettorato cattolico del Partito Democratico, o anche all'elettorato più femminista, sia un po' difficile da spiegare e lo apprezzo, però, ve lo dico con estrema chiarezza, non basta mettere una pezza su queste cose. Bisogna decidere se si è favorevoli o si è contrari. Non ci sono vie di mezzo e non ci sono mediazioni da questo punto di vista. Anch'io da cattolico lo dico: certi princìpi non sono assolutamente negoziabili. presidente Castellone, Il disegno di legge per chiedere che in Italia si faccia una norma per la gestazione per altri, solidale e altruistica, c'era già, l'abbiamo discussa ed è stata dalle opposizioni; una ha la mia prima firma, ma c'è anche il testo del senatore Scalfarotto e ci sono altri testi, ai quali voi avete chiuso completamente. *(Applausi)*. Invece la commercializzazione della gravidanza ma anche dei gameti è già reato. Presidente Romeo, lei neppure sa che è già reato. Stiamo parlando di un reato che già esiste e dell'estensione all'estero di un reato che, se non è considerato tale, non può essere fatta.

Basterebbe questa semplice considerazione a spiegare che è abbastanza assurdo pensare che si possa eludere la legge portando a termine la pratica della GPA all'estero. Eppure ci troviamo davanti tante mezze verità e miti da sfatare. In realtà, questo provvedimento sortisce un duplice effetto: da una parte, colma un vuoto normativo; dall'altra, non deve sfuggirci il significato ideale di questo provvedimento, che è disincentivare il ricorso alla GPA all'estero, chiarendo quello che è ovvio, ossia che farlo in Italia o fuori dall'Italia è esattamente la stessa cosa. Ho ascoltato molti interventi dei colleghi durante la discussione generale, ma non mi convincerete mai che si possa subordinare ad un contratto il legame unico, speciale e irripetibile che si crea nella gravidanza tra la madre e il nascituro. Non possiamo nasconderci che nella maggior parte dei casi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, la pratica della GPA non è solidale, ma avviene dietro compenso sfruttando la fragilità economica e sociale della madre surrogata: questo è del tutto inaccettabile e disumano. È vero che la GPA è legale in molti Paesi, ma in molti di questi Paesi è legale con pesanti restrizioni: penso all'Australia, al Canada, al Regno Unito, dove la GPA dietro compenso è sempre illegale. Quel che mi preoccupa maggiormente è il meccanismo speculativo della GPA. Mi riferisco alla pratica di coppie abbienti che, mosse dal desiderio sicuramente legittimo di avere un figlio, delegano la nascita ad una madre surrogata in un Paese povero. Mi domando: chi si preoccupa di tutelare la dignità e la volontà ultima di donne economicamente fragili? Per non parlare della tutela della loro salute durante la gravidanza. Veniamo ora al secondo mito da sfatare: la tutela dei bambini nati attraverso GPA. La trascrizione delle nascite è diventata via via più complessa nel decennio scorso; al momento per regolarizzare le adozioni di bambini nati attraverso GPA ci affidiamo a una sentenza della Corte di cassazione civile del 2019. La soluzione è quella dell'adozione in casi particolari, che consente l'adozione di minori a prescindere dallo stato di abbandono. È peraltro importante sottolineare, diversamente da quello che ho ascoltato poc'anzi, che il provvedimento in esame non avrà ovviamente valore retroattivo e, dunque, non avrà alcun impatto sui bambini nati attraverso GPA prima dell'entrata in vigore della legge, nemmeno su quelli in attesa di trascrizione della nascita. un falso mito, quello della tutela dei bambini, che fa il paio con quello della tutela dei genitori di intenzione. Qui è bene chiarire un aspetto: la genitorialità è un'aspirazione legittima, ma non possono farne le spese i diritti della madre surrogata e i diritti del neonato. La GPA è infatti una relazione complessa, che coinvolge i genitori di intenzione, la madre surrogata e il neonato. Quasi sempre il massimo delle tutele e del potere contrattuale va ai genitori di intenzione. Di potere contrattuale la madre surrogata ne ha ben poco, in quanto troppe volte è subordinata economicamente, e il neonato non ne ha affatto. Dovrebbe riflettere su questi rapporti di forza chi invoca il totem della tutela del bambino per chiudere il dibattito a favore della GPA. Una riflessione più attenta dimostra esattamente il contrario. Mi permetto infine un inciso sulla genitorialità. Non deve passare l'idea che la GPA sia l'unico modo di avere figli per coppie che non possono averne naturalmente. Esiste la procreazione medicalmente assistita, che, a differenza della GPA, è perfettamente legale in Italia. Ma non solo: la procreazione medicalmente assistita sarà inclusa nei LEA dal Sistema sanitario nazionale a partire dal 2025. Esiste poi il grande tema delle adozioni, che prima ha evocato il collega Delrio. Sono decine di migliaia in Italia i minori orfani o allontanati dai genitori in attesa di una nuova famiglia. Vero è che la pratica dell'adozione nel nostro Paese comporta tempi eccessivamente lunghi. Ma, allora, quello che il Parlamento dovrebbe prefigurarsi di fare in maniera *bipartisan* è snellire e ridurre la burocrazia e i tempi delle procedure di adozione. Da qui dovremmo partire: il Parlamento deve dare un contributo a un tema così delicato e importante, che riguarda la vita delle persone e delle famiglie. La gravidanza per altri non può essere la risposta o un modo per aggirare l'ostacolo. Mi avvio a concludere. Deve far riflettere l'ampio margine numerico con cui questo provvedimento è passato alla Camera, con numerose astensioni e persino con voti favorevoli da parte dell'opposizione. Gli ultimi sondaggi testimoniano che l'opinione pubblica è divisa, ma è divisa anche la sinistra progressista, di solito unita in difesa dei diritti. Ho molto apprezzato, nel dibattito alla Camera, l'intervento forte e sincero dell'onorevole Zanella di AVS. Divise sono anche le associazioni femministe; penso alla posizione contraria di "Se non ora, quando", penso al Convegno internazionale di Parigi del 2016 e anche alle varie sentenze della Corte costituzionale. Da ultimo ricordo che ad aprile di quest'anno il Parlamento europeo ha rivisto una direttiva del 2011: con questa revisione lo sfruttamento della maternità surrogata si inserisce nel novero dei reati che fanno capo al traffico di esseri umani. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, voterò a favore del provvedimento in esame.

Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, credo fermamente che certi provvedimenti non siano accolti con gioia. Riguardano il dolore, il dolore di chi viene ricattato per dare l'utero, la propria maternità, i propri sentimenti, le proprie affezioni potenziali. È sempre dolore, tantissimo, per chi scopre di avere i genitori in qualche modo lontani da sé, da tutti i punti di vista. Credo che solamente il piratismo di una certa sinistra permetta di dire: saremo contrari, però. Tuttavia in quel «però» c'è un mondo, c'è un universo di donne lontanissime ricattate dal bisogno, di persone irresponsabili che lucrano sia economicamente che nel potere su questi delitti, i cosiddetti crimini di pace. Presidente, lo rimando al mittente. Io sono nato due volte:

che lì ho capito che dovevo battermi per tutta la vita per quei diritti che qualcuno - anche Scalfarotto che stimo - ci nega

con gravi difficoltà di fare il medico, mi hanno sempre negato la possibilità di farlo facilmente all'università, ma ce l'ho fatta *(Applausi)*. Mi sono specializzato

a bisogni esterni. Ho sempre risposto all'etica, al diritto del bambino, sempre al centro della mia vita, ma anche al diritto della mamma e del papà. papà. Altrimenti il crimine di pace diventa qualcosa di ingovernabile, di fluido, di scivoloso e noi non ci possiamo prestare a questo. Quindi con molta determinazione, ma non con serenità, perché si parla di dolori, sempre, io dichiaro il mio voto favorevolissimo su questo provvedimento, che crea una distanza incolmabile

che si possa dire che saremo contrari, però. Questo però può uccidere l'anima della mamma lontanissima

ringraziando il presidente Meloni che indipendentemente da tutto, consapevole delle ragioni della sua scelta già nella precedente legislatura, aveva dichiarato questa realtà come come crimine universale e ha continuato a farlo. Poteva in qualche modo schivare, ma non lo ha fatto, e anzi ha aumentato la dose del suo sdegno su questa realtà.

vorrei iniziare citando la relazione a un disegno di legge presentato dalla Lega nella passata legislatura, la quale recitava che quel disegno di legge si prefiggeva di adeguare la disciplina vigente in materia di prostituzione, ne consentiva l'esercizio solo in abitazioni private, previa iscrizione nel registro tenuto dalla questura che attestasse l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. Dov'era allora la difesa della dignità delle donne, quando volevate ridurle a oggetti pronti per l'uso, quando volevate riaprire le case chiuse? Perché il presidente Romeo, allora, non rivolge la furia mostrata oggi contro il suo Gruppo? Perché non iniziare con il divieto di acquisto di prestazioni sessuali? Questa è la vostra ipocrisia. Volete non tutelare la dignità delle donne, ma colpire la loro autodeterminazione con gli stessi argomenti che un tempo usavate contro l'aborto. Qualcuno ha chiesto dove sono le femministe. Sono qua e combattono come cinquant'anni fa contro questo clima paternalistico che oggi punta la gestazione per altri e domani il diritto all'aborto. La senatrice Cattaneo ha ricordato bene che ci vuole il disvalore sociale comune per costituire un reato universale. «Cosa c'entra?»: ha urlato il collega Malan. C'entra eccome: sono i princìpi basilari del nostro ordinamento giuridico. È ridicolo prevedere un reato universale su condotte che sono lecite in gran parte dei Paesi europei, in Olanda, in Belgio, in Danimarca, nella Repubblica Ceca, in Grecia, in Portogallo, nel Regno Unito, in Ucraina, ma anche negli Stati Uniti e in Canada. Anche dal punto di vista pratico la legge non può funzionare. Come volete dimostrare che il reato sia stato commesso? In diversi ordinamenti giuridici, come in quello italiano, anche la madre può non riconoscere il figlio. Allora il padre biologico che si presenta all'anagrafe dovrà solo indicare la madre come sconosciuta e come proverete il reato? Con una rogatoria per avere dati sanitari da un Paese dove la GPA è lecita? Capite anche voi che non funzionerà. Oltre a decidere al posto delle donne, lo scopo di questa legge è quello di tenere vivi e alimentare i pregiudizi nei confronti delle famiglie arcobaleno. Avete capito che la battaglia culturale contro le unioni tra omosessuali è persa. Per questo avete spostato la vostra attenzione sul tema dei loro figli. Le coppie omosessuali non devono diventare famiglie come tutte le altre. Avete bocciato lo schema di regolamento europeo sui figli delle coppie gay e fatto una battaglia contro la registrazione delle famiglie arcobaleno nei registri comunali. Adesso volete far credere che il problema siano due uomini che vanno all'estero e si comprano un bambino di coloro che ricorre a questa pratica sono coppie eterosessuali. Sostenete che non c'è alcuna volontà di colpire i bambini, ma state dicendo a quelli che sono nati con la gestazione per altri che sono figli di un crimine universale, che i loro genitori sono peggio dei pedofili, perché qualcuno di voi ha detto anche questo: la GPA è peggio della pedofilia. Ci abbiamo messo anni ad allineare i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli dei figli nati in costanza di matrimonio, anni per dire che tra i figli non possono esserci discriminazioni. Voi, con un colpo di penna, volete portare indietro le lancette della nostra civiltà giuridica. È soltanto una norma cinica, che non ha alcun fondamento giuridico e che serve solo per alimentare un clima intimidatorio e di accerchiamento verso un pezzo della società italiana. Per voi deve esistere solo la famiglia tradizionale, un uomo e una donna, laddove la donna è tale solo se è in grado di procreare, come ha detto Bucci vostro candidato in Liguria. Se poi la donna non lavora, tanto meglio, come dimostrano i criteri per beneficiare del *bonus* Natale. Davanti a tutto questo scempio, il nostro voto sarà un convinto no.

per la modalità con la quale oggi abbiamo affrontato la discussione. Di fronte alla complessità dei fenomeni e anche all'elemento inedito che queste generazioni sono chiamate a dover affrontare in termini di regolazione e di legislazione, ci saremmo attesi un *surplus* di capacità di confronto, uno sforzo di comprensione reciproca, una possibilità di trovare nelle ragioni dell'altro un pezzo di verità per la composizione di un quadro complessivo. Signora Presidente, sui temi cosiddetti etici, nella cosiddetta Prima Repubblica, forze politiche che si erano contrapposte in maniera rilevante, profonda e significativa riuscivano sempre, anche nella distinzione di opinioni profondamente differenti, a far prevalere le ragioni dell'ascolto e il rispetto della volontà democratica. Questo Paese è stato retto per decenni da un partito di ispirazione cristiana, ma ciò non ha impedito alla Repubblica italiana di potersi dotare di una legislazione in materia di divorzio o di aborto, perché nella circostanza si realizzava e si praticava il concetto della laicità della politica. politica. Noi, vivendo un'era senza precedenti nella lunga storia umana, stiamo sostituendo allo sforzo del dibattito, del dialogo e del confronto, che è proprio della democrazia, l'esercizio del dogma, dell'ideologia, della chiusura pregiudiziale. Invece abbiamo di fronte degli appuntamenti che - mi verrebbe da dire fanno tremare le vene ai polsi. Signora Presidente, queste generazioni hanno sequenziato, per la prima volta nella lunga storia dell'umanità, l'intero genoma umano. Insomma, siamo gli architetti che possono maneggiare, per la prima volta nella storia, il DNA, e cioè un potere che fino a ieri era nelle mani della natura o di un essere trascendente, per chi ha la fede religiosa. Viviamo in un'epoca nella quale la simbiosi fra l'uomo e la macchina è in grado di generare le cosiddette *supermind,* cioè delle menti che siano capaci di svolgere compiti fisici e cognitivi a un livello superiore. Viviamo in un'epoca nella quale i confini tra vita e morte, che nell'antropologia, nella cultura, nella religione, nella storia dell'uomo erano sempre definiti con grande nettezza, sono diventati labili, perché l'introduzione della tecnologia nella nostra vita, dal suo concepimento alla sua fine, pone nuovi interrogativi etici, antropologici, culturali e quindi politici. Siamo anche in un'epoca nella quale ci sono nuove ideologie. alle ideologie transumanistiche, che immaginano che il *cocktail* fra scienza, farmacologia e tecnologia vada nella direzione di un potenziamento umano, fino al punto da superare malattie, invecchiamento, instancabilità psicofisica e produrre superintelligenza. Insomma, sullo sfondo tutte queste discussioni vi sono due questioni eterne dell'uomo che stanno entrando nelle nostre mani: l'eterna ambizione dell'uomo di rendersi immortale e l'eterna seduzione dell'uomo di sopraffare il proprio simile attraverso l'esercizio del potere. Abbiamo già visto una fase nella quale si volevano generare degli esseri umani perfetti e non è finita molto bene.

fondi d'investimento stanno lavorando sui temi della clonazione e delle piattaforme digitali tecnologiche per essere immesse all'interno di esseri viventi. Colleghi della destra, non vi dice nulla la parola Neuralink? Non vi dice nulla l'esercizio ideologico che Elon Musk sta facendo su questi temi, alla ricerca della civiltà perfetta, guidata da intelligenze potenziali artificiali e ibridate tra uomo e macchina? Insomma, stiamo vivendo un'era nella quale l'uomo rischia di essere un un oggetto e non più un soggetto. E noi come stiamo davanti a questa cesura epocale? Visto che la tematica di cui stiamo discutendo è un pezzo di questa evoluzione, noi avremmo potuto - e diciamo dovuto - esercitare la cultura del confronto, la riscoperta del limite e l'enfasi del reciproco ascolto, quella che Remo Bodei definiva la coltivazione del dubbio. dubbio. Il dubbio non è l'opposto della verità, ma è l'indice della capacità di pensare, e quindi di essere, di trovare una strada nella complessità della vita che stiamo vivendo. No, non l'avete voluto fare. Avete preferito una chiusura all'interno di uno spazio dogmatico, un pregiudizio ideologico, un rimpianto di un passato che in ogni caso non tornerà. Oggi quest'Assemblea ha scelto questa seconda strada, tradita peraltro da un esercizio muscolare che denota sempre una debolezza intima di fondo. Per questo, è un'occasione sprecata, anche perché nel merito, di cui dovremmo pur parlare ogni tanto, si è voluta sovrapporre a un'impalcatura giuridica già esistente un'inutile ostentazione di forza, portando la discussione su un terreno tutto ideologico. Lo dico in particolare ai colleghi dell'opposizione: non cadete nella trappola che oggi la destra ha voluto costruire, perché qui non si sta discutendo, anche se si vorrebbe far passare, della legge n. 40. Qui si sta discutendo di un'opzione, di una torsione, di un'imposizione panpenalistica e pretenziosa che parte dalla legge n. 40 per immaginare un'impalcatura giuridica di tipo nuovo. È per questo che noi siamo contrari, e non perché discettiamo nel merito della legge n. 40, su cui in una società, un partito o un gruppo liberale ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Sarebbe forse ora di uscire da questa idea totalitaria sulla base della quale il partito impone la linea su temi che afferiscono alla libertà individuale e al senso etico della visione della vita. *(Applausi)*. Questa impostazione ci porta a dei lidi che sono già stati battuti in passato e non è andata proprio tanto bene. Il tema, signora Presidente, è che dovremmo discutere di cosa stiamo portando oggi in esame. Come ricordato da molti colleghi, è il motivo per il quale noi voteremo contro convintamente e laicamente, perché vogliamo discutere nel merito e non perché qualcuno ci ha imposto la linea. Noi diciamo una cosa molto semplice e banale: quanto dichiarato in audizione da chi è venuto a darci la sua scienza giuridica, che ci ha detto che questa legge è inapplicabile per il principio di territorialità. Ma si è mai visto, signori sovranisti, fare una legge in una Nazione che vale per un'altra? Non si è mai visto. State superando il confine del sovranismo. Anzi, siete diventati dei globalisti. Altro che storie da questo punto di vista! poi un'altra questione che può sembrare tecnica, ma non lo è: il principio della doppia incriminazione. Stiamo definendo un principio in base al quale una persona che esercita una funzione in un altro Paese,

l'angolo. Signor Presidente, mi rivolgo ai signori della destra. Voi potevate scegliere di portare questo tema, insieme con tutti gli altri temi, sul piano dell'autorevolezza, che è qualcosa che si ottiene portando una propria posizione, ascoltando, convincendo gli altri che riconoscono la tua posizione. Avete, invece, preteso di passare dall'autorevolezza all'autoritarismo. Pretendete obbedienza incondizionata. incondizionata. Ma noi l'obbedienza incondizionata, per concetto di fondo, la vogliamo rimettere al centro di una valutazione di tipo diverso e crediamo, invece, invece, al concetto della laicità della politica a cui facevo riferimento. Rispediamo, dunque, al mittente le prediche di qualche ateo devoto, che, anche in quest'Aula, ci ha ricordato questi elementi e qualche elemento di elemento di figure zelanti, che poi, nella storia, diventano degli zeloti. Magari sarebbe interessante capire che cosa hanno fatto gli zeloti nella storia di quella religione che loro dicono di voler professare. Noi voteremo contro questo provvedimento, perché ci lascia un Paese più ingiusto, un Paese più ansioso, un Paese più cupo.

inutile, inapplicabile e con profili di forte incostituzionalità, di cui abbiamo già parlato a lungo. È l'ennesimo esempio, questo, di provvedimento manifesto, come del resto lo era stato il decreto rave, il decreto Cutro, il decreto Caivano e come fra poco sarà il disegno di legge sicurezza, con il quale questo Governo fa ancora una volta propaganda politica sulla pelle viva delle persone: in questo caso, però, dei bambini e delle bambine. provvedimenti tutti diretti a sottrarre diritti, ancora una volta, anziché estenderli; a togliere libertà, anziché aumentarla. Voi della maggioranza state trasformando questo Paese in una cittadella chiusa, arroccata, concentrata solo sulle proprie paure. Questo è quello che di fatto state facendo e dimostrando. Trasformare la GPA, che già in Italia è reato - come è stato detto più volte, ma evidentemente tocca ancora ricordarlo - in un reato universale è un abominio giuridico. Questo è chiaro a tutti, tranne a voi. Come abbiamo già detto in tanti, è pacifica l'assenza di un disvalore universalmente riconosciuto nella pratica della GPA, che è, difatti, consentita e pienamente lecita in circa 65 Nazioni, di cui sei in Europa. Europa. Non solo numerosi Paesi non vietano la GPA, ma addirittura la regolamentano, signor Presidente, e la promuovono all'interno dei propri sistemi sanitari. Viene così a cadere il presupposto fondamentale della giurisdizione universale, la presenza di un disvalore comune della condotta. È assurdo, colleghi, che questo provvedimento giunga in un momento in cui la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolineano che il nostro Paese continua a violare il diritto di figli e figlie di coppie omogenitoriali a essere riconosciuti all'anagrafe, nel rispetto del prevalente interesse del minore. Invece di concentrarsi sulle vere priorità - su questo tema sono: modificare la normativa sulle trascrizioni e, soprattutto, riformare la legge sulle adozioni, per introdurre un procedimento snello e consentire così di adottare anche ai singoli e alle coppie omogenitoriali questo Governo mette davanti a tutto l'ennesimo reato che verrà, con ogni probabilità, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, per assenza di ragionevolezza e proporzionalità e per violazione del principio di colpevolezza. Come potete guardare in faccia le persone che sono ricorse alla GPA e sostenere che debba essere reato universale una condotta che in altri Stati è perfettamente legale e regolata? Parliamo, colleghi, di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Belgio, Olanda, Portogallo e di altri Paesi ancora, cioè di democrazie consolidate. Io vi chiedo di immaginare concretamente cosa potrebbe succedere da domani ai bambini e alle bambine dopo l'approvazione di questo disegno di legge, ai cittadini italiani che magari sono all'estero da mesi sono all'estero da mesi o in questo momento rientrano in Italia con figli nati regolarmente all'estero da gestazione per altri, secondo le leggi di quel Paese e con un certificato di nascita che è un atto ufficiale. Si aprirebbe subito un procedimento giudiziario su quei genitori e, dopo un processo e una sentenza di condanna, la coppia potrebbe dovere scontare una reclusione fino a due anni e pagare una multa da 600.000 euro a 1 milione di euro, mentre il bambino o la bambina verrebbero allontanati dalla coppia. Con questa legge, quindi, esporremmo a procedimenti penali famiglie con bambini piccoli, semplicemente criminalizzando scelte procreative fatte all'estero, in Paesi dove queste pratiche sono legali e regolamentate. La verità, colleghi, è che si vogliono porre ostacoli di ogni genere alle coppie LGBT, quando invece a farne uso sono in maggioranza - lo dimostrano i dati - coppie eterosessuali, Presidente: nove coppie su dieci, secondo le statistiche. Questo disegno di legge - lo ribadisco - è un atto di smisurato disumanità verso quei genitori e quei bambini in carne ed ossa a cui voi vi ostinate a non voler riconoscere alcun diritto. Soprattutto per questo il voto dell'Alleanza Verdi e Sinistra sarà convintamente contrario.

Com'è stato più volte ricordato, la gestazione per altri è già vietata nel nostro ordinamento, in particolare dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. Con il disegno di legge in esame si sancisce invece il principio che, per quanto riguarda il cittadino italiano, la nostra giurisdizione si estende anche ai reati di maternità surrogata commessi all'estero, anche in territori dove questa pratica è consentita. Nella discussione odierna è risuonata più volte da parte dell'opposizione la questione della doppia incriminazione. Nella discussione della pregiudiziale ho parlato della violenza sessuale ai danni di un minorenne di anni quattordici per negare la necessità della doppia incriminazione, sulla quale invece hanno continuato ad insistere molti interventi dell'opposizione. Ritorno sull'argomento per chiarirlo meglio e fare un altro esempio, se vogliamo ancora più chiaro. Ho riflettuto, ad esempio, sul reato dei maltrattamenti in famiglia. In Italia questa fattispecie di reato ha un perimetro normativo piuttosto ampio e comprende comportamenti che, in altre latitudini o in altri Paesi, sono perfettamente leciti. Colleghi, consideriamo quindi un marito italiano che vive con la propria famiglia in Africa, dove commette atti di violenza e prevaricazione ai danni di moglie e figli, espressione là di potestà maritale e *ius corrigendi*. Se la coppia, dopo il soggiorno in Africa, torna in Italia, questo marito nel nostro Paese può ben essere punito dei suoi comportamenti violenti, anche se nel luogo in cui si sono realizzati erano perfettamente leciti. La deroga al principio della territorialità può aver luogo in quanto il nostro ordinamento tutela sommamente famiglie e minori. Esattamente lo stesso accadrà per la maternità surrogata quando questo disegno di legge sarà approvato. Quindi, credo che abbiamo superato il problema della doppia incriminazione. Veniamo quindi al merito del disegno di legge. Quello che mi stupisce, affrontando questo tema così delicato, è l'atteggiamento perlomeno incoerente dell'universo femminile che, in generale, non mi pare nel nostro Paese essere particolarmente sensibile, o quantomeno poco coeso rispetto ad altre problematiche. Le organizzazioni femministe, tendenzialmente di sinistra, che giustamente alzano la voce, si strappano i capelli e si indignano quando si parla di #MeToo, di sfruttamento del corpo femminile nella pornografia, condannano i compartimenti maschilisti, retaggio di un patriarcato retrogrado, oppure reclamano giustamente parità di opportunità professionali e di retribuzione fra uomo e donna, restano estremamente silenti sul commercio di neonati e sulla mercificazione della maternità che la pratica della gestazione per altri sotto sotto nascondono. Resto stupito anche di una certa titubanza della componente cattolica, che pure milita nel centrosinistra, di fronte alle problematiche poste con questo disegno di legge. Non mi si venga innanzitutto a dire che le donne che praticano la gestazione per altri lo fanno a scopo altruistico e di solidarietà umana: non ci credo, non lo ritengo plausibile, è del tutto irreale. Tutte le donne con cui mi sono confrontato, anche in previsione di questo intervento, all'interno della mia famiglia e all'interno delle amicizie, narrano di un legame profondissimo che si instaura tra gestante e nascituro nei nove mesi della gravidanza, qualcosa di misterioso e quasi soprannaturale; un legame fatto di sensazioni in comune, di odori, di palpitazioni, di sospiri, di sogni, in un rapporto simbiotico che resta indissolubile e indimenticabile per sempre. Non è naturale né normale, quindi, per una madre separarsi dal neonato subito dopo la nascita. Se lo fa - io credo - è solo per motivi economici, come lo facevano e ancora fanno purtroppo le donne - qualcuno lo ha ricordato anche nel corso del dibattito - che, per la loro che, per la loro inadeguata condizione economica o sociale, abbandonano subito dopo la nascita i figli per darli in adozione. Ma non è una libera scelta, la loro: è dettata dalle difficoltà della loro esistenza, dalla solitudine o dalla impossibilità di assicurare al figlio una vita dignitosa. Non mi si venga a dire che una donna istruita, benestante, affermata professionalmente, si presterebbe mai a portare in grembo per nove mesi un figlio per poi cederlo per mera simpatia umana a un'altra coppia, abbandonandolo per sempre. Quelle che si prestano a queste pratiche sono invece donne tendenzialmente povere, scarsamente istruite, di basso livello sociale, che vengono sfruttate e utilizzate come incubatrici dalle coppie ricche e viziate provenienti dal nostro Occidente opulento e decadente. Non vedo come si possa, quindi, negare che la gestazione per altri sia una pratica degradante che umilia la donna nella parte più bella e intima del suo essere, quella di creatrice e donatrice di una nuova vita. In diversi interventi di stamane sono state ricordate le pratiche aberranti cui accettano di sottoporsi le presunte volontarie, che stipulano, in cambio di somme di danaro, autentici contratti capestro anche in Paesi teoricamente civili. Sono Paesi che definisco teoricamente civili e avanzati, ma nei quali, in una sorta di darwinismo sociale, la tutela dei deboli e fragili è pressoché assente. Su questo non sono tanto diversi da quelli del Terzo mondo. Cosa poi dire del neonato? Qualcuno si chiede come potrà un nato attraverso la GPA mai accettare, raggiunta l'età della ragione, di essere stato oggetto di una transazione economica, anche se mascherata da rimborso spese? L'esperienza insegna che pressoché tutti i figli adottivi, spesso con profondo strazio della coppia dei genitori adottivi, vanno alla ricerca della madre e del padre naturali; talvolta abbandonano addirittura il contesto sociale dove sono stati cresciuti e ritornano nella patria di origine, subendo un misterioso ma insopprimibile richiamo della foresta. Un figlio o una figlia generati con la maternità surrogata vengono, quindi, privati della loro umanità più profonda e del diritto di conoscere i genitori biologici e naturali. Negli interventi di oggi si è sostenuto, infine, che la norma che stiamo per votare avrebbe per obiettivo penalizzare ingiustamente i bambini già nati: nulla di più falso. Intanto va precisato che, essendo norma penale, non ha effetti retroattivi e, quindi, non potrà mai incidere sullo stato di fatto ad oggi maturato. La norma, semmai, vuole evitare, nei limiti del possibile ovviamente, che donne deboli e fragili siano indotte, per motivi economici, a mettere al mondo bambini destinati a un turpe commercio e a contrastare il cosiddetto turismo riproduttivo, volto a eludere la nostra legislazione. Mi consenta, signor Presidente, una notazione finale su un intervento, quello della senatrice Pirro, che mi ha davvero creato turbamento. In questa delicatissima materia non è possibile gridare: l'utero è mio e faccio quello che voglio io. L'ovulo non è paragonabile a un rene o a un'unghia. L'ovulo femminile è una *spes vitae*. L'ovulo contiene in potenza un essere umano unico e irripetibile, titolare esso stesso di diritti; non se ne può fare quello che ci pare, e mi sorprende che una donna ne abbia così poca considerazione. Per tutti questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente il testo oggi all'esame dell'Aula. *(M5S)*. Signor Presidente, il Paese non ha bisogno di questa legge, che noi chiaramente non voteremo. Anzi, questa legge rappresenterà grave problema per alcuni cittadini di questo Paese, che oggi sono già discriminati. Cari colleghi, in questi due anni ormai ci avete abituati alla moltiplicazione e all'estensione dei reati; in due anni avete introdotto 15 nuovi reati, dal reato di *rave* al reato di invasione di terreni, al reato di stesa, al reato di rivolta in istituto penitenziario, al reato di detenzione degli orsi bruni marsicani. Oggi parliamo dell'estensione di un reato, partendo dal dato di fatto che la commercializzazione della gravidanza e la commercializzazione dei gameti in Italia è già reato, punito appunto dalla legge n. 40 del 2004. Vorrei provare a sgomberare un po' il campo dalla propaganda che è andata in scena questo pomeriggio, perché, vedete, la stessa collega Mennuni ci chiedeva di chiamare le cose con i termini giusti. Ebbene, il termine giusto non è utero in affitto, perché qui non si affitta proprio nulla. nulla. Quando c'è un affitto, si prevede anche un canone di affitto. Ma che costo, che prezzo si può mai dare a un dono che non ha valore, il dono di una vita? Non ci può essere alcun affitto e se c'è commercializzazione, come ho detto, è già reato. Ma, a mio avviso, è anche sbagliato parlare di maternità surrogata. Qui si parla di gestazione surrogata, di gravidanza surrogata. Forse non l'avete notato, ma la gravidanza e la maternità sono due cose separate e sono separate anche grazie alla legge n. 194 del 1978. E a chi, anche in opposizione, ha provato a dire che c'è un legame tra madre e feto, io dico: attenzione a non mettere in discussione questa separazione, che è stata sancita nel 1978. Oggi una donna in Italia, se gravida, può scegliere il parto in anonimato e non tenere il figlio può scegliere l'aborto. Questa libertà la difendo e la difendiamo, anche per tutte quelle donne che magari si sentono madri già nel momento in cui scoprono di essere incinte e non fanno neppure l'amniocentesi, perché sarebbero madri anche madri anche di un figlio con una malformazione. *(Applausi)*. È proprio la libertà che ti dà la consapevolezza della scelta di essere madre, perché la maternità è soprattutto una scelta. La maternità è un modo di stare al mondo, non è uno stato biologico. La maternità è cura, è guida, è accoglienza; la maternità è un dono e anche la gestazione solidale e altruistica è un dono. Se è gratuita, è un dono, il dono più grande che una donna possa fare ad un'altra donna o ad una coppia che non può concepire in modo biologico, perché magari la donna è nata senza utero, perché magari per un tumore ha subìto l'asportazione dell'utero. Se mia sorella, una mia amica o una persona a cui voglio bene mi avesse chiesto di aiutarla a diventare madre, io l'avrei fatto. La gestazione per altri, solidale e altruistica, è una pratica lecita. Infatti questa vostra legge non ha alcun senso, perché non risponde ai prerequisiti per prevedere che un reato possa essere universale. L'abbiamo detto in tanti: un reato, per essere universale, deve avere una doppia incriminazione, cioè deve essere reato sia nel nostro Paese che nel Paese in cui è stato commesso. Quindi non può essere reato universale una pratica che altrove è lecita. Un'altra caratteristica di un reato universale è la rilevante gravità

con una detenzione massima che va da sei mesi a due anni? Sapete voi stessi che non può essere un reato grave. Sono d'accordo però con voi su un punto Paese serve una legge che regolamenti la gestazione per altri solidale e altruistica, proprio per evitare ed arginare gli illeciti

senso. Colleghi, prima della legge n. 194 del 1978 l'aborto già esisteva. Le donne abortivano, ma lo facevano clandestinamente e abortendo perdevano la vita. Oggi la gestazione per altri solidale esiste e le coppie italiane fanno ricorso a quella pratica e non possiamo far finta che non esista. Sono sicura, Presidente, che quando, tra qualche anno, ripenseremo alla discussione di oggi in quest'Aula ci sembrerà surreale, così come oggi

E allora, quando ci occupiamo di temi che hanno una rilevanza etica così importante, noi davvero dovremmo lasciare fuori la propaganda e farci guidare di più dalla società che invece sui temi etici è tanto più avanti della politica. Dovremmo altresì farci guidare dagli esempi virtuosi di altri Paesi che hanno avuto il coraggio di legiferare su quella materia. Questo è quello che noi abbiamo provato a fare con il mio Gruppo parlamentare perché abbiamo studiato e approfondito le legislazioni degli altri Paesi sulla materia, cercando di prendere tutti gli esempi virtuosi e depositando una legge

una proposta di legge. Di essa io riprenderò solo alcuni punti. Il primo punto importante è riconoscere che la gestazione per altri solidale e altruistica è un dono. È il dono più grande che si possa fare e proprio perché è un dono che non può essere in alcun modo obbligatorio né commisurato con un valore, noi abbiamo previsto sempre la revoca del consenso da parte della gestante. proprio perché crediamo che il rischio alla rinuncia del consenso sia commisurato alla grandezza del dono. Un altro punto importante è la modifica che chiediamo di introdurre agli articoli 600 e 601 penale, in cui si tratta il reato di riduzione in schiavitù, chiedendo che quando c'è sfruttamento e gestazione per altri sotto sfruttamento, allora si parli di riduzione in schiavitù, il che riprende

tante tutele per la gestante. Per esempio la previsione che il materiale genetico non deve essere della gestante, che quindi non è la madre biologica, che deve avere dei figli viventi, e altre tutele per la coppia. la coppia. Presidente, in conclusione, quando trattiamo temi etici, anziché utilizzare la propaganda, dovremmo provare ad immedesimarci nelle storie e nelle vite di quelle persone che le vivono. Oggi in Italia ci sono 200 bambini nati da gestazione per altri e io vi invito ad ascoltare le storie di quei bambini e di quelle famiglie. A chi diceva che sta tutelando il diritto delle donne, io, da donna, vi dico che noi donne non abbiamo bisogno che ci tuteliate solo dal punto di vista riproduttivo. Noi donne vorremmo essere tutelate quando una donna su cinque entro i due anni di vita del figlio deve lasciare il lavoro perché non riesce a conciliare gli impegni lavorativi e gli impegni familiari. *(Applausi)*. Una donna vorrebbe essere tutelata quando in una posizione dirigenziale le viene sempre preferito un collega maschio che sicuramente ha più tempo da dedicare al lavoro. Una donna vuole essere tutelata in altro modo, Presidente. Invece, se proprio volete occuparvi di reati universali, occupatevi dei crimini di guerra e di condannare i criminali di guerra, quelli sì che sono reati universali E smettetela di fare propaganda sulla pelle delle persone e sulla pelle di bambini che sono nati da un atto di amore - perché sono sempre storie di amore - bambini che hanno il diritto di vivere nelle loro famiglie, qualunque tipo di famiglie esse siano.

cercando poi di ottenere, aggirando la legge, il riconoscimento giuridico e anagrafico del nascituro. Questa è una legge che va in questa direzione e in modo molto semplice diciamo che siamo d'accordo. Naturalmente, quando parliamo di maternità surrogata, stiamo parlando del consenso di una donna estranea al rapporto di coppia a mettere a disposizione il proprio utero per portare avanti la gravidanza altrui. Ne usufruiscono lo dico perché non vi è alcuna discriminazione, come è stato ricordato bene nella discussione generale dal collega Malan - in prevalenza delle coppie eterosessuali e poi anche delle coppie omosessuali, ma non vi è alcuna discriminazione: per noi qualsiasi sia la coppia ricorre a questa pratica, questa pratica deve essere giustamente considerata un reato. *(Applausi)*. Non ci sono forme di discriminazione di alcuna natura. Questo sembra quasi un pretesto tante volte evocato per cercare di fermare una legge e sarebbe più coerente dire che non si è d'accordo con la legge e questo sarebbe meglio per tutti. L'approvvigionamento, tra l'altro, di gameti e il reclutamento di donne sono gestiti da agenzie internazionali, che forniscono addirittura dei servizi legali e l'organizzazione dei viaggi. Pensate a cosa siamo di fronte, sicuramente a un gran *business*, su questo non c'è alcun dubbio. Non è altro che una forma di sfruttamento del corpo della donna, che porta ad una vera e propria compravendita di bambini e di bambine che vengono in tal modo trasformati in beni di consumo e in oggetti, il tutto per soddisfare i desideri di genitorialità di chi è pronto ad offrire, per soddisfare un proprio desiderio, ingenti somme di denaro a donne perlopiù finanziariamente e socialmente vulnerabili e quindi più facili da persuadere a prestare il proprio utero. Lo dico a lei, presidente Centinaio, naturalmente rivolgendomi alla vice presidente Castellone, che questa storia della maternità surrogata solidaristica e fatta con amore è la più grande ipocrisia che io abbia mai sentito in tutta la mia storia politica. chi ricorre a questa pratica perché lo fa e qual è l'obiettivo che vuole assolutamente raggiungere. Non è infatti un caso che i mercati di gravidanza surrogata più economici si trovino proprio nei Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con un basso livello di riconoscimento dei rischi e dei diritti. Come ho detto stamattina, si tratta di ricchi committenti che, per soddisfare un proprio desiderio, pagano donne povere, facendosi prestare l'utero e sfruttando il loro corpo. Questo è fondamentalmente la maternità surrogata, né più né meno, detto in modo molto semplice, senza star lì a girarci intorno. Si dimentica, così, che i figli non sono un diritto, ma sono un dono. Se crediamo davvero che sia giusto combattere tutte le forme di discriminazione, a maggior ragione dobbiamo fare in modo che nessun bambino venga discriminato, né possa essere comprato da ricchi committenti e che nessuna donna venga lesa nella sua dignità. Nella maternità surrogata la donna diviene strumento riproduttivo utile a soddisfare i desideri degli altri; è un attacco alla dignità umana, con l'essere umano trattato alla stregua di un oggetto, come ha ricordato anche di recente Papa Francesco.

e si evoca il diritto del fanciullo ad essere riconosciuto, però ci si dimentica della dignità della donna che viene lesa; poi altre volte, quando fa comodo, ci si ricorda del diritto di autodeterminazione e della libertà della donna di disporre del proprio corpo, dimenticando il diritto del bambino di conoscere le proprie origini, la propria identità biologica e storica e la propria madre.

che non sono disponibili per persone diverse da lui. La madre non può disporre del diritto dei figli. Questo è il punto che bisognerebbe mettere in evidenza. Così come i desideri dell'uomo non possono prevalere sui diritti di soggetti differenti. Non siamo molto lontani dal poterla definire la schiavitù del terzo millennio, impropriamente spacciata per progresso. Per questo motivo pensiamo sia doveroso considerarla un reato grave, da perseguire con adeguate sanzioni, anche a livello internazionale, proprio come avviene per la tratta e lo sfruttamento sessuale. Lo diciamo con chiarezza. Noi della Lega avremmo preferito che tale norma rientrasse nel codice penale per strutturare meglio e per dare maggior forza al reato ed è per questo che in Commissione abbiamo presentato degli emendamenti migliorativi. ci è stato detto che così facendo rischiavamo di perdere tempo, perché poi il provvedimento sarebbe dovuto tornare alla Camera e quindi, giustamente, per velocizzare e dare forza alla nostra iniziativa, abbiamo detto che andava bene, tanto ci saranno altre occasioni per poter

c'è il caso che l'inesperto e il dilettante (che è anche peggiore) di filosofia si metta a proclamare che il diritto consiste unicamente nel far tutti quanti il comodo proprio.

perché Marx si rivolterebbe nella tomba: dalla dittatura del proletariato alla dittatura del politicamente corretto e quindi del grande capitale. Oddio, capitalisti travestiti da comunisti. Non potete, dovete assolutamente smentire questa cosa, altrimenti non ci sarebbero davvero più dubbi e sarebbe davvero duro - e lo capisco - giustificare politicamente le vostre azioni. Ci saremmo aspettati un altro tipo di discussione, un altro tipo di intervento, pronto sì a contrastare la pratica dell'utero in affitto, magari proponendo soluzioni differenti; invece, da quello che abbiamo capito da certi interventi, magari non da tutta la sinistra, addirittura c'è qualcuno che la ritiene una pratica solidaristica. Noi no. Siamo favorevoli al disegno di legge. *(Applausi)*.

spesso con toni che, francamente, sono abbastanza mortificanti, perché quando si parla di questioni così delicate e difficili, che coinvolgono desideri e speranze che attengono alla concezione dell'uomo e della donna e della maternità, che producono anche divisioni e forti passioni, forse ci vorrebbe più serietà e meno tifo da stadio, come quello che abbiamo visto questa mattina in quest'Aula. quest'Aula. Nel nostro partito ci sono posizioni diverse sul tema della maternità surrogata e della gestazione per altri. Io, per esempio, sono tra coloro che condividono le parole che ha espresso al riguardo la Corte costituzionale, quando ha ricordato

se non indifferenza che avete nei confronti della tutela dei bambini e del corretto bilanciamento tra il divieto di maternità surrogata e la tutela dei bambini. In audizione abbiamo ascoltato tanti giuristi

un'opinione, ossia che questa legge che pretende di punire chi ha avuto un figlio con la gestazione per altri, anche quando la condotta sia stata tenuta in un Paese diverso dal nostro dove essa è consentita e lecita, è giuridicamente insostenibile. Questo ci hanno detto tutti i giuristi, anche quelli contrari. Ricordo, in particolare, la dottoressa Gabriella Luccioli, Presidente di sezione della Corte di cassazione, che per trent'anni si è occupata di questi temi

Anzitutto occorre sapere, perché forse non è stato ricordato adeguatamente, che la maternità surrogata in Italia è già reato ed è già punibile anche quando eseguita all'estero. Ripeto: è già punibile oggi. Non c'è bisogno di questa legge, perché si applica quella norma del codice penale che consente la perseguibilità di reati commessi all'estero a una condizione, ossia che il Ministero della giustizia chieda che si proceda. Questa disposizione, che subordina la procedibilità a una richiesta del Ministero della giustizia, ha una sua *ratio* e una sua stringente logica giuridica e politica, perché la regola che informa i rapporti di cooperazione e relazioni internazionali tra gli Stati (e soprattutto tra Stati democratici di tradizione e ispirazione liberale come il nostro) è quella della doppia incriminazione. Quella è la regola che informa i rapporti, per cui un reato commesso da un cittadino all'estero può essere perseguito se la condotta è considerata reato anche in quel Paese. Se invece la condotta in quel Paese è considerata lecita, come nel caso della maternità surrogata, che è regolamentata in molti Paesi civili e democratici, per procedere è bene che vi sia una valutazione politica che spetta al Ministero della giustizia, poiché una perseguibilità assoluta rischia di minare i rapporti con quei Paesi, all'insegna - e questo è il vero punto - di un paternalismo di Stato che trasforma l'Italia in giudice etico universale della moralità dei propri cittadini, in contrasto con i principi del liberalismo politico. *(Applausi)*. Questo è il punto: la vostra concezione del diritto penale. È proprio quello che accade con l'introduzione di questa norma. Non a caso, infatti, nonostante sia già perseguibile oggi a legislazione vigente, non risulta che mai una volta il Ministero della giustizia abbia esercitato tale facoltà, che pure è riconosciuta dalla legge italiana. Cosa succederà quando questa nuova norma si applicherà a condotte tenute in Stati dell'Unione europea dove la maternità surrogata è stata legalizzata? Come si concilierà la punizione dei cittadini italiani con i principi che informano l'Unione (la libera circolazione delle persone, l'uniformità di trattamento, la tutela dei diritti fondamentali)? Come si applicherà la norma a persone che hanno la doppia cittadinanza: italiana e, poniamo, di un altro Paese in cui invece è lecita, ad esempio il Canada? Cosa si farà in caso Ancora, è vero che il legislatore penale, in via del tutto eccezionale, può prevedere di punire in ogni caso, vale a dire a prescindere da una richiesta del Ministero della giustizia, reati commessi dai cittadini italiani ovunque essi siano compiuti, ma si tratta, in quei casi, di reati di particolare disvalore sociale, vale a dire di crimini contro l'umanità, rispetto ai quali il principio di universalità esprime la solidarietà internazionale tra gli Stati in favore di casi riconosciuti ovunque di interesse comune: come il genocidio, la pirateria, il terrorismo o gravissimi reati contro lo Stato. Non si tratta certo di reati come quello inerente la maternità surrogata, che è sproporzionatamente meno grave, tanto è vero che è punito con una pena bagatellare fino a due anni di reclusione e non è universalmente riconosciuto, considerata in particolare proprio l'eterogeneità delle regolamentazioni giuridiche di Stati di diritto e di democrazie liberali. Insomma, sul piano giuridico si tratta di una forzatura e dell'ennesima torsione del diritto penale, che molto ha a che fare con l'ideologia e poco o nulla con i principi liberali del diritto e con i buoni rapporti di relazione e cooperazione tra Stati democratici. Ma vi è di più e di peggio, perché voi ve ne infischiate dell'equilibrio che ci deve essere tra la punizione della maternità surrogata e la tutela dei diritti dei bambini, che sono i veri soggetti vulnerabili, indifesi e deboli, che vanno tutelati. Quando la Corte costituzionale ha definito la maternità surrogata una pratica che offende in modo intollerabile la dignità delle donne, non ha chiesto al legislatore di trasformare la condotta in reato universale per perseguire i cittadini italiani in tutto il globo terracqueo, come piace dire alla vostra Premier. La ha chiesto invece al legislatore qualcosa d'altro. Ha chiesto di occuparsi e di prendersi cura dei veri soggetti deboli e dimenticati di questa vicenda, i bambini, coloro che sono venuti al mondo grazie a queste tecniche e la cui tutela deve prevalere su ogni altra considerazione, su ogni esigenza di punizione, su ogni ideologia, su ogni strumentalizzazione. Questo è quello che ha chiesto la Corte, ricordando che il pieno riconoscimento del diritto di quei bambini è, in particolare, quello di essere accuditi fin dalla nascita dalle persone che possono meglio assicurare loro la cura; è il riconoscimento di quel legame di filiazione che li lega alle persone che, non solo hanno voluto la loro nascita, ma che concretamente esercitano la responsabilità genitoriale. Oggi quel diritto non è adeguatamente garantito. Questo ha detto la Corte, ma di tutto questo nel provvedimento al nostro esame non c'è traccia, perché, accecati dal vostro furore ideologico, ci si è dimenticati dei diritti degli ultimi, dei più deboli e indifesi. I bambini non solo sono stati completamente dimenticati da questa legge, ma addirittura rischiano di essere pregiudicati da un'applicazione rigorosa di sanzioni a carico dei genitori, ai quali dovesse essere riconosciuta la responsabilità genitoriale nel superiore interesse del minore. È questo il punto. Rischiano di essere pregiudicati i diritti dei bambini, lungi dall'essere riconosciuti. Per questo noi abbiamo votato a favore di tutti gli emendamenti e ordini del giorno che, anziché inseguire il paternalismo ideologico della destra, puntavano a dare migliori e più saldi diritti ai minori. Con questa legge, quindi, noi riteniamo si faccia un grave errore. A noi interessava ed interessa, a prescindere dalle soluzioni, dare un segnale chiaro: che in gioco qui ci sono, prima di ogni altra cosa, i diritti dei minori; che con quei diritti non si gioca per motivi ideologici e politici; che un legislatore attento, empatico e compassionevole di quelli dovrebbe occuparsi, non di altro. Con questa legge si va in una direzione diversa e opposta. Per noi è l'ennesima brutta pagina della politica; è l'ennesimo brutto capitolo della storia di questa legislatura e per questo il Partito Democratico voterà contro. signori del Governo, colleghi senatori, oggi concludiamo il percorso di un provvedimento normativo che non nasce oggi, ma nasce nella vecchia legislatura, e la prima firma di questo disegno di legge è di Giorgia Meloni. Coroniamo, in questo percorso e in questo giorno, una battaglia che non finisce sicuramente qui, ma che è l'inizio di un grande cammino che restituisce la dignità e la difesa delle donne, la dignità e la difesa dei bambini e la custodia dello stesso senso dell'umanità. Sono emozionata e anche orgogliosa di intervenire in dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. Ringrazio l'onorevole Carolina Varchi, che è la prima firmataria di questo disegno di legge nell'attuale legislatura. Ovviamente i ringraziamenti vanno alle due Commissioni di competenza che hanno lavorato e alla relatrice Susanna Campione che ha ha svolto un grande lavoro *(Applausi)*. C'è stato un grande dibattito nei due rami del Parlamento, ma anche nel Paese, e questo succede quando i provvedimenti toccano la carne viva delle persone. Ognuno ha portato la propria visione e la propria discussione, ma credo che oggi sia stato fatto un passo importante ed un avanzamento sul piano dei diritti e della dignità dell'essere umano. Proprio rispetto a questo dibattito, vorrei fare una prima semplice considerazione: la narrazione che è stata fatta in questi giorni e in questi mesi, soprattutto dalle opposizioni, alcune volte con affermazioni lontanissime dalla realtà, non aiuta il cittadino che vuole seguire da casa il dibattito parlamentare. La maternità surrogata, o gestazione d'appoggio, o gestazione per altri (GPA) non è una pratica solidale. Si tratta di una particolare tecnica che ha bisogno comunque di un contratto, ha bisogno delle regole, ha bisogno di una fecondazione *in vitro* e quindi, alla nascita di questo bambino, la consegna dello stesso alla coppia o al singolo che lo hanno commissionato. Quindi, per facilitare tutto ciò, in questo contratto si cancella qualsiasi tipo di legame tra la donna surrogata e il bambino stesso. L'ovocita è quello di un'altra donna: c'è una fecondazione assistita, c'è la cosiddetta donatrice che viene scelta sul catalogo. Lo abbiamo già detto stamattina: si possono scegliere tutte le caratteristiche legate alla genetica, all'aspetto fisico, alle caratteristiche anche intellettive. È un vero contratto commerciale. Quindi, i protagonisti sono la donatrice, la madre surrogata, l'uomo che fornisce lo sperma, la coppia, il singolo committente, i professionisti, gli avvocati, i medici e addirittura le banche di biomedica: questo è l'utero in affitto, checché se ne dica. Stiamo parlando in realtà di esseri umani e quindi non di un'automobile, non di un jeans e neanche di un accessorio che completa l'*outfit* per una serata. È una pratica obbrobriosa. Si parla di commercializzazione dei corpi delle persone. Com'è stato detto, in Italia il reato era già riconosciuto dalla legge n. 40 del 2004. In realtà lo estendiamo a tutti quegli italiani che negli anni - e in tanti anni - hanno favorito il turismo procreativo. In Italia abbiamo già sentito anche alcuni esponenti della minoranza dei quali apprezzo gli interventi che sono stati differenti rispetto a quelli del loro partito. Alcune giurisprudenze importanti hanno usato parole durissime verso la surroga. La stessa Corte di cassazione parla di maternità surrogata che offende in modo indelebile la dignità delle donne e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando di fatto la mercificazione delle donne *(Applausi)*, e sistematicamente di donne che vivono in condizioni economiche disagiate. Quindi, si va all'estero, si commissiona un bambino e si porta in Italia, raggirando la legge. Fratelli d'Italia ha voluto portare avanti con coerenza e determinazione questo impegno e oggi diciamo basta a qualsiasi tipo di utero in affitto. In Italia è vietato l'utero in affitto in qualsiasi forma Oggi, come donna e come madre, esprimo grande soddisfazione, perché le donne e i bambini non sono merce di scambio perché le donne povere non si sfruttano e soprattutto perché la genitorialità non è un contratto commerciale. Da donna impegnata nelle istituzioni sono altrettanto soddisfatta, perché in realtà stiamo dando un quadro certo di diritto che consente l'efficacia di una legge dello Stato. Stiamo rispondendo soprattutto ai sindaci coraggiosi, perché ce ne sono quei sindaci che, attenendosi alla legge, in questi anni non hanno trascritto gli atti prodotti all'estero. Io sono tra quelli. Ci si è trincerati dietro un dibattito pubblico per mesi, però vi do una notizia, cari colleghi della minoranza: a nessun bambino è stato negato il diritto dall'ordinamento italiano. Gli unici diritti a rischio sono quelli calpestati quando, piuttosto che parlare di bambini, parliamo di bambini come merce di scambio *(Applausi)*, di articoli e di oggetti da prendere su un catalogo.

Presidente, la delicatezza di questo argomento non è un alibi per non affrontare lo stesso. Noi lo abbiamo affrontato con tutta la necessaria determinazione. Oggi finalmente in quest'Aula si scrive una bellissima pagina di storia. A Fratelli d'Italia non interessa l'ideologia e allora vogliamo ribadire con forza che la maternità non ha nulla a che vedere con questa pratica disumana commerciale. Non possiamo avallare con azioni e anche con omissioni questa nuova forma di schiavitù della donna. Non vogliamo che siano avallate e comunque cancellate varie battaglie femministe. Sono infatti curiosa di vedere poi, al momento concreto, come voteranno le tante femministe che sono sedute dall'altra parte dell'Aula. Ho apprezzato l'intervento della senatrice Valente, che stimo soprattutto per l'onestà intellettuale rispetto a quello che ha detto sulla GPA, perché le battaglie personali non possono essere cancellate dal contenitore politico al quale si appartiene, e quindi l'onestà intellettuale va premiata, come quella di altri colleghi che sono intervenuti a questo riguardo.

perché ha rappresentato le istanze di tutto questo Gruppo politico prima ancora della dichiarazione di voto da me svolta. Nelle pregiudiziali, le frasi che ho ascoltato dai colleghi di opposizione sono state le seguenti: è un provvedimento bandiera; è un provvedimento incostituzionale; è un furore ideologico, un rigurgito di omofobia; legge sbagliata, violenta, demenziale; fiera dell'ipocrisia, ha detto una mia collega. Il collega Verini chiede addirittura la resa ad una visione della società colorata. Io mi rifiuto. *(Applausi)*. Il collega Scalfarotto poi, dopo un intervento alquanto importante che ha fatto ieri rispetto alla mia collega che era intervenuta, ha paragonato tutti i parlamentari che sono seduti da questa parte dell'Aula e soprattutto gli italiani ad un gregge, perché ha detto testualmente

ci vorrebbe una giornata per replicare a questa giornata importante di interventi. Ovviamente non commento sulla confusione espressa in maniera teatrale e plateale, a cui ci ha abituato la senatrice Pirro, perché ha confuso l'utero con il bambino. È curioso quando, nel secondo intervento, ha detto che le donne devono essere libere di poter lasciare il bambino: un bambino non si deve lasciare e non si deve abbandonare;

avete perso un'occasione. Capisco l'imbarazzo di chi magari non la pensa come il partito di appartenenza su certi temi etici, come questo. ripetere in quest'Aula e ormai sono due anni che ci sentiamo dire, soprattutto da esponenti del PD, che abbiamo perso un'occasione, quando in realtà in due anni abbiamo approvato numerosi provvedimenti nell'interesse dei cittadini, mi dispiace dirlo, non lo comprendo. Ci spieghi il PD perché, quando ha governato pur non vincendo le elezioni da anni e decenni, non ha mai disciplinato materie importanti come questa. Gli italiani ci hanno eletto per fare le norme, per scrivere le norme; fatevene una ragione. Questa è una norma necessaria, a tutela della dignità della donna, dei diritti dei bambini, delle origini e delle identità. Questo Governo a guida Meloni e questa maggioranza parlamentare di centrodestra continueranno a lavorare con coerenza e a dare risposte sugli impegni presi in campagna elettorale. Nel dichiarare il voto convinto e favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ribadisco e sottolineo l'impegno che ci siamo presi con gli italiani: lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani. Lasciamo ai progressisti e al segretario del PD, paladina delle battaglie creative, le passerelle, i microfoni e i riflettori dei palcoscenici musicali. Fratelli d'Italia con questo provvedimento recupera un *vulnus* normativo e dice no alla violenza sulle donne non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni dell'anno. Viva le donne e il loro ruolo centrale, come ribadito da più parti e dal nostro Papa. Viva i bambini e il loro diritto, che è prioritario, ad avere una madre e un padre.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 163, 245 e 475.

con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024*** La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica di quattro atti internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Si tratta di strumenti normativi che finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile 2023. A seguito di quell'appuntamento internazionale nel febbraio 2014 l'Italia ha sottoscritto questa serie di intese con la BERS e l'Ucraina allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga Nova Kakhovka sul fiume Dnipro nell'oblast meridionale di Kherson, a partire dalla realizzazione di un progetto di cooperazione a favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono rispettivamente un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Nello specifico, gli accordi in via di ratifica definiscono i termini di un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del fondo rotativo per la cooperazione e lo sviluppo gestito da Cassa depositi e prestiti, tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, dal valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità addizionali di fondi provenienti direttamente dalla BERS. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

supporto militare e politico, ma di occuparsi anche in prospettiva della ricostruzione. La presenza della comunità internazionale accanto all'Ucraina deve concretizzarsi deve concretizzarsi anche in un sostegno economico ed infrastrutturale che sia anche di medio e di lungo periodo. L'accordo al nostro esame facilita questa possibilità strategica e per tale ragione voteremo a favore della ratifica.

il richiamo a un impegno straordinario perché si riescano a portare le parti al tavolo per trovare una soluzione condivisa in quella zona martoriata dell'Europa. Presidente, con il suo permesso, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia a tutti e tre i disegni di legge di ratifica in oggetto, il n. 1228 perché certamente contribuirà ad aumentare l'interscambio commerciale tra Italia ed Egitto, n. 1229 perché contribuirà ad aumentare il partenariato economico tra Italia - e quindi Europa - e Ghana e ci auguriamo per l'intera regione dell'Africa occidentale, e il n. 1230 che ratifica quattro accordi tra Italia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Ucraina e per ricostruire e ripristinare le centrali idroelettriche ucraine che purtroppo, nel frattempo, sono state danneggiate dall'azione di un conflitto insensato. Bene ha spiegato la relatrice, quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia senza intervenire ulteriormente.

Il 14 ottobre a Milano si è svolto un convegno in cui erano presenti anche il sindaco di Mykolaiv e alcune nostre aziende che stanno già collaborando in in sede di progettualità per la ricostruzione di quella città. Credo che sia doveroso aiutarli in termini economici e sostenerli quanto più possibile per quel che riguarda la popolazione civile,

segnale di una proficua e attenta politica estera sia in termini di sviluppo, sia in termini di difesa del nostro Paese. Per quanto riguarda questa specifica ratifica tra l'Italia e la Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione dell'Ucraina, evidentemente qui il ripristino di alcune centrali idroelettriche è assolutamente importante per iniziare quel percorso di ricostruzione. Dichiariamo pertanto il nostro voto favorevole, augurandoci anche che questo possa essere d'auspicio per una fine veloce del conflitto.

perché dà il segno - ne parlavamo ieri anche alla presenza della Presidente del Consiglio - di come noi non diciamo abbastanza di quanto stiamo facendo per aiutare, dal punto di vista economico e della ricostruzione delle infrastrutture strategiche, l'Ucraina, perché tutto il dibattito, anche mediatico, è sempre ed esclusivamente sugli aiuti militari, che rappresentano certamente una parte importante, ma meno del 50 per cento degli aiuti e del sostegno che noi diamo al popolo ucraino e al Governo dell'Ucraina. È per questo che mi permetto di spendere qualche parola in più per sottolineare l'importanza del lavoro che abbiamo fatto. Non era scontato: rischiavamo di perdere queste risorse e abbiamo dovuto accelerare. Ringrazio anche la Presidente della 3a Commissione, perché abbiamo lavorato insieme, a tappe forzate, per arrivare velocemente ad approvare questo, che è un accordo anche innovativo

un accordo sia con la banca che con il Governo ucraino, ma anche di mettere in contatto le società che partecipano, in particolare la principale società idroelettrica ucraina. Questo

della brutale aggressione russa, che nel 2023 ha colpito la diga nella regione di Kherson che rifornisce di acqua tutta quell'area, creando un disastro naturale davvero imponente. Il fatto è che

che ospiterà la conferenza sulla ricostruzione. Mi son preso qualche minuto in più per sottolineare come l'Italia aiuti e sostenga prevalentemente con aiuti economici e di ricostruzione delle infrastrutture energetiche, ma purtroppo questo è un tema molto poco sottolineato. Oggi facciamo dunque un passo in avanti rispetto al lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi e penso possa essere sottolineato, non solo da noi, non solo da quest'Assemblea, ma anche da chi segue e ci ascolta, quindi da parte dei *media* e dei giornali italiani.

effettivo di solidarietà all'Ucraina: quando ci si schiera moralmente, politicamente e geopoliticamente, ci sono tanti fatti che seguono. *Acta non verba*, si diceva un tempo in latino. un segno effettivo e, se ci pensate, i quattro accordi che oggi ratifichiamo nascono direttamente da quella conferenza che volle il Governo nel febbraio 2024, a due anni dall'invasione russa

accordo si indica la strada della ricostruzione e del ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, ma tutto questo serve a consolidare e a finalizzare un impegno assunto dal nostro Paese.

che lo stesso schema può essere la base di future collaborazioni nella definizione del cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse. Penso per esempio al Piano Mattei e a quello che l'Italia, non soltanto con le parole,

e, un domani, anche collaborando con il Continente a noi vicino.

Il testo prevede l'istituzione di un'agenzia trinazionale dotata di personalità giuridica, operante nell'alveo di un'organizzazione internazionale, GCAP per l'appunto, deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di cosiddetta sesta generazione,

Italia, Regno Unito e Svezia, ma che diventa Italia, Regno Unito e Giappone (ed anche questa è una proiezione europacifica), e può essere, tra l'altro, aperta all'inclusione e alla partecipazione di ulteriori Paesi. L'organizzazione istituisce un'agenzia che avrà sede in Inghilterra, nella città di Reading. Il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea era stato inizialmente curato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un *memorandum* del 2020

della realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione. Cosa significa? È un sistema integrato con sistemi cooperanti non pilotati, con satelliti e altri assetti militari. Sono tutti elementi collegati tra di loro da una rete intelligente che è basata su un'architettura *cloud*, cioè nuvola, dedicata di intelligenza artificiale, di *data link* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli di sesta generazione sono destinati a sostituire gli attuali, cioè gli Eurofighter, a partire dal 2035. La vita operativa prevista sarà estesa fino alle ultime decadi del secolo in corso. Molti di noi, quindi, non li vedranno finire. Le aziende capofila sono Leonardo - ovviamente -, la britannica Bae Systems e la giapponese Mitsubishi. Per l'Italia si prevede, tra l'altro, la partecipazione di altre aziende di livello internazionale. Pensiamo, per esempio, a MBDA Italia, Elettronica e Avio, oltre a ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese. Proprio perché la cosa ha una certa importanza cerco di non essere così veloce come accade di solito con questo tipo di ratifiche. La relazione illustrativa, che invito a leggere, sottolinea come il programma abbia l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* del settore di cui parlavo, anche centri di ricerca e università, puntando alla realizzazione di un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive in ambito industriale e accademico. Il GCAP si prevede possa realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *knowhow*.

andranno a concordare i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione e supporto logistico), che comunque non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto nelle linee di finanziamento dedicate di cui al decreto di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento dello Stato maggiore della difesa n. 36 del 2021, a cui si fa riferimento. Su questo volevo dire che l'atto di Governo recante lo schema di decreto ministeriale a cui ho fatto cenno è relativo allo sviluppo di un'architettura complessa e interoperabile,

ed è stato approvato ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)* del codice dell'ordinamento militare. La Commissione difesa del Senato esaminò il provvedimento già nell'autunno del 2021, formulando, il 20 dicembre del 2021, un parere favorevole.

la sede sarà in Inghilterra, ma ci sarà una parametrazione, una equilibratura proprio negli organi dirigenziali, che quindi sistemerà ed equilibrerà la partecipazione di tutti i Paesi. si stabilisce che, alla eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Il testo, come è ovvio, non presenta profili di incompatibilità con la normativa pertanto, il Senato tutto ad approvare questo che, strategicamente, verso il futuro del nostro Paese, tanto in termini di difesa quanto in termini di partecipazione e di copartecipazione con gli alleati, risulta fondamentale per i prossimi decenni.

l'occasione è significativa per porre all'attenzione dell'Assemblea e del Governo, oltre che della Presidenza, una riflessione che parte dalla condivisione, almeno per quel che riguarda il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, di questo percorso, che il relatore ha bene illustrato, ma che pone un elemento che stride in maniera significativa con l'attualità. Signor Presidente, noi stiamo approvando un disegno di legge che istituisce un'organizzazione internazionale per finalità di difesa, di sicurezza, di tutela del nostro ordinamento. Questo percorso ha seguito una linea retta molto puntuale, molto precisa, molto corretta dal punto di vista delle relazioni e dal punto di vista dell'autorizzazione parlamentare. È una Convenzione fra Stati che è stata sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 fra Italia, Giappone e Regno Unito. L'ambasciatore del Giappone è intervenuto in audizione in Parlamento e ha spiegato le questioni e le motivazioni che il relatore ha ricordato e oggi il Parlamento è chiamato a dover ratificare. Perfetto. Mentre noi seguiamo questo percorso fra Stati sovrani, siamo costretti a dover leggere sui *media* e sui giornali che non meglio precisati che non meglio precisati livelli istituzionali del nostro Paese starebbero chiudendo degli accordi di carattere militare e di sicurezza con un soggetto privato per il trasferimento di dati del nostro apparato di sicurezza e del nostro esercito su un *device* privato che si chiama Starlink, che è di proprietà del signor Elon Musk. Allora, ne approfitto per porre al Governo, alla Presidenza e all'Assemblea una semplice riflessione: com'è che nelle relazioni tra Stati il Parlamento è giustamente centrale e nel momento in cui qualcuno decide, non so dove, negli Stati maggiori, alla Farnesina o alla Presidenza del Consiglio di potersi avvalere di una struttura privata, che peraltro non è neppure soggetta alla giurisdizione delle nostre strutture nazionali, tutto questo noi lo si debba apprendere aprendo un giornale? Ne approfitto pertanto per chiedere che, su quello che sta avvenendo nei rapporti fra il Governo e la struttura di Starlink, con particolare riferimento al tema dell'impiego dei satelliti con finalità di sicurezza e militari, ci sia la necessaria attività di coinvolgimento preventivo del Parlamento, da cui arrivi poi una valutazione successiva. Non scodellateci qui cose già fatte, perché noi non staremo a ratificare in maniera silente questioni di sicurezza nazionale. Signor Presidente, noi stiamo discutendo di recepire una ratifica che, come diceva il senatore Alfieri, forse meriterebbe una discussione un po' approfondita sul tema.

delle spese militari e qui siamo di fronte a una spesa molto rilevante. È chiaro che oggi si costituisce l'Agenzia, però c'è un valore dietro di circa 9 miliardi.

Noi abbiamo sempre pensato e detto che, anziché sviluppare ogni Paese la propria strategia, se vogliamo costruire, ad esempio, un'Europa che conti nel mondo, non basta farlo dal punto di vista commerciale, ma andrebbe fatta una cessione, in particolare sul terreno della difesa. Ogni Stato fa da sé, tant'è che c'è un altro progetto, diverso da questo fatto dall'Italia con la Gran Bretagna e con il Giappone: ce n'è uno fatto dalla Francia e dalla Germania. È dimostrabile, andando avanti così, che l'Europa non conterà mai nulla sulla scena internazionale, se ogni Stato pensa di andare in questa direzione. Se l'Italia pensa addirittura di mettersi con Paesi che sono usciti dall'Unione europea, mi pare anche questo un segnale non accettabile. Infine, alcuni articoli che sono usciti pongono il problema vero: noi stiamo parlando di costruire le future armi, perché dovremo difendere la democrazia dall'attacco della Cina in particolare, ma anche di altre aree emergenti del mondo. Ora, se noi pensiamo,

se noi pensiamo che la democrazia si difenda coi cacciabombardieri di sesta generazione, credo che non faremo un buon servizio alle nuove generazioni.

qualche dubbio dovrebbe venire a ognuno di noi.

ed è previsto un esborso economico di oltre 9 miliardi. Questo programma è il proseguimento di un *memorandum* del 2021 in cui gli attori principali di allora erano Svezia, Italia, Gran Bretagna e Giappone. In seguito, la Svezia si è sfilata dal programma ed è rimasto in piedi solo l'accordo tra Giappone, Gran Bretagna e Italia. Dal punto di vista tecnico, non c'è nulla da dire, anzi direi che secondo me il Governo ha proseguito nei giusti modi; non ha effettuato gli errori che, secondo me, sono stati effettuati durante la progettazione e gli accordi sugli F-35. Mi spiego. Andiamo a creare una agenzia intergovernativa che si occuperà dall'inizio alla fine, quindi dalla progettazione alla messa in opera e all'industrializzazione di tutto quel che riguarda la costruzione di questo velivolo di sesta generazione, ossia un velivolo tecnologicamente più avanzato degli F-35. C'è stato un *iter* che io condivido pienamente. Questa agenzia servirà per controllare tutto ed è costituita in parti egualitarie e paritarie dai tre Stati citati; non ci sono *partner* di diverso livello, come invece fu per l'F-35. Dove sta la problematica? La problematica, secondo me, sta nel fatto che non siamo più in ambito europeo. Il senatore Magni prima ha citato un programma che Francia e Germania parrebbe stiano progettando

Ricordo a tutti noi che anche il rapporto Draghi indica nel comparto difesa quello su cui investire massicciamente al fine di garantire appunto la nostra difesa. L'Italia cosa sta facendo? Concludendo un accordo con Giappone e Gran Bretagna, che non sono ovviamente nell'Unione europea, temo che debba finanziare

alle porte, vicinissime e meno vicine. Credo che possa anche essere utile pensare, da qui ai prossimi ottant'anni, di andare a sostituire quello che è tutto il nostro comparto aereo. Ma, in questo momento in cui il ministro Giorgetti chiede sacrifici a tutti e chiede a tutti i Ministeri un taglio del 5 per cento

per quanto sia anche condivisibile l'obiettivo, sembra che ci stiamo andando ad infilare in un problema più grosso di quello che cerchiamo di risolvere. la seguente: io so benissimo che questo programma è aperto anche agli altri Stati europei che in futuro vorranno parteciparvi, ma è stato tastato il terreno di quanti Stati europei vogliano, possano e abbiano la necessità di partecipare al programma, al fine che anche le nostre industrie e quindi i nostri lavoratori partecipino al finanziamento che ovviamente l'Unione europea darà per i programmi del comparto difesa? Io credo che ci stiamo andando a isolare e a sopportare un costo che in questo momento non ci possiamo permettere, un costo di denari che per il popolo italiano sarebbe meglio - secondo me e secondo noi - andare a distribuire per difendere le parti sociali più deboli, per investire in sanità, scuola e formazione. Credo che forse fermarsi un attimo per ragionare e temporeggiare su questo programma sia dovuto. Per questo annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. Signor Presidente, sono in totale disaccordo con quanto ha detto il collega precedente e ritengo invece che questa, più che una ratifica internazionale, sia un vero e proprio accordo accordo strategico con altri Paesi alleati e amici, come lo sono il Regno Unito e il Giappone. Il GCAP rappresenta, per il nostro Paese, un'opportunità

Voglio anche sottolineare come questo programma permetta all'Italia di rafforzare le relazioni internazionali. Questo non è più un programma europeo, ma è un programma globale, tra l'altro fatto con attori che sono in un'area del globo, l'Indo-Pacifico, sempre più strategica nel contesto geopolitico internazionale. Per i motivi che ho elencato, il nostro Gruppo voterà favorevolmente.

Signor Presidente, dicevo prima che non è una ratifica banale, ma è una ratifica che va specificata nel suo oggetto. Qui non stiamo parlando del programma in sé, che è stato già approvato, e poi tornerò a dire quando lo è stato e da chi è stato proposto. Noi oggi ratifichiamo l'istituzione di un'organizzazione internazionale che dovrà definire sede, comitato direttivo, responsabilità, guarentigie e privilegi dei funzionari e di chi ci lavorerà al suo interno per ragioni di sicurezza. Quindi, ci stiamo occupando di tutt'altro. miliardi, ma poi è sempre molto difficile andare a definire l'impatto, dal punto di vista economico-finanziario, di un progetto così rilevante. Sono tutte cose che sono state definite in un altro provvedimento. Oggi parliamo di altro e, quindi, faccio fatica a capire le ragioni di votare contro la definizione e la ratifica di un'organizzazione internazionale che tutela le persone che stanno all'interno. Però ognuno fa le sue scelte, evidentemente. Su quello oggi votiamo. È poi anche l'occasione, giustamente, di parlare in Aula di questo progetto. È un progetto che vede la nascita nel 2019, certamente in ritardo - come diceva il collega senatore Magni - rispetto al progetto franco-tedesco,

progetto. Se noi vogliamo investire sull'autonomia strategica - ed è bene che l'asse franco-tedesco lo capisca, essendoci un tema di convergenza che dovremo affrontare - il primo passaggio è cercare di diventare autonomi dagli Stati Uniti. È evidente che il progetto F35 è interamente basato su tecnologia e su investimenti prevalentemente del nostro principale *partner* dal punto di vista della sicurezza, e cioè gli Stati Uniti. Per quello noi abbiamo iniziato a investire su vari settori, su vari dispositivi, su vari sistemi d'arma, a geometria variabile. Noi dovremo andare in prospettiva a costruire un sistema unico. un sistema unico. Siamo dentro una dimensione diversa rispetto al passato e questo non è l'aereo del passato, della quarta generazione di Eurofighter, che noi dovremo andare a sostituire. Noi oggi parliamo più correttamente di una piattaforma aerea di sesta generazione, non è l'aereo in sé, meccanico, costruito come era in passato. Contano molto di più e incidono nei costi gli investimenti nell'elettronica, nei satelliti e nei sensori. La parte elettronica conta oggi molto di più dell'investimento sull'aereo in sé e ha ricadute enormi sul settore civile. Tanto che, per fare tutto questo, si è creato un laboratorio scientifico in Italia

Certamente noi dovremo lavorare per una convergenza maggiore dei sistemi d'arma a livello europeo e costruire la difesa europea. tecnologicamente sul nostro sistema, rimarremo sempre dipendenti dagli Stati Uniti e quell'idea di autonomia strategica e di difesa europea rimarrà un'ipotesi velleitaria.

altresì investire in difesa. Il benaltrismo non mi convince. Noi dobbiamo investire nella difesa, trovare più soldi, investendo anche sulla difesa europea se vogliamo giocare un ruolo nel mondo e non piangere lacrime di coccodrillo quando ci ritiriamo dall'Afghanistan o in Medio Oriente non siamo capaci di investire fino in fondo il nostro capitale politico a livello europeo. Serve parlare il linguaggio della verità. Facciamo questo dibattito, portiamolo nelle Aule parlamentari e parliamo in maniera seria dei temi della difesa. Se diventa tutto dibattito ideologico, non faremo mai un passo in avanti in questo Paese.

credo che oggi stiamo scrivendo una pagina di storia sia per la nostra industria aerospaziale sia per il futuro della nostra Aeronautica militare, con l'approvazione di questo provvedimento,

alla Seconda guerra mondiale, quella con i motori sulle ali. Oggi andiamo, con questo GCAP Tempest, di fatto a tentare di realizzare per il 2035 un aereo che ci porterà fino alla fine del secolo; un aereo dotato appunto dei collegamenti con la rete, di intelligenza artificiale, che quindi possa essere avanguardia tecnologica rispetto a quella di chissà chi altro. Credo che tutto questo non possa che essere oggettivamente guardato in maniera positiva da tutto l'arco parlamentare. Dopodiché oggi, soprattutto nelle dichiarazioni di voto, ho sentito alcuni interventi rispetto ai quali - il Presidente mi permetterà - vorrei fare alcune sottolineature. Il senatore Enrico Borghi ha tirato fuori dai cassetti voci che non c'entrano nulla con questo provvedimento; articoli di giornale che, onestamente, mi sembravano completamente fuori luogo e decontestualizzati rispetto al testo che stiamo analizzando. Posso riconoscere coerenza al senatore Magni rispetto alle posizioni politiche che la sua forza politica ha preso in passato; posizioni che non ho mai condiviso e che condivido ancora meno oggi rispetto allo scenario internazionale. Ma una cosa non mi convince, e cioè andare ad analizzare gli Stati *partner* rispetto a una collocazione non c'entra assolutamente nulla rispetto alla collocazione geopolitica dell'Italia del futuro, perché qui stiamo parlando di un piano industriale per costruire aerei tecnologicamente avanzati di sesta generazione. Al netto del fatto che stiamo parlando di due Paesi occidentali, onestamente non si capisce perché questo non si possa fare con coloro i quali mettono a disposizione risorse e investimenti. di investimenti, senatore Marton, è dimostrato che ogni euro investito in difesa produce ricchezza complessiva e, quindi, posti di lavoro, entrate fiscali, quindi la capacità di aiutare il bilancio dello Stato più che in qualsiasi altro settore venga investito. Lo dimostra la storia; lo dimostrano le tecnologie che abbiamo in tasca; lo dimostra il futuro di tutti quei progetti che nascono in ambito difesa e che poi ci troviamo nella vita di tutti i giorni. Anche la demagogia spicciola che ho sentito nel suo intervento, e che - mi permetta - non è da

nella *governance* di questo progetto la Svezia con il Giappone a modificare l'impianto. Credo che, nell'impianto complessivo, questa sostituzione sia oggettivamente residuale rispetto alla portata del progetto. Vedremo come si svilupperà. Senatore Alfieri, va benissimo approfondire questi temi anche in Commissione; nulla osta, per quanto mi riguarda, anche verificare con affare assegnato come avanzeranno queste cose per andare verso quel progetto e quella visione che il Presidente del Consiglio ha affermato più volte con forza, ovvero far sì che l'Europa, pur in un quadro occidentale, pur nell'ambito delle forze della NATO, possa avere una propria gamba europea e, nel momento del bisogno, possa non essere del bisogno, possa non essere dipendente dall'Alleanza occidentale, ma avere più autonomia decisionale quantomeno per i territori che ci circondano. Per tutti questi motivi evidentemente il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del provvedimento.

in realtà il titolo denuncia già il contenuto del provvedimento. Vorrei solo aggiungere che il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale di riferimento per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi mediterranei, mediante il trasferimento via mare di soli veicoli rimorchiati, contribuendo così

non vengono rispettati e l'Egitto è uno di quelli. Per noi la ferita di Giulio Regeni è ancora sanguinante e per questa ragione ci asterremo.

vengono presi in carico da altre motrici. Ciò risponde a un'esigenza degli operatori, perché si evitano costi di assicurazione e controversie

i rimorchi ognuno nel proprio Paese, c'è un tema di minore impatto sulle assicurazioni e di minore inquinamento da parte dei veicoli egiziani. Si tratta, quindi, solo di un accordo tecnico fatto dai rispettivi Ministeri e, pertanto, il voto del Gruppo

tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016. L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale complesso e piuttosto lungo, oltre a essere finalizzato a porre le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano, attraverso la progressiva rimozione di barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, punta a garantire al Ghana un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazioni economiche e commerciali complessive dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica complessivamente in poco meno di 14.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, 2025, essenzialmente ascrivibili a spese di missione. In conclusione, si propone, non essendoci contrarietà rispetto a obblighi internazionali, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

vorrei ricordare in quest'Aula Mariella Gramaglia, morta dieci anni fa, il 15 ottobre. È stata una femminista, giornalista, scrittrice, parlamentare negli anni Novanta nella Sinistra Indipendente, assessore alle pari opportunità del Comune di Roma nella Giunta Veltroni. È stata anche docente presso la facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo. Nata ad Ivrea, ha studiato a Torino. Venne a Roma, dove scoprì il femminismo come lei scrisse - quando i cuori delle donne hanno cominciato a cantare, solo quando ne avevano voglia loro. Il suo ultimo libro, «Fra me e te», scritto con la figlia, è un dialogo epistolare tra una madre e una figlia sui diritti delle donne, le cose conquistate, le cose che non andavano negli anni in cui c'era il movimento Se non ora, quando? Di Mariella Gramaglia il primo ricordo che ho è dopo Chernobyl, in un intervento in un seminario bellissimo, «Scienza, potere, coscienza del limite». Io ero una ragazza ci consegnò allora la parola cura. «Sulla scorta del vocabolario - disse - ho verificato che la parola Cura ha un duplice significato che ben si attaglia al nostro problema: da un lato vuol dire "angoscia e ansia", dall'altro, pensiero attento e costante. Da un lato dunque rappresenta un'emozione, per l'altro, lo sforzo concreto intelligente di governare l'emozione stessa.». Mariella Gramaglia è stata una visionaria. È stata una persona che arrivava prima. Oggi della parola cura abbiamo fatto sapere e riflessioni. È stata un assessore attentissimo alle persone. È suo il numero 060606, che è un servizio del Comune di Roma semplice, che dà risposte a tutti i cittadini. Lei diceva che, per essere un amministratore, ci vogliono soprattutto costanza e attenzione. Mariella voleva che si rispondesse a ogni *mail* o lettera - era la responsabile della comunicazione - possibilmente telefonando. Era un modo coerente con la sua idea della politica, il suo modo di abitare il mondo. una donna curiosa e coinvolta dalle vicissitudini delle umani genti, un'attenta tessitrice di relazione e connessioni: un modo di essere che tanto servirebbe oggi a questa politica così urlata.

come parte integrante dei nostri valori democratici. Marco Borella, un apicoltore comasco, ha avuto l'ardire di esporre, sul suo banchetto autorizzato, in un'area mercatale, una semplice scritta: «Stop bombe a Gaza. Stop genocidio». È un messaggio di pace, un appello alla riflessione su una situazione di conflitto che sta lacerando vite e famiglie lontane, ma che ci tocca profondamente nel cuore. Eppure, invece di ricevere cori di approvazione o semplicemente un confronto rispettoso, è stato punito con una multa di 430 euro per violazione dei commi 1 e 11 dell'articolo 23 del codice della strada. La scritta "Stop bombe a Gaza. Stop genocidio" sul banchetto di Marco Borella arrecherebbe disturbo visivo agli utenti della strada, distraendo l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione in un'area mercatale. È evidente che dietro questo intervento ci sia una volontà di reprimere chi ha il coraggio di esprimere il proprio pensiero, di sottrarre il nostro discorso pubblico a quei temi scomodi che richiamano la nostra coscienza. Ciò che è accaduto a Desio è non un'esazione burocratica, ma un abuso di potere, un attacco alla libertà di espressione, un gesto che mina le fondamenta della nostra democrazia. Un messaggio contro le bombe può davvero essere considerato un problema? La risposta è un secco no: fino a che punto siamo disposti, quindi, a tollerare la repressione del dissenso in nome di un presunto ordine pubblico? Tutti noi dovremmo prendere una netta posizione contro atti di questo genere, che manifestano non solo una mancanza di sensibilità nei confronti di questi temi urgenti, ma anche una scarsa comprensione del valore della libertà di espressione. In conclusione, voglio chiamare tutti noi a difendere il diritto di espressione per le proprie opinioni, anche quelle scomode. Chiamo quindi tutti noi a riflettere sull'importanza di una società in cui i messaggi di pace non vengano puniti, ma accolti e discussi, perché la vera forza di una democrazia si misura nel rispetto della diversità di pensiero. La vicenda però ha avuto un lieto fine in qualche modo, perché poco fa si è conclusa con un provvedimento in autotutela dei Carabinieri di Desio che hanno annullato la multa. La democrazia diventa più forte accogliendo il dissenso e la diversità di pensiero. *(Applausi)*.